L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato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

In considerazione del ruolo centrale che le riforme occupano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del regolamento dell'Unione europea n. 241 del 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo ritiene che in questa occasione il PNRR possa integrare il PNR. Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, il DEF espone il quadro relativo all'anno 2020 e le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni fino al 2024. Con riferimento al 2020, richiamando le stime ufficiali dell'Istat, il DEF evidenzia come il PIL abbia registrato una caduta pari all'8,9 per cento in termini reali, una contrazione dell'attività economica senza precedenti in tempi di pace. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica e delle riforme della politica di bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche prospettate all'interno del PNRR, che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2021 e adottate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio in data 31 marzo 2021. La previsione di crescita tendenziale del PIL in termini reali per il 2021

è prevista pari al 4,5 per cento nel 2021, 4,8 nel 2022, 2,6 nel 2023 e 1,8 nel 2024. Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, i dati riferiti al 2020 attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a 156,9 miliardi, corrispondenti al 9,5 per cento del PIL, inferiore al livello del 10,8 per cento previsto dalla NADEF. Lo scostamento rispetto alle precedenti stime è attribuibile prevalentemente alla revisione del saldo primario per circa 20 miliardi; vi concorre inoltre la nuova stima della spesa per interessi per circa un miliardo. A sua volta, la revisione del saldo primario è dovuta in parte a un miglioramento delle entrate per 3,6 miliardi e in misura prevalente a un miglioramento delle spese per 16,4 miliardi rispetto alle precedenti previsioni. Per quanto attiene al quadro previsionale a legislazione vigente, quindi tendenziale, il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2021 un indebitamento netto pari al 9,5 per cento del PIL (circa 165 miliardi). Rispetto al 2020, nel 2021 il saldo rimane costante in termini di PIL: a un peggioramento del saldo primario (meno 0,2 per cento) corrisponde un analogo miglioramento della spesa per interessi (più 0,2 Per gli anni successivi si stima un decremento dell'indebitamento netto rispetto al 2021 sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL, con riduzioni costanti in ciascun esercizio: meno 100 miliardi nel 2022, meno 69,6 miliardi Per quanto riguarda il quadro programmatico di finanza pubblica, si segnala in particolare che esso tiene conto del prossimo decreto di sostegno all'economia che utilizzerà il nuovo scostamento di 40 miliardi nel 2021, 6 miliardi nel 2022,

quindi, espansiva nel prossimo biennio tramite un forte impulso agli investimenti per poi intraprendere un graduale percorso di consolidamento fiscale - dal 2024 in poi - a condizione che le ipotesi sull'evoluzione dell'epidemia e sulle condizioni di contesto internazionale dello scenario di base restino valide. Per quanto riguarda l'evoluzione del rapporto debito pubblico-PIL, la stima preliminare per il 2020 indica un livello del 155,8 per cento inferiore al livello del 158 per cento previsto nella NADEF 2020 e dal documento programmatico di bilancio 2021. Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con un andamento dei saldi di cassa migliore delle attese. Il fabbisogno del settore pubblico a fine 2020 si è attestato infatti al 9,5 per cento del PIL anziché all'11,8 per cento atteso a settembre 2020. Un ulteriore contributo è stato fornito dalla revisione in lieve rialzo della previsione del PIL nominale. Per quanto riguarda le determinanti della variazione del rapporto debito-PIL, Il DEF evidenzia innanzi tutto come, per l'operare per l'operare congiunto di fattori ciclici e discrezionali, sia venuto meno nel 2020 l'effetto positivo dell'avanzo primario in presenza di un peggioramento dell'indebitamento netto di otto punti percentuali. Quindi, alle previsioni per effetto del perdurare delle ripercussioni economiche della crisi da Covid-19, il rapporto debito-PIL non subirà l'inversione di tendenza prefigurata nella NADEF 2020, che prevedeva per il 2021 un valore pari al 155,6 per del PIL - ma invece aumenta fino al 159,8 per cento nel 2021. Il quadro tendenziale aggiornato è infatti peggiore rispetto a quello della NADEF 2020 a causa sia dello scostamento di bilancio richiesto lo scorso gennaio per finanziare il decreto-legge cosiddetto "sostegni", sia della nuova richiesta di scostamento annessa a questo DEF. Per quanto riguarda gli anni successivi dell'orizzonte di previsione fino al 2024, l'inversione di tendenza del rapporto debito/PIL inizia già a partire dal 2022, con un obiettivo programmatico pari al 156,3 per cento da ottenere grazie al calo del fabbisogno del settore pubblico (-6,8 punti percentuali rispetto al 2021) e alla maggiore crescita del PIL nominale Il rapporto è previsto in ulteriore calo nel 2023 (155 per cento) e nel 2024 (152,7 per cento) principalmente grazie ad una riduzione del disavanzo primario e di un miglioramento della crescita del PIL nominale.

Quindi, alle previsioni per effetto del perdurare delle ripercussioni economiche della crisi da Covid-19, il rapporto debito-PIL non subirà l'inversione di tendenza prefigurata nella NADEF 2020, essendo stimato in aumento fino al 159,8 per cento nel 2021. Il quadro tendenziale aggiornato è infatti peggiore rispetto a quello della NADEF 2020 a causa sia dello scostamento di bilancio richiesto lo scorso gennaio per finanziare il decreto-legge cosiddetto sostegni, sia della nuova richiesta di scostamento annesso a questo DEF.

probabilmente se non si legge con grande attenzione quello che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha scritto,

Unitamente al Documento di economia e finanza, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del Piano di rientro verso l'Obiettivo di bilancio di medio termine, denominato OMT, ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid. La relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, la cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio, il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. Il Governo evidenzia preliminarmente che per l'anno in corso la Commissione europea ha deciso l'applicazione della cosiddetta *general* *escape clause*, che assicura una temporanea sospensione delle regole di bilancio per assicurare agli Stati membri un maggior spazio di manovra al fine di sostenere le spese sanitarie necessarie ad affrontare la pandemia e a contrastare gli effetti recessivi della crisi pandemica. Questa relazione segue una serie di analoghe relazioni presentate nel corso degli anni 2020 e 2021, con le quali il Governo ha richiesto alle Camere l'autorizzazione a reperire risorse attraverso un maggiore indebitamento netto per fronteggiare la crisi pandemica. In particolare, con le autorizzazioni approvate a marzo, aprile, luglio e novembre dello scorso anno, il Parlamento ha consentito il ricorso a un maggiore indebitamento pari a circa 108,3 miliardi di euro per l'anno 2020, 32,4 miliardi per il 2021,

A ciò va aggiunta l'ulteriore autorizzazione approvata in occasione dell'esame della Nota di aggiornamento al DEF 2020, da cui deriva un maggior *deficit* pari a circa 25 miliardi per il 2021, 12 miliardi di euro per l'anno 2022 e lo scorso gennaio, su richiesta del Governo, il Parlamento ha autorizzato un ulteriore scostamento di bilancio pari a 32 miliardi di euro per l'anno 2021. Queste risorse sono state impegnate nel bilancio delle pubbliche amministrazioni per finanziare una serie di misure contenute nei provvedimenti approvati a partire dal marzo 2020. In particolare, circa 108 miliardi per l'anno 2020, 31 miliardi per il 2021 e 35 miliardi per il 2022 hanno finanziato le misure recate dai decreti-legge cosiddetti cura Italia, liquidità, liquidità, rilancio, cosiddetto agosto e cosiddetto ristori. Adesso, a questi utilizzi, vanno aggiunti quelli della legge di bilancio, che ha fatto ricorso a maggior *deficit*. Il maggiore indebitamento netto autorizzato lo scorso gennaio ha consentito di finanziare per circa 32 miliardi di euro nel 2021 le misure recate dal decreto 183 del 2020, il cosiddetto proroga termite relativo ai rischi sanitari da Covid-19, e il cosiddetto ristori 2021. Questi ultimi due provvedimenti sono attualmente in corso di esame presso le Camere. Con questa Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento Stiamo indebitando l'Italia, un attimo di silenzio! Faccio una fatica terribile; ho avuto anche il Covid. Faccio fatica a parlare!

azione di disturbo, però ha ragione. Vi prego di seguire con attenzione la collega. Prego, senatrice Faggi.

si sente solo quello che dice lei. Vada pure avanti. FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Con la presente relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'Obiettivo fissando il nuovo livello dell'indebitamento netto, in precedenza pari a -11,8 per cento del PIL nel 2021,

All'attuazione dei prossimi interventi per fronteggiare la crisi pandemica è quindi destinato un ammontare, in termini di maggiore indebitamento netto, pari a 40 miliardi di euro per l'anno 2021, a 6 miliardi per l'anno 2022, a 4,5 miliardi per il 2023, a 4,35 miliardi per il 2024 per il 2024 e a circa 6 miliardi di euro annui in media dal 2025 al 2034. Questi importi sono comprensivi, per gli anni dal 2021 al 2033, della spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo autorizzato. Dal 2034 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi. La mia relazione si conclude qui. Ho fatto un quadro di quanto indebitamento abbiamo, che, a conti fatti, ammonta a circa 200 miliardi, che dovremo ovviamente restituire. A questi si aggiunge un quadro economico che deve tenere presente anche il PNRR il *recovery fund*, con la necessità assoluta di provvedere velocemente, nei prossimi mesi, a delle riforme strutturali che tengano presente la pubblica amministrazione, soprattutto lo snellimento burocratico di tutte le documentazioni, i progetti e i disegni di di legge finalizzati a un miglioramento della situazione. In difetto di questo, in mancanza di riforme strutturali di ogni grado e di ogni tipo, mi sento di concludere che questo indebitamento sarà solo ed esclusivamente indebitamento, perché non avremo la forza e la capacità di riuscire a restituirlo, essendo troppo lenti, troppo burocratizzati, con una legislazione troppo rallentata, che non permetterà, nel momento in cui chiederanno la restituzione di questi soldi, di avere gli strumenti per poterlo fare. Tutte le relazioni contenute in questi *dossier*

prevedendo che con la vaccinazione e con la remissione della malattia si possa a poco a poco tornare a una vita normale. Sicuramente sarà così,

da questa situazione, qui nei Ministeri, qui come noi legiferiamo, saremo destinati solo ad avere i debiti. La storia lo dice: dopo le pandemie ci sono le carestie.

Signor Presidente, allo stato attuale il DEF si presenta come una mera dichiarazione di intenti, impossibile da valutare, in quanto manca il Piano nazionale delle riforme. Io già ieri in Commissione, nell'intervento in discussione generale, ho fatto riferimento a questi aspetti. Anche perché ricordo che Fratelli d'Italia

perché ricordo che Fratelli d'Italia presentò una risoluzione riferita proprio al metodo e non al merito, che chiaramente fu bocciata dall'attuale maggioranza. è stato tutto rinviato al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche questo, però, non è allegato al DEF, come richiedemmo anche qualche settimana fa, e che ancora non conosciamo a pochi giorni dalla sua consegna in Europa. Nella lettera inviata dal presidente Draghi al presidente del Senato Alberti Casellati si legge, infatti, che il DEF non reca il PNR in quanto il Governo procederà, successivamente, alla trasmissione del solo PNRR, che, ad ogni modo, ad oggi non è ancora pervenuto e di cui, pertanto, ignoriamo i contenuti. Proprio in sede di discussione del PNRR, Fratelli d'Italia aveva chiesto che quest'ultimo fosse allegato al DEF. Almeno oggi avremmo avuto qualcosa di cui discutere. Senza PNR né PNRR, il DEF di cui stiamo parlando in quest'Aula oggi Va inoltre rilevato che, rispetto alla normativa vigente, in questo documento, oltre al PNR, non è presente una lunga serie di documenti, quali il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, previsto dall'articolo 3 della legge n 196 la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, previsto dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 196; la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui al comma 9 dell'articolo 10 della legge n. il documento sulle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome; la relazione sui bisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip; la relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa del Ministero del ciclo 2018-2020, il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile previsti dall'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge n. Quanto ai contenuti, nel DEF si dà larga importanza alle conseguenze dovute alla crisi pandemica, in particolare alle cosiddette seconda e terza ondata di Covid-19 e ai necessari interventi di contenimento. Si potrebbe aprire un lungo capitolo di discussione circa il fatto che una recrudescenza della pandemia dopo l'estate era attesa e che, tuttavia, il Governo Conte 2 si è fatto trovare impreparato. Né certamente poteva fare di meglio per la terza ondata il Governo Draghi, che ha scelto di mantenere gli stessi Ministri, pur rimuovendo la figura del commissario straordinario all'emergenza, dimostratosi del tutto inadeguato. Il DEF affida le speranze di una ripresa dell'economia al contenimento della pandemia, possibile solo con una massiccia campagna vaccinale. A tal proposito, va sottolineata la confusione del Governo che, nella premessa del DEF, ipotizza di somministrare i vaccini all'80 per cento della popolazione entro l'autunno. Tale termine, nelle pagine successive, è più specificamente indicato come fine di settembre, un orizzonte che non coincide con il più vasto periodo autunnale di cui sopra. Tale termine viene aggiornato qualche riga dopo in ottobre, in caso di *gap* nelle forniture delle dosi, come quella registrata nei primi mesi di campagna vaccinale. Su questo aspetto va sottolineato il tempo perso, vista la gestione del piano di vaccinazione da parte del precedente commissario straordinario, più proiettato sull'acquisto delle primule che sull'effettiva necessità di vaccinare nel modo più rapido possibile, partendo chiaramente dai più fragili. Tuttavia, anche con un buon andamento della campagna vaccinale il DEF prevede che il periodo di restrizioni non sia finito, tanto che dice testualmente che non può escludersi che nei prossimi mesi il contenimento dell'epidemia richiederà di valutare talune e restrizioni alle attività che comportano maggiori rischi di contagio. Quindi, si prevedono ancora restrizioni che questa volta, però, potrebbero non trovare più alcun sostegno economico dal momento che sempre nel DEF, a proposito del cosiddetto decreto-legge sostegni-*bis*, con l'attuale scostamento richiesto di 40 miliardi, si legge che l'auspicio del Governo è che, grazie ad andamenti epidemici ed economici sempre più positivi nei prossimi mesi, questo sia l'ultimo intervento di tale portata. di Fratelli d'Italia è che il Governo si assuma invece la responsabilità di far ripartire le imprese, imponendo dei protocolli di sicurezza rigidi. L'apertura in sicurezza non può però più essere posticipata. Si contesta, a tal proposito, anche l'affermazione contenuta nel DEF secondo cui il sistema economico, al netto delle interruzioni operative, sembra aver raggiunto una forma di coesistenza con il virus*.* Si riscontra - prosegue il DEF - una maggiore resilienza dell'economia, verosimilmente riconducibile anche alla capacità di adattamento degli operatori sul piano sia delle scelte produttive e organizzative, che dei comportamenti sociali. parallelamente le misure restrittive, anche nelle loro forme più stringenti, appaiono meno nocive per l'attività economica di quelle della prima fase dell'emergenza. Quanto scritto in queste poche righe è di una gravità inaudita. Se l'economia italiana si fosse adattata al virus, non avremmo oggi le manifestazioni di piazza in cui tanti operatori non chiedono più *bonus* o sostegni, ma quanto di più di più onesto ci sia e cioè poter lavorare. Fin troppe attività sono ancora chiuse a causa delle restrizioni; altre sono aperte, ma con limitazioni; altre non riapriranno proprio a causa del perdurare dell'emergenza. Vogliamo sperare che l'affermazione di cui sopra - e che giova ripetere - ossia che parallelamente le misure restrittive, anche nelle loro forme più stringenti, appaiono meno nocive per l'attività economica, non sia la scusa che il Governo cerca per continuare a mantenere restrizioni senza più ragioni (una su tutte, il coprifuoco). Venendo ai dati economici, nel 2020 l'economia italiana ha registrato una caduta di PIL pari all'8,9 I dati congiunturali dei primi mesi dell'anno in corso indicano che, dopo la flessione registrata nel quarto trimestre del 2020 (meno 1,9 rispetto al trimestre precedente), il PIL ha continuato a contrarsi, sebbene in misura più lieve rispetto al calo congiunturale registrato nella parte finale dell'anno scorso. Nonostante si registrino segnali positivi dal comparto industriale, appaiono meno rosee le prospettive per il settore dei servizi, mentre si mantengono contratti i consumi.

favorita dal blocco dei licenziamenti e dalla cassa integrazione Covid. Per contro, però, va rilevata la diminuzione del tasso di partecipazione al mercato del lavoro; in pratica, il mercato degli inattivi

Secondo il DEF, in virtù degli stimoli economici e del contenimento della pandemia, il PIL recupererebbe del 4,5 per cento quest'anno e del 4,8 per cento nel 2022, per poi crescere per cento nel 2024. Nel DEF si sottolinea che si tratta di tassi di incremento mai sperimentati nell'ultimo decennio, che permetteranno all'Italia di tornare ai livelli di PIL pre-crisi nel 2023. se ciò può sembrare una vittoria, va sottolineato che il PIL del 2019 restava più basso del PIL precedente la crisi del 2008. Avendo a disposizione i fondi del Next generation EU e i 30 miliardi di euro del fondo complementare istituito dal Governo per realizzare progetti complementari, ma rimasti esclusi dal Piano nazionale, è ipotizzabile che si possa fare di più per il prodotto interno lordo nazionale. Richiedono una riflessione a parte le dinamiche demografiche rispetto al rapporto debito-PIL, illustrate nel quarto capitolo, in cui si legge che, ipotizzando invece una progressiva riduzione del tasso di fertilità cento a partire dal 2020, si osserva un incremento del rapporto debito-PIL marcato nel lungo periodo. L'invecchiamento della popolazione, unito alla diminuzione della popolazione, in particolare di quella giovane, per una riduzione del tasso di natalità,

modo nel DEF, pur sottolineando i rischi che un invecchiamento della popolazione comporta in termini di costi pensionistici, non si prevede una riforma del sistema.

crescita più alta delle previsioni, che invece ipotizzavano rimanesse quasi stabile, al 42,3 per cento. È significativo che nell'anno della pandemia, del calo dei consumi e dei redditi, ciò che è aumentato sono le tasse. Auspichiamo sia vero quanto riporta il DEF, ovvero che nel 2021 la pressione fiscale scenderà al 41,3, per arrivare al 40,9 nel 2024. Va segnalata, inoltre, la questione delle regole di bilancio. Il Documento di economia e finanza e il ministro Franco hanno confermato che il Patto di stabilità e crescita resterà sospeso anche nel 2022, mentre probabilmente tornerà in vigore nel 2023, salvo discussione annunciata in merito. Su questo punto manca un impegno del Governo a far sì che il Patto di stabilità o le nuove regole sui vincoli di bilancio tornino in essere solo al termine dell'erogazione dei fondi compresi nel Piano nazionale di riforme; altrimenti potrebbe verificarsi una doccia fredda, in particolare per gli enti locali. Quanto, invece, allo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro, necessario per sostenere le misure contenute nel decreto-legge sostegni-*bis*, il Governo chiede al Parlamento di fidarsi e di accettare al buio, un po' come firmare un assegno in bianco. Apprezziamo l'intento dichiarato dal Presidente del Consiglio di fornire ulteriori aiuti alle imprese. Ma, se guardiamo indietro a quanto avvenuto in occasione dei decreti ristori 1, 2, 3, 4 e all'attuale decreto sostegni, che stiamo discutendo...

Va sottolineato, infine, come per la crescita e il rilancio il Documento di economia e finanza introduca alcune riforme, a partire da una riforma fiscale, di cui però non si conoscono i contenuti: non è chiaro se si riferirà alle persone fisiche o al costo del lavoro, piuttosto che ad altri settori. In definitiva, le previsioni del DEF fanno affidamento sul PNRR e sul decreto sostegni-*bis*, ma entrambi sono documenti che al momento non conosciamo e ciò rende questo Documento di economia e finanza vago, timido e incolore.

la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Pertanto, l'esame del documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo, relativo alla Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012,

la mia forza politica ha sostenuto il Governo Draghi. La risposta che mi sono data è stata un atto che risponde agli indirizzi e ai motivi per cui si è deciso di fare questo tipo di scelta. Sarò breve, perché ovviamente sappiamo tutti che siamo in una situazione particolare, con la sospensione temporanea delle regole di bilancio, con degli indebitamenti - lo ricordava prima la collega - che non sarebbero stati neanche immaginabili fino a un paio di anni fa, con la sospensione delle regole per gli aiuti dello Stato e con la prospettiva del Piano di resilienza che verrà analizzato la prossima settimana.

delle previsioni con riferimento agli indebitamenti e alla previsione generale macroeconomica comunque prudenti. Quello che vorrei far notare ai colleghi è che si è sempre detto che i Governi

ma c'è anche una valutazione che si riferisce ai rischi collegati che è stata, tra l'altro, esaminata e sottolineata anche dal documento depositato dall'Ufficio parlamentare

significative. Per esempio - lo dico perché è sempre stato un punto sottolineato anche da Forza Italia - Confindustria ha espresso delle

in prima linea nella guerra alla pandemia - ha sottolineato come la previsione complessiva delle risorse è quella che ci si aspettava, indipendentemente poi da alcune correzioni.

vuoi perché calcola anche le ipotesi di rischio e vuoi perché ha un quadro complessivo anche di sostegno da parte delle categorie che evidentemente hanno prima condiviso il testo,

Noi abbiamo bisogno di una tipologia di impostazione che risponda a queste necessità, ossia che abbia una visione complessiva e sappia dare determinate risposte, sapendo che viviamo sì in un momento particolare, ma che un domani i Governi che verranno dovranno affrontare il debito. Se questo Governo riesce nell'intento fondamentale di tirarci fuori

ridiscuterà i parametri con cui si sta insieme in Europa, con tutte le conseguenze del caso. Ecco perché la visione prospettica è fondamentale ed ecco perché ritengo che, se le forze politiche con grande fatica con grande fatica ma in forma responsabile seguono questo percorso, lo fanno proprio perché c'è una necessità di visione prospettica che tenga conto del quadro di oggi, dei rischi di domani, ma anche della necessità di far crescere il nostro Paese. *(Applausi)*.

La prima è sul Governo Draghi che, nonostante numerose difficoltà, mostra una qualità di lavoro molto buona: corretto, efficace e tempestivo nelle decisioni, autorevole e credibile. Sullo strappo di ieri per un'ora di *lockdown* in meno, resto alle cronache: il Governo era compatto, il capo di un partito di maggioranza no; è sempre grave, ma non è la stessa cosa. La seconda considerazione è sul ruolo del Parlamento, in un tempo nel quale le sue funzioni si sono largamente ridotte. Nella sorta di stato di eccezione permanente che stiamo vivendo, è legittimo che il Governo assuma più forza e maggior peso, ma non è questo il punto. Il punto è emerso nella seduta di ieri, quando le riserve del presidente Romeo sul cosiddetto disegno di legge Zan contro l'odio discriminatorio hanno aperto tra di noi un dibattito sul tema, vitale per il Senato, del margine che resta al Parlamento per legiferare su questioni diverse dai provvedimenti anticongiunturali del Governo. Apro una parentesi anche riferendomi all'intervento di ieri del senatore Quagliariello: gli anni Settanta, anni di terrorismo e di maggioranza di emergenza, sono stati ricchi di grandi riforme istituzionali e di grandi leggi fortemente divisive sui diritti civili. Anzi, ripensando a quegli anni con gli occhi di oggi, possiamo dire che fu proprio quell'interagire tra misure antiterrorismo, provvedimenti economici, decisioni istituzionali e nuovi diritti civili a salvare l'Italia da una catastrofe assoluta. Questo tema, che poi è il tema della complessità della vita, si ripropone adesso anche per noi. In questo contesto, il Documento di economia e finanza che stiamo esaminando con lo scostamento di bilancio, assieme alla relazione, al Piano nazionale di ripresa e all'ultimo rilevante decreto-legge, acquista un rilievo che va oltre le cifre molto importanti che questi provvedimenti espongono. Stanno qui, nella concomitanza di emergenze, urgenze e scadenze indifferibili, le fondamenta degli interrogativi sui margini rimasti al Parlamento, al di là dell'approvazione degli atti del Governo. Da mesi il Senato lavora a scartamento ridotto, come se vivessimo in un altro mondo, tranquillo e lontano dai drammi del mondo reale. La partita si gioca tutta tra la società italiana e il Governo e di questa partita il Parlamento è spettatore privilegiato, ma pur sempre spettatore. Nel mondo è nato un cambiamento che non si è ancora stabilizzato e sulla scacchiera mondiale resta incerto l'esito della partita tra le grandi e le medie potenze. In una fase così delicata, nell'Europa post-Brexit e con l'uscita di scena della cancelliera Merkel, le opportunità offerte dall'autorevolezza della Presidenza Draghi dovrebbero suggerirci di fare del Senato il centro di un grande dibattito politico sulle due questioni, squisitamente parlamentari, alle quali è legato il nostro futuro: l'Europa e la democrazia. Invece il Parlamento non solo ha perso gran parte del suo potere legislativo, ma ha anche rinunciato ad aprirsi ai grandi confronti politici che potrebbero dar forma al suo ruolo di indirizzo sulle prospettive del Paese. La sfida tra le democrazie e i sistemi autoritari finirà non con un compromesso, ma solo con vincitori e vinti. La vicenda tra Draghi ed Erdogan, nella quale sto totalmente dalla parte del è solo un ultimo segno, non minore, di quanto sia aspro questo confronto. Qualche giorno fa il presidente Biden, che ha già annunciato una conferenza mondiale sulla democrazia, testualmente, che i nostri figli e i nostri nipoti faranno le loro tesi di laurea su chi avrà avuto più successo e su chi avrà vinto tra democrazia e autocrazia. La XVIII legislatura, la nostra, non sarà costituente, come pure avrebbe potuto essere. Auguriamoci che lo sia la prossima, pur così diversa dalle precedenti, per il ridotto numero dei parlamentari. Nei confronti di chi verrà eletto nel nuovo Senato abbiamo numerosi doveri, non solo di adeguare la Costituzione e il Regolamento alla riduzione del numero dei senatori, ma anche di lasciare una traccia sulle future riforme. Il Governo Draghi si è insediato pressato da due urgenze, la lotta al Covid e le scadenze del *recovery plan*, ma senza riforme strutturali neanche i miliardi dell'Europa ce la faranno mai cavare. Il Governo sta lavorando alle riforme del sistema economico, tutte misure necessarie, indispensabili e urgenti, ma ancora più in alto c'è la grande questione del riassetto dei poteri dello Stato, del Parlamento e del Governo. Sono queste le pietre angolari traballanti del nostro sistema istituzionale che, da mezzo secolo, tengono l'Italia in una crisi permanente e che, a cascata, bloccano l'intero apparato dello Stato. Occuparcene, oggi, è il primo dovere del Parlamento, non del Governo. Questo è il nostro spazio: scegliere tra una democrazia robusta ed efficiente e un sistema fiacco e inconcludente, destinato a soccombere nella sfida con l'autoritarismo. Dobbiamo impostare con franchezza e onestà intellettuale un calendario dei nostri lavori che preveda sessioni di lavoro capaci di restituire al Senato il suo ruolo di indirizzo. Solo un quadro istituzionale solido potrà garantire successo al DEF, al PNRR, alla prossima legge di bilancio e ai tanti decreti di sostegno. Un dibattito franco e onesto significa che sull'Europa dobbiamo saper scegliere dove stare, tra un'Europa di Nazioni e un'Europa federale, tra un'unione tecnocratica e un'unione politica, tra i pieni poteri della Polonia e dell'Ungheria e la democrazia. Significa che la nostra Costituzione, a sua volta, deve scegliere tra bicameralismo perfetto, bicameralismo differenziato e monocameralismo; tra parlamentarismo all'italiana, semipresidenzialismo alla francese e cancellierato alla tedesca. Significa che dobbiamo esprimerci su cosa resti del XXI secolo, della divisione dei poteri e dello Stato di diritto. Significa, infine, che la democrazia deve sapersi difendere dal potere antidemocratico delle grandi multinazionali private. Signor Presidente, dibattere sull'Europa e sulla democrazia è strettamente connesso alle vicende drammatiche della crisi. Né il DEF né il PNRR saranno mai in grado di salvarci senza una forte impalcatura delle istituzioni e nemmeno se la nostra democrazia non saprà crescere in efficienza. Egualmente, nel nuovo mondo, nessuna Nazione europea potrà mai essere da sola un attore globale. Solo una struttura federale ci può salvare. Oggi, con il Governo intento a battere la crisi, occuparci dell'Europa e della democrazia è un dovere di noi parlamentari, è solo nostro. Accontentarci del pur rilevante compito della conversione dei decreti-legge del Governo ci caricherebbe sulle spalle una pesante responsabilità nei confronti delle future generazioni. *(Applausi)*. La ringrazio, senatore Zanda, per il suo intervento che, al di là del merito, sul quale si può convenire o dissentire, riconcilia con la qualità degli interventi di questo Senato. È iscritto Signor Presidente, ho buttato via l'intervento che avevo preparato, perché preferisco stare sulla scia di quanto ha sostenuto ora il senatore Zanda. infatti, due modi per stare nel dibattito di oggi: un modo corretto è rimanere legati ai dati e alle prospettive di natura finanziaria ed economica; un altro, di di supporto, è comportarsi da senatori e, quindi, di provare a intravedere cosa potrebbe accadere in un mondo completamente rovesciato. Se la pandemia si fosse conclusa a pochi mesi dal suo inizio, nulla sarebbe accaduto. Ma ormai dobbiamo cominciare a pensare a come gestire effetti continuativi della pandemia, ancorché ciascuno di noi venga vaccinato. è positivo il Piano che il Governo presenta, così come questo quadrilatero che è fatto di misure di emergenza, riforme strutturali, PNRR e interventi pubblici, ma senza dimenticare l'architettura istituzionale,

tra il marzo 2020 e l'aprile 2021, considerato lo scostamento annunciato dal Governo di fine aprile, i Governi italiani hanno già impegnato una somma pari a 202 miliardi di euro, mesi abbiamo già esaurito il PNRR. Sappiamo quindi che il PNRR non può essere considerato decisivo per ribaltare, in una condizione storica rovesciata, le sorti dell'Italia. Non ho molto tempo e, quindi, vado per capitoli, con la premessa che bisogna abituarsi a convivere durevolmente con gli effetti della pandemia. Pertanto, in primo luogo i sostegni non possono essere dati a tutti: a Nencini non può essere dato alcun sostegno per l'acquisto di un monopattino, né di una bicicletta; bisogna scavare all'interno e premiare e sostenere chi ha più bisogno. Le imprese farmaceutiche o alcune imprese che hanno prodotto alimentari non possono godere degli stessi sostegni di piccole e medie imprese che sono in crisi e bisogna mettere più soldi per queste

o diversamente non saremo in grado di governare una fase durevole degli effetti della pandemia. L'ultima questione riguarda Queste misure, signor Presidente, rappresentanti del Governo, certo che appartengono a uno Stato, certo che servono agli italiani, ma sarebbe sconsiderato,

con un solo Ministro delle finanze e un'unica politica economica e di difesa, o altrimenti, nella sfida fra Stati Uniti e Cina, l'Europa non avrà alcuna possibilità di scampo. Saremo un mercato, metteremo denari per superare la fase dell'emergenza pandemica, ma non avremo alcuna felicità alla fine del nostro destino. Di questo deve parlare il Senato della Repubblica italiana: deve, cioè, proporre una seduta il cui titolo sia rifare l'Italia, come pensiamo che debba essere,

per tre anni ho iniziato ogni mio intervento salutando la Presidenza, il Governo e i colleghi. Questa volta, invece, invertirò l'ordine e lascerò il Governo per ultimo perché è direttamente al Governo che mi rivolgo,

perché, nonostante i proclami di quasi cinque anni fa, la ricostruzione non verrà finanziata per intero. A diversi colleghi qui dentro potrei dire: «Ve l'avevo detto!». Glielo avevo già detto quasi cinque anni fa, ma non è questo il punto. è che quegli accolli, che in qualche caso saranno importanti nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro, avrebbero potuto essere abbattuti utilizzando i vari *bonus* attualmente vigenti: il *bonus* sisma, il *bonus* facciate, il superbonus e i vari *bonus* previsti in questo momento. Tuttavia, mi riferiscono che un parere dell'Agenzia delle entrate - di cui sono stato messo a conoscenza di recente e che non ho letto non ho letto - prevede l'impossibilità di doppio finanziamento; quindi, con riferimento agli edifici che ebbero un contributo per la ricostruzione dopo il terremoto di Marche e Umbria del 1997, si prevede che prevede che non possano beneficiare degli attuali bonus. A mio parere, invece, l'Agenzia sta sbagliando, perché la ricostruzione non dovrebbe essere disciplinata da princìpi generali e ordinari: implicitamente questo divieto è già stato superato dal fatto che effettivamente la ricostruzione verrà finanziata anche questa volta. Inoltre, non si tiene conto della specificità delle norme che disciplinavano la ricostruzione del 1997. Entro così nel dettaglio. La disciplina generale della ricostruzione pesante era contenuta nella legge n. 61 del 1998, che non riconosceva il 100 per cento del costo, perché veniva dato un contributo secondo un computo metrico, e quindi impropriamente a piè di lista,

percentuale che ovviamente si riduceva per i redditi più alti. Quindi, prima considerazione: essendo previsto un accollo, è evidente che c'era la partecipazione del privato, come è evidente che sarebbe arbitrario escludere dal beneficio dei *bonus* chi andasse a ricostruire adesso. Seconda considerazione: la ricostruzione del 1997 non pagava il miglioramento o l'adeguamento sismico, ma dava un contributo per il ripristino del danno. Vorrei sapere, allora, se qui dentro c'è qualcuno che pensa che intervenire esclusivamente per il ripristino del danno in un edificio del 1500, del 1600 o del 1700, in uno dei tanti centri storici interessati da quella ricostruzione, possa essere motivo di esclusione da un ulteriore intervento, visto che, non essendoci stati né l'adeguamento né il miglioramento sismico - se escludiamo i casi di demolizione e ricostruzione - è chiaro che diventa arbitrario escludere quelle fattispecie. È evidente, infatti, che in un edificio del 1500 a cui si ripristinano solo i danni non si eliminano le criticità, rendendolo quindi vulnerabile alla nuova sollecitazione. Un'ultima considerazione è che la ricostruzione - come ho detto prima - era distinta in pesante e leggera; quella leggera, nelle Marche, ad esempio, era disciplinata dalla legge n. 121, che prevedeva un contributo massimo di 60 milioni. Ciò Ciò significa che in molti casi si dava un contributo di poche migliaia di euro. Sembra giusto a tutti i colleghi in quest'Aula che, per aver percepito qualche migliaio di euro vent'anni fa, ora si sia esclusi dalla possibilità di percepire un *bonus*? Io sono d'accordo sul fatto che bisogna contribuire al rilancio dell'economia e, quindi, concordo sul *bonus* e sul *superbonus*, sul *bonus* facciate, sul *bonus* sisma ed anche sul *bonus* giardini.

proprietà degli edifici, di socialità. Quelle popolazioni poi furono costrette ad abbandonare i propri luoghi di nascita e andare in qualche casa a centinaia di chilometri - e da un punto di vista sanitario - in quelle zone è più che raddoppiato il consumo di ansiolitici - e quindi in termini anche sanitari l'impatto del terremoto è stato notevole? Dopo tutto questo, troviamo giusto escludere quelle persone dalla possibilità di beneficiare, appunto, dei contributi previsti per chi fa un intervento ordinario discrezionale adesso? Quello che chiedo, quindi, non è un trattamento di favore: chiedo di non discriminare quelle popolazioni. E preciso che tutto quello che sto dicendo è contenuto nell'osservazione ad un parere, non è disciplinato dal DEF. Per questo ci siamo attivati come Gruppo e come ufficio legislativo, ma chiedo al Governo di rendere inutile quel lavoro. A noi non interessa mettere una bandierina su un provvedimento a prendercene i meriti: a noi interessa solo ed esclusivamente risolvere un problema. Quindi, rendete inutile il lavoro che stiamo facendo adesso; intervenite prima voi; date un parere autentico all'Agenzia delle entrate; evidenziate che la ricostruzione è speciale e deve essere gestita secondo non i principi ordinari dell'ordinamento, ma secondo le necessità specifiche della ricostruzione. Superate questo problema e sarò il primo ad essere

la crisi pandemica che ha sconvolto non solo l'organizzazione sanitaria, ma anche la struttura stessa di tutte le collettività coinvolte, con i conseguenti sconvolgimenti economici e sociali che ognuno ogni giorno ha toccato e tocca con mano, condiziona le scelte programmatiche di ogni Governo. Priorità ovviamente deve essere data alle misure in materia sanitaria. Se le stesse saranno efficienti, efficaci, adeguate e orientate nella giusta direzione, si ripercuoteranno con effetto domino sulla ripresa economica, sulle riaperture delle attività e degli esercizi commerciali, sul rilancio dell'occupazione e più in generale sulle modalità del vivere la quotidianità e sul ritorno ad una convivenza sociale non più dettata da distanziamenti e isolamenti. Massima attenzione e priorità devono essere rivolte alla campagna vaccinale, ad una sua più adeguata organizzazione, o meglio riorganizzazione, ad una sua migliore omogeneizzazione sull'intero territorio nazionale, alla disponibilità di un numero di dosi vaccinali finalmente sufficiente per farla decollare e riuscire a raggiungere fasce sempre più ampie della popolazione, permettendo in tal modo entro l'autunno di raggiungere l'immunità di gregge o di massa. Tutto ciò rappresenta, in ogni caso, il punto nodale da considerare e premessa vincolante per gli altri provvedimenti. Nel campo sanitario sono inoltre indispensabili - come anche previsto dal Governo - un rafforzamento ed una più ottimale organizzazione del Sistema sanitario nazionale, cercando - da un lato - di compensare le carenze e le criticità emerse ed evidenziatesi in modo così eclatante e drammatico durante la pandemia - di avere una struttura sanitaria che dia sempre maggiore rilevanza alla prevenzione, con un particolare riconoscimento all'importanza della riabilitazione e del reinserimento sociale e lavorativo del paziente non più acutamente malato. una nuova visione prospettica della risposta sanitaria che sia sempre più commisurata ai bisogni reali dei cittadini, in cui un punto basilare è rappresentato dall'assistenza territoriale e di prossimità e fondata su un'organizzazione che non sia più eccessivamente centralizzata, ma capace, anche con l'aiuto della telemedicina, di ridurre il sovraccarico dei pronto soccorso e delle corsie ospedaliere. Essa deve essere capace di dare, inoltre, la massima attenzione alle patologie croniche, con tutti i risvolti familiari e sociali, alla disabilità, con le molteplici e complesse problematiche che la accompagnano, le quali non devono rappresentare più le necessità del singolo, ma coinvolgere tutta la collettività. Tutta la missione salute compresa nel PNRR, con il grande risalto dato all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, come d'altronde a tutti gli assi strategici in cui il Piano si sviluppa, richiede ovviamente impegni economici e investimenti importanti. Non dimentichiamo, tra gli obiettivi previsti, anche l'ammodernamento necessario delle strutture sanitarie, delle attrezzature e delle apparecchiature tecnico-scientifiche in esse operanti, condizione quest'ultima sempre più irrinunciabile, visti i grandi progressi della scienza e della tecnologia nei percorsi diagnostici aggiornati e nelle nuovissime tecniche terapeutiche utilizzate per patologie prima mai diagnosticate precocemente o ritenute non trattabili o aggredibili. Da ciò scaturisce la necessità di un ulteriore scostamento di bilancio, resosi necessario per contrastare non solo l'emergenza Covid, come già detto, ma - ribadisco - per una profonda opera di rinascita del nostro Paese, una nuova primavera dello sviluppo e della crescita economica. Dopo la difficile, lunghissima e durissima resilienza l'Italia, in un contesto europeo sempre più aperto, più sensibile e più solidale alle esigenze, alle necessità e alle problematiche dei singoli *partner*, può e deve intraprendere la strada maestra della ripresa. A proposito di Europa, non posso non fare un passaggio sul contratto - che non esagero a definire capestro - siglato dal commissario europeo della salute con i vertici della Pfizer il 20 novembre scorso, pubblicato ieri dal giornale spagnolo «La Vanguardia». Al di là del prezzo di listino più alto di quello preventivato, a colpire sono soprattutto due aspetti. Il primo è l'assenza di penali previste a carico dell'azienda in caso di inadempienza o ritardi nella fornitura delle dosi di vaccino e del loro numero; il secondo, ben più grave secondo me, è la dettagliata esclusione di responsabilità di Pfizer da eventuali danni a terzi. Una volta che il vaccino è consegnato ai singoli Paesi, decade qualsiasi ipotesi di risarcimento, anche per eventuali reazioni o effetti collaterali non descritti nella scheda tecnica del farmaco.

dopo questo dovuto passaggio, concludo dicendo che è mia convinzione affermare che sia fondamentale e condizione irrinunciabile il corretto utilizzo delle risorse recuperate e indirizzate verso programmi di investimento condivisi, capaci effettivamente di incidere sulla qualità della vita dei cittadini per poter guardare con una nuova e ritrovata fiducia al futuro. Facciamo sì che, con il contributo di tutti, quell'inno di speranza «andrà tutto bene», che più di un anno fa alleggiava nella triste atmosfera del primo *lockdown*, possa diventare una concreta certezza oggettivamente realizzabile. *(Applausi)*.

svolgere un'analisi su un documento particolarmente importante per le istituzioni di un Paese: il DEF. Quest'ultimo però è un documento che, come avrò modo di dimostrare, certifica innanzitutto il fallimento della precedente esperienza di Governo. Come il *recovery plan*, il PNRR, è stato un po' il *casus belli* che ha fatto cadere il Governo Conte, il DEF rappresenta la fotografia che ne certifica il fallimento. Perché lo dico? Mi rivolgo proprio al nuovo Governo: state attenti a non inciampare sugli stessi ostacoli che hanno certificato il fallimento del Governo Conte. Le libertà costituzionali, onorevole Sottosegretario, Sottosegretario, che il Governo Conte ha violato ripetutamente, in disprezzo dei lavoratori e dei cittadini italiani, quelle libertà costituzionali, ahimè, nonostante la posizione ferma e decisa di Fratelli d'Italia, continuano a essere violate anche dal suo Governo, onorevole Sottosegretario. Non è accettabile che si continui con i coprifuoco, non è accettabile che le persone vengano controllate se rientrano a casa alle dieci e mezza di sera. Non è accettabile! Non è accettabile, signor Presidente, che si continui con *lockdown* immotivati. Imparate da Stoccolma, imparate da Madrid, città che non rappresentano il terzo mondo e che sono messe meglio di Milano, meglio delle nostre metropoli. Questo dovete fare, se avete un minimo di dignità e di rispetto per questo Paese. E invece no, invece si continua: chiusura alle

quelle che avete previsto nel decreto sostegni sono elemosine, e li tenete chiusi. Ebbene se violando le libertà costituzionali il Governo Conte è caduto, violando le libertà costituzionali, onorevole Sottosegretario, il Governo Draghi certamente non farà molta strada, ma soprattutto - ahimè - non ne farà il nostro Paese. Per quanto riguarda il debito pubblico, i numeri certificano che quest'anno arriveremo intorno al 160,5 per cento nel rapporto debito-PIL. Gli appassionati di storia economica ricorderanno che i livelli di rapporto debito-PIL che questo DEF purtroppo certificherà, per gli sbagli dei Governi precedenti e anche di questo Governo,

Voglio ricordare, a titolo di confronto, che durante la Seconda guerra mondiale o durante la crisi del 1929 il rapporto tra debito pubblico e PIL era di poco superiore all'85 Cerchiamo di capire dove state arrivando. Ebbene, in questo problema del debito, quali sono le prospettive che potremmo cercare di derivare dal DEF? Sono alquanto misere, signor Presidente, perché, per poter uscire dal debito e per migliorare il rapporto debito-PIL abbiamo bisogno anzitutto di una cosa: di crescita. Ebbene si può pensare seriamente e razionalmente alla crescita, nel momento in cui non parliamo di politiche agrarie e di politiche industriali

Questa è la crescita: coniugare le politiche agrarie e industriali per lo sviluppo del Paese. Nulla di tutto ciò, purtroppo, possiamo rinvenire nelle politiche che deriviamo dalla lettura prospettica del DEF. Ma anche sui grandi temi cosa state facendo? Vorremmo delle risposte sulla proprietà immobiliare. Ieri c'è stata una maratona di Confedilizia per testimoniare un grido di dolore della proprietà immobiliare italiana di fronte a situazioni assurde. Penso ai sedici mesi di blocco degli sfratti. Voi avete addossato alla proprietà immobiliare italiana un ruolo di *welfare* che spetterebbe allo Stato. Voi lo avete addossato al cittadino: è ingiusto, è incostituzionale! Voglio pensare anche ad altro. Voglio pensare a quello che non state facendo per due pilastri dell'industria italiana. Penso all'Ilva, al polo della siderurgia. Le nostre imprese stanno oggi combattendo con la crescita dei prezzi delle materie prime, anche perché noi non abbiamo più una leva determinante nel polo della siderurgia italiana. Ma non basta l'Ilva, che dovrebbe essere il primo pilastro a sostegno della nostra impresa. Grazie, invece, anche agli attacchi vergognosi che pochi anni fa il primo partito presente in Parlamento ha fatto all'unica industria siderurgica italiana, avete rovinato e state rovinando tutta l'industria italiana! E non ve ne preoccupate, onorevole Sottosegretario! Cosa state facendo per ridare all'Ilva quella dignità di cui lo Stato italiano necessita, di cui l'economia italiana necessita? Un altro caposaldo per la ripresa del Paese il turismo e state distruggendo anche l'Alitalia. State continuando a distruggere anche l'Alitalia, che è un cardine essenziale per lo sviluppo turistico del nostro Paese. Ecco perché, quando vogliamo parlare di crescita, nel leggere i numeri fantastici, mi viene quasi da dire, che proiettate nelle previsioni del 2021, 2022, 2023 e 2024, dovrebbe venirmi da ridere, ma invece mi viene da piangere. Signor Presidente, cosa vogliamo dire sul debito pubblico nato nel 2020 e sul debito pubblico che sta nascendo nel 2021? Ricordo che, tra i 70 miliardi di queste

altrimenti non ne usciremo. Do atto al presidente Draghi di avere fatto, almeno tra le righe, qualche accenno alla necessità di smuovere il Patto di stabilità

voglio sottolineare due punti. Innanzitutto, la gravità della mancanza del PNR e, soprattutto, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarebbe un fondamento del DEF, ma noi non lo conosciamo. Già sappiamo, purtroppo, che il Parlamento non entrerà nel merito, ma semplicemente lo apprenderà, così come, da quanto mi risulta, lo apprenderanno passivamente anche i Ministri e i partiti di Governo. È inaccettabile, un grave *vulnus* democratico. Infine, concludo davvero con una fotografia del... Concludo dicendo che il DEF fotografa, in modo inequivocabile, anche le critiche che noi abbiamo rivolto al Governo, perché perché le entrate tributarie, come le entrate generali dello Stato, sono diminuite nel 2020, come era ovvio prevedere, ma sono però aumentate in rapporto al PIL. Ciò vuol dire che avete addossato alla classe produttiva del Paese, alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, ai professionisti e alle imprese, il 99 per cento degli effetti drammatici di questa crisi. Lo certifica il DEF.

colleghi, discutiamo il Documento di economia e finanza 2021 in una fase molto difficile. Il 2020 è stato l'anno della peggiore recessione dal Dopoguerra, mentre il 2021 sarà l'anno dell'avvio del recupero, la ripresa è ancora parziale e soprattutto molto diseguale. I settori manifatturiero e dell'edilizia sono tornati a crescere e il digitale è esploso, mentre il terziario fa molta più fatica, con interi settori che hanno subito perdite tremende e impiegheranno molto tempo prima di riguadagnare i livelli di prima di prima della pandemia. È in gioco la tenuta sociale e democratica del Paese e l'Italia ha il dovere di stare vicina a chi sta soffrendo la crisi: crisi: i precari lasciati a casa, i cassaintegrati, gli studenti costretti alla didattica a distanza, le donne e i giovani che sono i primi perdenti di questa crisi. ai commercianti, agli artigiani e ai piccoli imprenditori, obbligati a limitare o sospendere le proprie attività senza poter contare su una rete di protezione adeguata. Abbiamo il dovere morale di comprendere i sentimenti di questo popolo di lavoratori: il disagio, l'umiliazione, la rabbia e la paura di non farcela. Abbiamo il dovere politico di rispondere con fatti concreti. signor Presidente, ma dobbiamo farlo in sicurezza e in modo irreversibile, tenendo conto della realtà e non delle *fake news*.

Il Governo ha deciso ora un calendario di riaperture, assumendosi un rischio ragionato, come ha detto il presidente Draghi. Il dovere delle forze che sostengono la maggioranza e il Governo è aiutare e aiutare e condividere questa scelta e non di giocare al più uno e al distinguo dopo aver votato e condiviso le scelte in Consiglio dei ministri. Dobbiamo rispondere con i fatti, il che significa accelerare la campagna di vaccinazione e aiutare chi è in difficoltà finché dura l'emergenza. Il cosiddetto decreto sostegni, che abbiamo iniziato a discutere in Commissione bilancio, è stato concepito prima dell'ultima ondata di contagi, delle nuove misure restrittive e delle nuove chiusure. Il Partito Democratico è stato tra i primi a chiedere che le risorse del nuovo scostamento che voteremo oggi vengano destinate alle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi e a quella parte del mondo del lavoro che più sta soffrendo le conseguenze della crisi. Il Governo ha risposto positivamente e nel DEF ha scritto, nero su bianco, cosa verrà inserito nel nuovo decreto. L'impianto ci convince perché va nella direzione giusta; è necessaria una nuova tornata di ristori, facendo arrivare i soldi il più rapidamente possibile. Il fattore tempo sconsiglia di cambiare meccanismo rispetto al primo decreto sostegni, perché è meglio replicare in automatico per far arrivare i soldi prima e, semmai, aggiungere robusti interventi che riducano i costi fissi, gli affitti, le bollette e le tasse comunali. È necessario intervenire sulla liquidità

Dobbiamo iniziare a ragionare su un intervento strutturale perché non ci sarà ripresa finché migliaia e migliaia di aziende saranno schiacciate da quei debiti o dovranno sacrificare i nuovi investimenti per pagare la quota capitale e gli interessi del debito che hanno contratto in questi mesi. Signor Presidente, la sfida più difficile della politica economica in questa fase è tenere assieme l'emergenza e il rilancio dello sviluppo, che è la via maestra per riportare sotto controllo il debito, che è arrivato al 160 per cento del PIL. Il DEF si pone esattamente questo obiettivo: da una parte, lo scostamento (i 40 miliardi che devono finanziare quello che noi abbiamo chiamato il decreto imprese, lavoro e professioni), dall'altra, la scommessa per il futuro, lo *shock* di investimenti pubblici e le riforme strutturali da discutere e approvare in pochi mesi. Spendere tutti i 237 miliardi del PNRR entro il 2026 comporta un cambio di passo radicale per la pubblica amministrazione nel nostro Paese. Negli ultimi sei anni abbiamo realizzato 243 miliardi di investimenti. Nei prossimi sei anni vogliamo aggiungere altri 154 miliardi di spese aggiuntive (il 65 per cento in più). Noi possiamo scrivere il Piano nazionale per la ripresa più bello d'Europa, ma se continueremo a impiegare 16 anni per realizzare le grandi opere, come accade oggi nel nostro Paese, non andremo da nessuna parte. *(Applausi)*. È per questo che, contestualmente alla presentazione del PNRR, è necessario intervenire sulla normativa, sulla *governance* per l'attuazione del Piano. È necessaria una catena di comando chiara, un coordinamento stretto tra chi realizzerà queste opere. Bisogna snellire le procedure, la capacità di progettazione va migliorata, i funzionari vanno responsabilizzati, vanno cambiate le modalità di monitoraggio e di rendicontazione. Dobbiamo inoltre valorizzare il ruolo del Parlamento anche nella fase di attuazione. Credo che l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale che controlli, verifichi e dialoghi con il Governo nella fase di attuazione del Piano sia indispensabile, così come indispensabile è predisporre canali attraverso cui le parti sociali, la società civile e i singoli cittadini possano accedere alle informazioni, interloquire con le amministrazioni, controllare l'*iter* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Signor Presidente, il mondo dopo il Covid cambierà profondamente e rifare l'Italia oggi è... esattamente come cento anni fa, dopo un altro Dopoguerra. Le riforme servono per il cambiamento e il DEF le indica per titoli: pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza, ammortizzatori sociali e fisco. Sono temi politicamente potenzialmente divisibili. Per realizzare queste riforme servirà una chiara assunzione di responsabilità delle forze che sostengono questo Governo e una forte capacità di sintesi politica del Governo e del Presidente del Consiglio. L'Italia ha bisogno di un patto per la ricostruzione, di un patto sociale, come quello che nel 1993 portò il Paese fuori

il proprio contributo di idee. È necessario che lo stesso avvenga da parte di tutte le forze politiche e sociali perché, oggi più che mai, abbiamo il dovere di mettere al primo posto l'Italia e di fare tutto quanto è necessario - *whatever it takes*, direbbe il Presidente del Consiglio - per aiutare l'Italia a ripartire.

promulgazione del sistema codicistico (1942) che costituisce ancora l'architrave del nostro sistema giuridico. Invece

servendo all'aperto sia parecchio difficile, almeno per un mese o due, e che occupare gli spazi, strade e parcheggi, ingeneri discussioni che vanno anche alle mani. Faccio presente al Governo (che rimane rappresentato) un altro problema, quello del rinvio del termine dell'approvazione dei conti consuntivi dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio: so che c'è un dibattito in corso e chiederei un'accelerazione e una definizione. Ma veniamo ai numeri del Documento sono numeri che fanno rabbrividire. C'è una contrazione delle entrate fiscali, evidentemente per le concessioni date di rateizzazione, dilazione e rinvio e anche perché

Ripeto queste cifre che in Assemblea sono note a tutti, proprio perché fanno rabbrividire. Eppure ci sono segnali contrastanti: i BOT e i BTP e cinquant'anni nelle aste dei giorni scorsi sono andati a ruba, con un interesse dello 0,75 per cento per i primi quattro anni che poi cresce leggermente. Ci sono state richieste da tutto il mondo. L'Italia gode ancora di una certa fiducia, per una serie di motivi. Abbiamo, però, la capacità di rimborso, che ci hanno insegnato a scuola, del debito pubblico, del debito con l'Europa, del debito con la Banca

Le classi dirigenti di oggi, quelle non politiche della pubblica amministrazione e il CEO capitalismo, non capiscono più queste cose perché lavorano sugli algoritmi e non conoscono più la realtà.

Se si sviluppa il lavoro come deve svilupparsi, pubblico e privato, ci saranno dei problemi per l'ambiente, perché, prima di arrivare all'economia circolare, al rimboschimento, a tutti i propositi che facciamo e che sono largamente condivisibili, lavorare

è una bestemmia: si può proporre e può essere segno di un cambiamento, di una regolarizzazione dello stato di fatto. Quali sono gli umori della gente? La gente che parla con noi ci chiede

I privati hanno voglia di investire, ma vogliono certezze. È stato approvato ieri il decreto per le riaperture e si sono ingenerate delle discussioni. È l'inizio di una qualche certezza, per la quale ci vuole anche un po' di fortuna. Soprattutto occorre che il presidente Draghi - o chi per lui - acquisti vaccini in tutto il mondo a qualsiasi prezzo. Poi la struttura dell'Italia è in grado di vaccinare.

Purtroppo viviamo in un momento in cui, per colpa o per merito dei *social*, delle televisioni e dei giornali, c'è troppa polemica. Ma questa è la società, questo è il mondo e questi sono i tempi. Sta passando l'idea che

Non c'è stata riduzione della spesa pubblica, ma ci sono alcune richieste assurde da parte di settori che non sono stati toccati. Questo mi fa dire che la crisi che c'è nella società è anche molto prepolitica: non dipende soltanto da noi, ma da un cambiamento in atto in una

ancora oggi, nel 2021, l'Italia resta un Paese tristemente spaccato a metà, con un divario tra Nord e Sud divenuto sempre più ampio ed evidente nell'attuale momento di grave crisi sanitaria ed economica che tutti stiamo vivendo. In questo contesto, il Documento di economia e finanza non solo si configura come un importante strumento per rilanciare l'economia, ma può anche essere la cornice per iniziare a colmare lo storico *gap* tra le due Italie e per permettere di mettere concretamente il Mezzogiorno al centro di un quadro di sviluppo e di crescita nazionale. Il Sud ha bisogno di investimenti seri e di lavoro, non di misure assistenziali. Noi vorremmo che il reddito di cittadinanza si trasformasse in reddito di lavoro. Il Sud ha bisogno di interventi finalizzati soprattutto ad un vitale protagonismo delle giovani generazioni. Un capitale prezioso che purtroppo è andato perdendosi nel corso degli anni: ragazze e ragazzi costretti ad emigrare per trovare delle opportunità e spazi di affermazione. Occupazione, maggiore partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro, sanità, servizi essenziali, scuola, pubblica amministrazione e infrastrutture sono solo alcune delle priorità che devono accompagnare le misure che il Governo intende mettere in atto per il Mezzogiorno d'Italia. È necessario pertanto un progetto solido e di medio periodo, con azioni mirate e precise tese allo sviluppo del Mezzogiorno attraverso una serie di opere strategiche. Mi riferisco per esempio all'Alta velocità, con la realizzazione delle infrastrutture necessarie a dare una piena omogeneità nei collegamenti. Ma penso anche alla messa in sicurezza di strade e autostrade, al porto di Gioia Tauro, scalo centrale del Mediterraneo, e ad interventi per potenziare le aree produttive, il turismo, il commercio, l'imprenditorialità. Solo attivando le risorse di ciascun territorio e scommettendo sulla coesione e solo investendo sul capitale umano, riportando al Sud i cervelli che abbiamo perso, si può sperare di rilanciare la nostra Nazione. È evidente allora che c'è bisogno di un nuovo scenario economico anche per il Mezzogiorno d'Italia, con le medesime opportunità e le stesse prospettive di sviluppo dati al Centro-Nord. L'Italia cresce solo se cresce il Sud: lo stesso presidente Draghi lo disse da governatore della Banca d'Italia. senza il traino del Mezzogiorno il nostro Paese continuerà ad arretrare rispetto all'Europa e al resto del mondo. Concludo il mio intervento. Per raggiungere questi obiettivi, i sindaci del Sud hanno dato vinta alla Rete del *recovery* Sud: ci ritroveremo il 25 aprile a Napoli, città medaglia d'oro al valor militare per la lotta al nazifascismo, per chiedere con forza che al Sud sia dato quello che spetta al Sud, sperando che questa ricorrenza sia anche la festa della liberazione dalle divisioni del Paese, con una parte dell'Italia che avanza e con un'altra che arretra, e sperando che i cittadini del Sud siano pienamente considerati cittadini italiani, con gli stessi diritti e gli stessi doveri che ci rendono e ci fanno sentire i figli di un'unica Nazione, l'Italia. Governo, onorevoli colleghi, dall'analisi del DEF emerge la necessità e l'urgenza di mettere in campo politiche di rilancio per il Paese, considerando non solo misure tampone, ma misure strutturali. Lo scenario macroeconomico dell'economia italiana resta soggetto a diversi fattori di incertezza e le risorse dei vari scostamenti e del Next generation EU devono essere utilizzate per rimettere il Paese nella condizione di riprendersi e innovarsi, per non correre il rischio di rimanere indietro rispetto agli altri Paesi, europei e non. Quindi la sfida che abbiamo di fronte è quella di far ripartire il Paese nel più breve tempo possibile. importante e forte impatto per un ritorno alla normalità sarà sicuramente dato dalla necessità che la campagna vaccinale possa svolgersi senza troppe problematiche, arrivando al più presto all'immunità di gregge. I vari rappresentanti delle categorie, che abbiamo audito, hanno tutti evidenziato la gravità della situazione e il fatto che le risorse stanziate dai vari decreti-legge ristori e sostegni sono insufficienti. Siamo al settimo scostamento di bilancio: ciò significa che vi è continuamente la necessità di liquidità per le imprese. A questo si aggiunge la necessità di migliorare ulteriormente i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, garantendo il pagamento dello *stock* di debito pubblico. Non basta la liquidità, se non viene affiancata dalle riforme urgenti e necessarie, *in primis* quelle della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco, altrimenti le risorse stanziate per gli investimenti rischiano di non sortire gli effetti sperati. Ad acuire ulteriormente le criticità, si sono aggiunti la difficoltà di reperimento delle materie prime e l'aumento dei costi delle stesse. Paradossalmente alcuni settori si trovano con le commesse che non possono essere erogate per questo ulteriore fenomeno. Uno dei settori trainanti e più colpiti durante questa pandemia è sicuramente quello del turismo, che, come sappiamo bene, pesa per il 13 per cento del PIL. L'ultimo aggiornamento del quadro dei danni lo ha fatto Confturismo-Confcommercio: dal primo marzo a fine maggio si stima che nelle strutture ricettive ci sarà un calo di oltre 31,6 milioni di presenze, con una perdita stimata di 7,4 miliardi di euro. Per l'anno 2020, l'Italia ha avuto 219 milioni di presenze in meno, con gravissime conseguenze sull'occupazione. Tante imprese hanno chiuso e non riapriranno e tante stanno svendendo le loro attività, frutto del lavoro di una vita. Il rischio maggiore è che dall'estero si venga a fare acquisti dei nostri marchi storici e delle nostre aziende. Ad aprile 2021 la percentuale di imprese fortemente a rischio di usura, che hanno subito pressione per vendere le proprie aziende, è del 12 per cento e sono a rischio usura 36.000 piccole aziende del commercio, alloggi e pubblici esercizi. Questo emerge da un'analisi recente di Confcommercio. Per questo serve sostenere in maniera forte il comparto, prevedendo ristori adeguati, inclusivi e tempestivi col prossimo decreto, prevedendo moratorie creditizie e fiscali e misure per le locazioni commerciali. Servono interventi urgenti per dare più liquidità a questo sistema. Rendere le imprese forti e salde, con prospettive future, permette di richiamare coloro che momentaneamente non hanno un lavoro, hanno finito l'assegno di disoccupazione o sono in cassa integrazione. L'incremento ulteriore di posti di lavoro persi è di un milione, l'incidenza della povertà cresce, sia in termini di nuclei familiari, che in termini di individui, che salgono a 5,6 milioni. Anche qui poi l'analisi sulla difficoltà, che riguarda le varie strutture familiari, si diversifica tra famiglie più o meno numerose. È evidente che l'incertezza economica influisce negativamente anche sulle politiche di natalità che si vogliono mettere in atto. Concludendo, sicuramente la pandemia ha colto impreparata la nostra Nazione e ha evidenziato le carenze strutturali causate dalle scelte politiche passate e le criticità, che sono più evidenti se facciamo paragoni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Questo ulteriore scostamento di bilancio dovrà essere accompagnato dalla riapertura delle attività e da un ritorno alla normalità, che come Lega auspichiamo avvenga al più presto. L'estate è alle porte e serve urgentemente una programmazione certa, con linee guida e protocolli, ma soprattutto coordinamento, affinché il turismo possa ripartire evitando corsie preferenziali nelle località estere. Il comparto è a forte rischio, con ricadute sull'intera filiera, e di conseguenza sulle casse dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, con relative difficoltà poi a sostenere i costi dei servizi da erogare ai cittadini. È evidente che le vaccinazioni e le riaperture sono gli ingredienti fondamentali per riappropriarsi del nostro futuro *(Applausi)*. PRESIDENTE.

i dati programmatici del DEF ci dicono che alla fine del periodo di programmazione il tasso di disoccupazione scenderà, ma per attestarsi all'8 per cento l'occupazione, che ha segnato un calo del 10,3 per cento nel 2020, crescerà con percentuali sovrapponibili a quelle del rimbalzo stimato del PIL, ma si attesterà sempre al 4-5 per cento ogni anno e non riuscirà a recuperare il numero di occupati precedenti la crisi nemmeno alla fine del periodo di programmazione. Si tratta, in termini numerici, di 2 milioni di persone che resteranno fuori dal mondo del lavoro ancora nel 2024. Confindustria ha evidenziato come l'Italia registri un livello più basso della media europea in spese per politiche attive, mentre vede una spesa più alta in politiche passive. Bisogna quindi improntare le nostre politiche in materia di lavoro ad una maggiore occupabilità dei lavoratori.

non si può guardare solo a quanto succede in Italia, ma anche a cosa avviene negli altri Paesi e questo ci obbliga a colmare lo *skill gap* che si è generato creando un aumento spaventoso dei disoccupati, ma anche degli inattivi e di coloro che non cercano lavoro. numeri ci hanno posto di fronte alla necessità di guardare al lavoro e soprattutto al capitale umano con occhi prospettici. Le persone, non solo gli investimenti e le aziende, dovranno essere i protagonisti sia della transizione ecologica che di quella digitale, e per farle partecipare a queste due grandi transizioni è necessario formarle, quindi è necessario prepararle a quelle nuove professionalità che richiedono le attività che saranno generate sia dai capitali provenienti dall'Europa sia della programmazione economica di questo Documento di economia e finanza. Per questo riteniamo che gli investimenti debbano avere come obiettivo prevalente il capitale umano, cioè la formazione permanente per ampliare le competenze e l'educazione delle imprese e dei lavoratori. In quello che è stato definito debito buono ci deve essere quello impegnato per formare in modo più puntuale i nostri giovani, ma anche per riqualificare con nuove competenze coloro che sono già nel mondo del lavoro e che vogliono e possono partecipare a questa grande e straordinaria fase di transizione. Dall'inizio della pandemia si sono impegnate, e parzialmente spese, risorse, tra politiche attive e passive, pari al contenuto economico del PNRR, ora è necessario impegnare le risorse disponibili in modo sapiente. Un tema imprescindibile per uscire dalla crisi, e che sono sicuro assumerà sempre più importanza, è la valorizzazione del capitale umano su larga scala, impegnando risorse nella formazione. A beneficiare dell'aumento di valore del capitale umano, a tutti i livelli, sono le stesse aziende che, come ha dimostrato un recente studio di McKinsey, quando vengono ritenute dagli investitori più dinamiche, vedono crescere il valore stesso della propria capitalizzazione. Per concludere questo breve intervento, ritengo che l'impegno assoluto del Governo e del Parlamento debba essere rivolto alle politiche attive del lavoro, indirizzate alla valorizzazione del capitale umano quale risorsa imprescindibile del futuro del nostro Paese e delle nostre imprese. Solo così - ritengo - si potrà colmare quel *deficit* che si è venuto a creare con la pandemia. Per guardare al futuro con occhi sicuramente più fiduciosi c'è necessità di interventi veramente incisivi sulla formazione. Presidente, credo che questo discorso abbia bisogno di tempo; non mi è stato concesso, ma ritornerò sul concetto del capitale umano quale

Signor Presidente, il testo del DEF approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 aprile conferma l'avvio di un piano di profonda revisione del sistema tributario italiano. Per quanto riguarda la riforma fiscale, si inizierà dalla seconda metà del 2021 e sarà una delle misure collegate all'attuazione del *recovery plan*. Il sistema fiscale italiano risulta essere ancora troppo complesso e iniquo per i contribuenti. Per questo motivo è necessaria una sua riforma organica con il contributo e l'impegno di tutte le forze politiche. Il DEF non entra nei particolari di quella che sarà la riforma fiscale a venire, anche perché il Governo attenderà il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef e il prezioso patrimonio di audizioni che le Commissioni congiunte finanze del Senato e della Camera hanno raccolto negli ultimi mesi nell'ambito della stessa indagine. Dall'indagine conoscitiva sulla riforma Irpef sono emersi alcuni punti di interesse, sui quali le forze politiche dovranno confrontarsi, tra cui il ruolo da dare all'imposta personale, redistributivo o *pro* crescita o entrambi contestualmente; la scelta del modello di imposta onnicomprensivo, quindi ricondurre tutte le forme di produzione di reddito al sistema progressivo oppure migliorare l'attuale sistema duale, magari semplificandolo e riducendo il numero di aliquote sostitutive che sono oggettivamente numerose. Ancora, la scelta dell'unità impositiva, quindi conservare l'attuale sistema di tassazione individuale o individuare, ad esempio, il nucleo familiare come soggetto passivo d'imposta. È necessario stabilire e stabilizzare le nuove regole in materia di imposta personale e in materia di imposta in generale; ma questo non basta. Stiamo assistendo a un cambio epocale determinato dall'uso della tecnologia e da come la stessa abbia cambiato il nostro modo di vivere. Questa rivoluzione sta avvenendo anche senza aver stravolto le regole. Sulla riforma fiscale occorre, quindi, tener conto di questo, ovvero del fatto che lo stravolgimento epocale che stiamo vivendo non si è determinato a causa di uno stravolgimento delle regole, ma a causa della nascita di nuovi strumenti tecnologici che ci hanno fatto declinare quelle vecchie regole in modo completamente nuovo, diverso (alcuni usano il termine «spettacolare»). Questo è il ragionamento che dovremmo traslare nella riforma fiscale. Le regole sono necessarie, ma non sono l'elemento più importante; e un eccesso di regole - lo abbiamo sperimentato - può alimentare ulteriore complessità e paradossalmente può alimentare proprio quelle distorsioni che si vorrebbero contrastare: l'elusione fiscale, l'evasione e la corruzione. Le regole, quindi, devono essere semplici e funzionali all'utilizzo virtuoso della tecnologia. La tecnologia deve essere resa facilmente fruibile e deve essere facile da usare, esattamente come le più comuni applicazioni che utilizziamo nella vita quotidiana e, cosa importante nel fisco, la tecnologia non deve essere utilizzata contro i cittadini e i contribuenti, con una logica punitiva che abbiamo visto non aver mai funzionato, ma deve essere utilizzata per i cittadini, per semplificare il nostro ruolo di contribuenti, vedere le nostre imposte calcolate in modo semplice e immediatamente misurabile. Questo anche per dare finalmente l'esatta e tangibile misura della pressione fiscale, per poter monitorare la nostra situazione fiscale in tempo reale, semplicemente guardando il cellulare che teniamo in mano. Ripeto, il nostro modo di vivere negli ultimi anni è cambiato perché sono cambiati gli strumenti, le *app*, non perché sono cambiate le regole. Nel parere al DEF espresso dalla Commissione finanze del Senato, tra le osservazioni, è emersa la necessità di implementare una infrastruttura digitale che garantisca la certificazione dei crediti d'imposta ed una loro ampia circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi, anche alla luce dell'introduzione del superbonus 110 per cento e degli altri crediti d'imposta cedibili, compresi quelli maturati dalle imprese per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle zone economiche speciali e quelli in beni strumentali. Ieri l'Istat ha certificato un fatto molto importante: la produzione nel settore delle costruzioni ha superato a febbraio il periodo pre-Covid, il superbonus e i bonus in edilizia e soprattutto la possibilità di cedere i crediti fiscali derivanti da questi bonus, nonostante il perdurare delle chiusure e della pandemia, nonostante la complessità tecnica dalle misura che ancora dobbiamo superare, stanno producendo i loro effetti concreti, si sono caricati un intero settore economico sulle spalle e lo stanno portando fuori dalla crisi. I cittadini intendono occuparsi del bene più prezioso che hanno, la propria casa, e lo vogliono fare declinando la vera transizione ecologica, vorrebbero cioè rendere la propria casa completamente autonoma dal punto di vista energetico e alimentare i propri bisogni energetici con la luce del sole. Dallo studio della Luiss Business School e da OpenEconomics, uno studio rilanciato il 10 marzo dal Dipartimento politiche economiche di Palazzo Chigi, è emerso che il superbonus porterebbe nel lungo periodo un effetto positivo sui conti pubblici, considerando il gettito aggiuntivo dell'IVA e dell'Ires ottenuto per effetto degli investimenti indotti dal superbonus, quindi effetti positivi sulla crescita economica con ritorno positivo anche per le casse dello Stato. Del resto, già a dicembre del 2019 l'ufficio studi della Camera, in collaborazione con Cresme, aveva fatto emergere come gli incentivi per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nel ventennio 1998-2019, considerando tutto il gettito prodotto dallo stimolo all'economia in termini di IVA, Irpef, IRAP e oneri sociali, abbiano prodotto un saldo positivo di poco meno di 8,7 miliardi di euro. Chiedo, servono altre prove; le timidezze e i tentennamenti che si intuiscono, provenienti da qualche struttura ministeriale appaiono del tutto incomprensibili: il superbonus non deve essere brutalmente e banalmente degradato a mera spesa improduttiva, dobbiamo renderci conto che coniugando la cessione dei crediti fiscali con l'efficientamento energetico, con il bene più prezioso che abbiamo, la nostra casa, e con il settore delle costruzioni, abbiamo imboccato la strada giusta da seguire, dobbiamo solo darle una sistemata, renderla magari più sicura, ma quella è la strada che ci porterà fuori dalla crisi economica. *(Applausi)*.

col segnalare quanto già anticipato dal senatore Calandrini nella relazione di minoranza a questo provvedimento: il Documento di economia e finanza arriva sostanzialmente monco,

qui non li troviamo, non c'è alcun allegato, si è persa la possibilità addirittura di allegare a questo Documento il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come noi chiediamo da mesi ormai. Lo abbiamo fatto in tutti i modi, lo ha fatto la nostra *leader*, lo abbiamo fatto in Commissione, l'hanno fatto i Capigruppo alla Camera e al Senato, credendo fosse fondamentale riuscire a discutere di questo tema prima del 30 aprile, data ultima entro la quale il nostro

che l'Europa ha già bocciato con un sorriso, dicendoci di tornare a settembre, come quando un alunno è poco preparato ma ci prova lo stesso. È drammatico, perché in questo momento avremmo voluto poter discutere del tema, invece questo PNRR è rimasto nei cassetti di Città della Pieve e probabilmente arriverà l'ultimo giorno utile, di modo che questa fastidiosa opposizione che mette a nudo tutte le criticità di questa amplissima maggioranza non possa esprimersi sul merito e nemmeno sul metodo. Questa è la prima denuncia che facciamo da questi scranni perché - lo abbiamo detto il giorno dell'insediamento del Governo Draghi - noi saremo molto più leali di gran parte della vostra maggioranza e in questi giorni ce ne stiamo rendendo conto. Noi diciamo la stessa cosa da sempre; non abbiamo mai cambiato idea e gli italiani cominciano a riconoscerci questa coerenza, che non è strumentale ad aumentare la nostra È semplicemente il metodo che ci siamo dati senza chiedere nulla in cambio per essere utili a questa nazione e continuiamo su tale solco, convinti, come siamo, che paghi. Capisco però che, a volte, i lavori parlamentari siano interpretati come una rottura di scatole e capisco che, quando la maggioranza è talmente ampia, la minoranza è trattata come un qualcosa che, se non ci fosse, sarebbe meglio, in barba a qualsiasi tipo di democrazia nel mondo. Ricordo che non esiste nessuna democrazia dove non esiste opposizione, anche se qui parrebbe così. Gli appelli all'unità nazionale devono essere assolutamente accolti, altrimenti chi non li accoglie, secondo i vostri *standard*, diventa un alieno, qualcuno che non ha nulla a che fare con la democrazia. Invece, la democrazia risiede proprio in questi banchi. Sono questi i banchi che rappresentano la democrazia, perché quelli rappresentano il Governo

Ricordo a tutti che abbiamo già votato un *recovery* *fund* perché con la votazione dello scostamento di oggi sono 200 miliardi che questo Governo ha avuto a disposizione per cambiare le sorti di questa nazione.

uno studio della CGIA di Mestre - non occorreva nemmeno che voi portaste il DEF per capirlo - solo il 4,5 per cento dei fatturati delle imprese sono stati ristorati con le vostre operazioni e con i 200 miliardi che avete chiesto alle generazioni future. Alla faccia della sostenibilità! Aprendo una parentesi sulla sostenibilità e ricordando che oggi è la giornata mondiale della terra,

distratti nel momento in cui atti come il Protocollo di Kyoto andrebbero discussi oggi. Ripeto: è un atteggiamento che ormai vi riconosciamo e che ci rendiamo conto essere così. Detto questo, anche questa volta, con assoluta e massima responsabilità, che ci ha sempre mosso, voteremo magari lo scostamento, metteremo a disposizione ulteriori risorse, convinti e sperando che le tante proposte che Fratelli d'Italia ha fatto per una volta vengano accolte.

15 aprile ha approvato il nuovo Documento di economia e finanza che prevede un ulteriore scostamento di bilancio di altri 40 miliardi. nelle precedenti occasioni, come Gruppo parlamentare, abbiamo espresso con chiarezza e coerenza la nostra linea politica. Per sconfiggere oggi la pandemia e fronteggiare questa grave crisi economica è necessario fare sicuramente debito, a patto però - lo abbiamo ribadito più volte - che si tratti di debito buono e indirizzato nella maggior parte a investimenti e, soprattutto,

ha sempre tenuto. Nella lotta al virus siamo oggi a una linea di svolta, possiamo dirlo, perché a livello internazionale e nazionale è partita con grande forza la campagna vaccinale, tant'è che tutte le riviste e tutti gli scienziati dicono che sicuramente in autunno avremo raggiunto l'immunità;

del nostro Paese è assolutamente sostenibile. È essenziale quindi lo stimolo alla crescita degli investimenti pubblici, con interventi che operino il necessario rafforzamento delle infrastrutture del nostro Paese. Si va proprio nella direzione che noi sosteniamo da debito sì, ma debito buono e finalizzato agli investimenti che hanno un effetto espansivo e moltiplicatore sull'economia. La linea che viene tracciata e che è stata tracciata in questi mesi va anche nella nostra direzione. Le prospettive di ripresa e di crescita a breve termine sono fortemente condizionate dal successo della campagna vaccinale e dall'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'aspetto chiave è oggi l'accelerazione sul piano dei vaccini. Le Regioni in questo momento hanno hanno un ruolo molto delicato e importante, perché hanno delle tabelle di marcia per quanto riguarda il piano vaccini. Bisogna spingere anche da parte delle Regioni, tant'è che il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, lo ha ribadito e ha invitato le Regioni a dare una forte

al quale si aggiungerà nelle prossime settimane il decreto-legge sostegni due. In questo mese ci sarà un apporto di sostegno economico al Paese di ulteriori 70 miliardi di euro, che saranno importanti e vitali non soltanto per il sostegno all'economia, ma anche per il rilancio che in

un grande risparmio delle famiglie italiane. Quindi, c'è una importante massa di denaro data dal risparmio. Perché gli italiani in questo momento sono andati sulla strada del risparmio? Proprio per l'incertezza economica. Noi oggi dobbiamo cominciare a ripercorrere una strada, che è quella della fiducia. Solo attraverso la fiducia noi oggi possiamo riprenderci, utilizzando quel risparmio delle famiglie nei consumi, che è un fatto perché, attraverso un'azione forte sui consumi, possiamo riprendere in mano il Paese e, quindi, percorrere la strada della ripresa economica. Pertanto, è importante cominciare,

vi dico che c'entra moltissimo, perché salvaguardare la biodiversità, sempre più a rischio, e combattere il cambiamento climatico sono tra le sfide più importanti, che, se vinte, non fanno altro che salvaguardare la salute dei nostri cittadini. L'Europa in questi giorni ha raggiunto un accordo,

Se noi riusciamo a vincere questa sfida, riusciremo ad avere anche più salute. Quindi, è un tema importantissimo. Anche il DEF, che prevede una programmazione della politica economica e di bilancio del nostro Paese non può distaccarsi dai temi sanitari. Infatti, nella costruzione e nei cardini posti a sostegno del DEF, molto poggia sul tema poggia sul tema della sanità, come ad esempio la campagna di vaccinazione, della quale tutti stiamo parlando e che, per fortuna, si sta avvantaggiando grazie all'arrivo di ulteriori dosi. La campagna di vaccinazione, infatti, è uno dei temi sui quali punta anche il DEF. Addirittura, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha messo, tra i rischi delle previsioni economiche di breve e lungo termine, l'avanzamento della campagna vaccinale. Un aspetto chiave per la ripresa economica è legato anche alle riaperture.

delle case della comunità, l'assistenza domiciliare integrata, lo sviluppo delle cure intermedie mediante ospedali della comunità, interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, l'ammodernamento tecnologico e digitale: abbiamo sentito parlare tantissimo della telemedicina. Ancora, le cure tecnologiche avanzate e poi anche la ricerca sanitaria, nonché il trasferimento tecnologico e la formazione connessa alla suddetta ricerca. Sono tutti temi incentrati nella Missione 6, con fondi messi a disposizione. Ricordo che, nel Documento di economia e finanza, proprio per far diventare strutturali questi cambiamenti, vi sono anche collegate delle leggi delle leggi importanti. Una di questa è l'attuazione del patto della salute 2019-2021 per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Tra gli altri disegni di legge, richiamo alla nostra attenzione quello sull'attuazione dell'autonomia differenziata regionale, che in questo periodo, con tutte le diversificazioni di applicazione del sistema sanitario dal senatore Zanda, che ha fatto un discorso di altissimo rilievo,

Dobbiamo identificare precise responsabilità di chi avrà il compito di attuare i progetti, con tracciamento delle stesse e senza cadere nell'indeterminatezza e nella generalizzazione delle responsabilità, come purtroppo sempre accade. Anche su questo l'Europa si aspetta da noi, come Paese, uno scatto di maturità, visto che siamo abituati a non monitorare

dall'esigenza di dare discontinuità rispetto al precedente Governo Conte-*bis,* che si era manifestamente dimostrato incapace non solo di governare, ma ancor più di gestire l'emergenza coronavirus. Si tratta di una discontinuità che il presidente Draghi, insieme ai suoi Ministri, ha prontamente dimostrato con i fatti e negli atti, a cominciare dalla sostituzione del commissario per l'emergenza Arcuri e azzeccando la nomina del generale Figliuolo, i cui risultati si stanno vedendo in maniera visibile, giorno dopo giorno. La discontinuità si è vista anche quando ha cambiato il vertice della Protezione civile e quando, in maniera trasparente, ha deciso di affidare al prefetto Gabrielli i servizi segreti, al contrario di quanto aveva fatto Conte, che voleva tenerli per sé in maniera quasi gelosa. Ha segnato la discontinuità

con la spesa di ben 500 milioni di euro, che erano conservati in un cassetto, mentre le imprese del settore erano in sofferenza.

La discontinuità c'è stata anche quando sono state sbloccate 58 opere pubbliche per 66 miliardi di euro, con la nomina dei corrispondenti commissari. A proposito di opere pubbliche,

Speriamo che i responsabili vengano assicurati subito e con certezza alla giustizia. *(Applausi)*. Discontinuità c'è stata anche rispetto alle riaperture. È giusto infatti ricordare qui che, se si è parlato di zona gialla dal 26 aprile, è perché la Lega e Matteo Salvini hanno insistito in questi giorni e in queste settimane verso questa direzione; diversamente non avremmo avuto nemmeno la zona gialla dal 26 di aprile. A proposito di riaperture, bisogna dire candidamente che per le attività il vero sostegno, il sostegno auspicato, è la loro ripartenza. Dobbiamo fare in modo che, rispetto alle ideologie, prevalgano la responsabilità, la concretezza, nonché la volontà e l'indirizzo dell'Italia reale che sta sul territorio. Quello che oggi la Lega sta facendo è portare in seno al Governo la volontà dei sindaci, dei governatori - di destra, di sinistra, di centro - che spingono perché si apra il più possibile e il prima possibile. Discontinuità è anche questo scostamento, perché qualche settimana fa si parlava ancora di 20 miliardi. Matteo Salvini aveva detto che erano insufficienti, che avrebbe voluto almeno il doppio e abbiamo 40 miliardi di scostamento per le imprese, per le partite IVA. Adesso aspettiamo che a fine mese venga approvato il decreto sostegni-*bis*, in modo da dare subito risorse vere

ce ne sono per il 2021 altri 30 per le opere pubbliche, per mettere in piedi un piano parallelo al PNRR, con una previsione fino al 2023 di ben altri 70 miliardi di euro. È vero, il presidente Draghi ha lanciato la sfida e noi la raccogliamo. Questo scostamento significa la scommessa del debito buono, quello che serve a far crescere il Paese e che non deve essere soltanto visto nella cifra notevole e importante che lo caratterizza - per l'appunto 40 miliardi di euro ma, soprattutto, per il dopo. Se, infatti, sapremo spendere bene questi soldi e accompagnare queste risorse con riforme importanti nel nostro Paese, a cominciare dall'azzeramento del codice degli appalti, saremo in grado di rientrare di questo debito subito, bene e senza la necessità di attuare una manovra correttiva. Si diceva che questo è il tempo di dare i soldi agli italiani e non di prendere i soldi dagli italiani. È anche il tempo di liberare le risorse e non di vincolarle. A questo proposito, tanto per chiarire in quest'Aula, anche alla luce del dibattito di ieri, il Governo Conte non esiste più: non esiste più, è andato a casa perché incapace di gestire questa maledetta e brutta pandemia sotto ogni punto di vista, economico, sanitario e sociale. Facciamo chiarezza anche su un altro aspetto. Se arriveranno i soldi del PNRR, non è per merito di Conte, che non ha meriti, ma semplicemente perché l'attuale Governo, guidato da Draghi, sta lavorando in maniera assidua per recuperare i ritardi e i disastri che anche in questo ambito il Governo Conte ha fatto. Per concludere, perché la Lega è al Governo? Il nostro *leader* lo ha sempre detto in maniera chiara e candida: potevamo stare fuori ad aspettare che la nave affondasse, invece abbiamo deciso di starci per il bene dell'Italia, per l'interesse degli italiani. Vogliamo farlo, non per il gusto di governare o di annoverare qualche Ministro o qualche Sottosegretario in più, ma per determinare un'inversione di tendenza, per salvare il nostro Paese. Vogliamo farlo con responsabilità, con concretezza e con realismo. No, quindi, all'ideologia, a quell'ideologia che fa vedere sempre e comunque rosso; vogliamo farlo con coraggio, perché non vogliamo vivacchiare, ma vogliamo decidere. Vogliamo farlo

si inserisce in un quadro particolare. Infatti, accanto all'approvazione del Documento, autorizzeremo un margine ulteriore di scostamento di 40 miliardi di euro, che confluirà in un decreto-legge emergenziale, di prossima emanazione, il decreto sostegni-*bis*, che avrà un impatto in termini di indebitamento netto nel 2021, mentre l'impatto sul *deficit* degli anni successivi varierà fra 4 e 6,5 miliardi all'anno, volti soprattutto a finanziare investimenti pubblici con risorse aggiuntive a quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Proprio il PNRR contiene una specifica sezione dedicata alle riforme, coerentemente con il regolamento dell'Unione europea n. 2021/241, che integra così il programma nazionale di riforma, precedentemente inserito nel DEF, che ora invece si compone di sole due sezioni: il programma di stabilità e l'analisi e le tendenze della finanza pubblica. È chiaro che stiamo discutendo di un Documento, non di un testo di legge. Infatti, il contenuto del Documento di economia e finanza segue un *iter* preciso, non trovando un'applicazione concreta e immediata; però ha un'importanza fondamentale, perché rappresenta il punto di partenza di tutte le misure finanziarie ed economiche individuate dal Governo e proposte all'Europa. Leggendo il Documento è facile individuare la direzione verso il sostegno a famiglie e imprese e il rilancio, da garantire attraverso gli investimenti pubblici e privati. Con questo Documento si indica la strada economica e finanziaria che l'Italia deve intraprendere, si delineano gli obiettivi e le strategie a lungo termine, per una politica monetaria espansiva, da realizzare accrescendo il potenziale di sviluppo e rilanciando gli investimenti pubblici e, contemporaneamente, incentivando quelli privati nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, della digitalizzazione e soprattutto delle infrastrutture, materiali e immateriali. Buona parte delle risorse dello scostamento, infatti, sono destinate a sbloccare lavori sulle infrastrutture, per un valore complessivo di 66 miliardi di euro, ma non bastano, in assenza di validi progetti. È indubbio che sia necessario semplificare la normativa sulle opere pubbliche, con un lavoro che sia parlamentare prima che del Governo, evitando - come purtroppo sta accadendo la nomina di troppe commissioni tecniche e teoriche, molto spesso avulse dalla realtà pratica, dai territori e dalle stesse imprese, le cui esigenze, ora più che mai, devono essere tenute nella giusta considerazione per consentire un effettivo sostegno, che non sia pura assistenza, ma permetta la tutela del lavoro di qualità e il mantenimento dei livelli occupazionali.

che consentiranno il potenziamento anche delle assunzioni nel settore, e conferma la volontà di attuare la semplificazione delle procedure e migliorare la *governance* del piano di rilancio infrastrutturale. Rilanciare quindi gli investimenti per le opere pubbliche e sbloccare risorse importanti è un segnale forte di voglia di ripresa, che non si può ignorare. È vero che la crisi pandemica ha sconvolto il quadro economico e sociale mondiale, ma non si può negare che l'Italia retto lo scossone determinato da questo sconvolgimento grazie ai sacrifici di tutti gli italiani, che ringrazio a nome di Italia Viva. In particolar modo, ringrazio gli imprenditori, gli autonomi, le partite IVA e i professionisti che hanno faticato, molto più di altri, a rispettare regole e decisioni legittime e necessarie, dettate dalla protezione della salute, ma penalizzati molto più di chi, grazie ai provvedimenti assistenziali esistenti, ha continuato a sopravvivere, in una condizione certamente difficile, ma stabile nel complesso, perché fondamentalmente uguale a quella precedente la pandemia. È urgente, colleghi, attuare riforme per una politica fiscale efficiente, in grado di calibrare gli interventi per compensare difficoltà così diverse e, nello stesso tempo, rassicurare le famiglie, riducendo il desiderio di risparmiare per contrastare le incertezze. Non possiamo poi non riconoscere il significativo sostegno fornito dalla politica monetaria europea per gli interventi che hanno stabilizzato i mercati, evitando un inasprimento delle condizioni finanziarie; politica monetaria si è rafforzata insieme a quella di bilancio, intervenuta a difesa dei redditi del settore privato, consentendo alle banche di sostenere l'economia reale. La risposta comune da parte delle autorità europee e le opportunità offerte dalle politiche economiche espansive in atto costituiscono un valore da tener presente e da non vanificare, occorrendo invece dare continuità e fornire certezza al sistema economico. Ora dobbiamo aumentare gli investimenti produttivi, rilanciando per questa via l'economia europea, per dare stabilità a quella italiana e alla finanza pubblica, attraverso un impulso serio allo sviluppo e alla crescita. Solo così potremo riemergere dalla crisi con un'economia più forte e con un onere del debito più sostenibile.

insieme a molti colleghi ho fatto notare che col prossimo scostamento avremmo superato la barriera psicologica dei 200 miliardi; oggi è arrivato quel giorno. Vorrei ricordare che sono 400.000 miliardi di vecchie lire, così suona sicuramente in maniera più forte. Allora sgombriamo il campo: erano necessari quegli scostamenti? Assolutamente sì. Sono stati utilizzati al meglio delle possibilità? Assolutamente no. Come Lega, non ci siamo sottratti prima dall'opposizione e non lo stiamo facendo sicuramente oggi, convinti che non ci sia un debito di per sé sbagliato, negativo o cattivo, ma che dipenda da come le risorse vengono impiegate. Questo è il contributo che responsabilmente vorremmo dare, perché essere responsabili significa anche dire lealmente come la si pensa nell'interesse del Paese.

ai tempi e alle regole della ripartenza. È chiaro infatti che, per ogni settore che scegliamo di far ripartire, facciamo anche una scelta: possiamo risparmiare

conseguenza e un nesso causale fra le scelte sulle riaperture e l'impiego delle risorse attuali e di quelle che magari saranno ancora necessarie. È stato richiamato poco fa quello che ha detto il presidente Draghi sulla necessità di un rischio calcolato. Vogliamo che quel rischio calcolato, che tutti insieme stiamo decidendo di affrontare,

Poco fa il collega Misiani, al quale va riconosciuta l'onestà intellettuale, sostanzialmente ha detto due cose: la prima è che il decreto-legge sostegni

in una logica differente. Quel richiamo che egli mandava a questo pezzo di maggioranza lo estendiamo anche all'altro pezzo di maggioranza: siamo coerenti e facciamo esempi chiari.

Allo stesso modo, viviamo in un Paese che parla di far ripartire le fiere, i teatri e cinema, ma non è che il cinema al chiuso, a debita distanza, in una sala cinematografica, che era giusto far ripartire, sia diverso

e fare in modo che quel futuro, che vorremmo tutelare per noi e per i nostri figli e che vorremmo costruire con una ripartenza, non avrà fisicamente nessuno a viverlo, né in termini di aziende, che chiuderanno ben prima, non avendo comunque le risorse sufficienti a rimanere in piedi per altri mesi e altri anni, né in termini di cittadini, perché permettetemi di dire che anche da questo passa

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati ad esprimerci sul DEF 2021, in un contesto sanitario ed economico molto difficile. Il documento di economia e finanza è il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che delinea, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche. È opportuno sottolineare che la Commissione europea ha stabilito una clausola per meglio coordinare le politiche di bilancio volte a garantire agli Stati membri un maggiore spazio di manovra, per sostenere spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemica e le misure per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee, causati dalla diffusione del Covid-19. In futuro è ormai sempre più chiaro che le assurde impalcature finanziarie alla base del Patto di stabilità e del *fiscal compact* non potranno più riproporsi, per come le abbiamo conosciute finora. Il DEF 2021 è privo del Programma nazionale di riforma (PNR), in quanto in questa fase delicata il Piano nazionale di ripresa e di resilienza integra il programma di riforma previsto dai regolamenti europei e dalle norme nazionali. Nella giornata odierna siamo chiamati anche a esprimerci attraverso la votazione sullo scostamento di bilancio e quindi sull'indebitamento per ulteriori 40 miliardi di euro, nell'anno 2021. Il Governo richiede inoltre l'autorizzazione, per 6 miliardi di euro annui, per il periodo che va dal 2022 al 2033, finalizzati a finanziare spese per investimenti pubblici *extra* PNRR. Il nuovo scostamento da 40 miliardi di euro sarà utilizzato per un nuovo provvedimento di sostegno all'economia e alle imprese. In particolare, il sostegno economico sarà indirizzato al sostentamento dei lavoratori autonomi e delle imprese più colpite dalle restrizioni adottate per contenere il contagio. Dobbiamo essere fortemente consapevoli del rischio che il nostro Paese ha corso e, allo stesso tempo, della quantità e della qualità dello sforzo profuso, a partire dal Governo Conte II, l'Esecutivo che ha posto le basi e gli schemi per tutti gli interventi odierni. Attraverso la lettura del DEF non possiamo che renderci conto della qualità e quantità dello sforzo messo in campo dal secondo Governo Conte e da ultimo dall'attuale Esecutivo. Dal decreto-legge cura Italia del marzo 2020 all'imminente decreto sostegni *bis* sono state recuperate risorse fresche per più di 200 miliardi di euro, attraverso gli scostamenti di bilancio di volta in volta votati dal Parlamento. Dallo stesso DEF, inoltre, constatiamo che il PNRR italiano da qui al 2026 metterà in campo 237 miliardi di euro, comprensivi del PNRR vero e proprio, dei fondi aggiuntivi per finanziare investimenti *extra* PNRR e dei fondi React-EU. Il combinato disposto di risorse interne ed europee porta quindi il conto finale di quelle reperite per proteggere cittadini, famiglie e imprese e per rilanciare il Paese con investimenti *green* e digitali intorno ai 450 miliardi di euro. Siamo consapevoli che il PNRR è uno degli strumenti fondamentali per programmare investimenti e interventi necessari al Paese, per rispondere alla crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da Covid-19; è doveroso ricordare allo stesso tempo l'importanza e l'urgenza di completare o innescare riforme quali quella della pubblica amministrazione, del fisco, della giustizia e del mercato del lavoro, che non sono complementari, ma un supporto fondamentale per garantire il successo del PNRR. Per ripartire, l'Italia necessita infatti di una pubblica amministrazione più moderna e funzionale (andrei oltre il termine "semplificazione"),

di spendere unicamente per creare valore per i cittadini e di farlo in modo sostenibile, sul piano sia finanziario sia ambientale. Pensiamo a una riforma fiscale che possa ristabilire un buon rapporto tra Stato e cittadini, creando un'intesa sana e collaborativa tra le parti, in grado di ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale, favorendo i pagamenti elettronici e riducendo i costi delle transazioni *cashless.* Il MoVimento 5 Stelle, già nella relazione delle Commissioni riunite 5a e 14a sul PNRR, è riuscito a far inserire una proposta molto innovativa, con l'avallo delle altre forze politiche, per immettere un'ingente massa di risorse finanziarie nell'economia. Mi riferisco all'implementazione di una piattaforma informatica per certificare e far circolare gli innumerevoli crediti d'imposta immessi nel sistema economico a partire dal superbonus e dagli altri *bonus* edilizi. crediti fiscali che, inseriti in autentici conti correnti fiscali, dobbiamo poter usare come mezzi di pagamento di beni e servizi. La stessa proposta era già stata recepita in un altro atto parlamentare, ovvero il documento finale dell'indagine conoscitiva sul superbonus svolta dalla Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Insisteremo senza sosta sul punto, perché la libera circolazione dei crediti d'imposta, fissata a partire dal superbonus, è un'opportunità enorme per rendere immediatamente fruibili i crediti d'imposta stessi e per mettere ingenti risorse in mano a cittadini e imprese. Parlare di moneta fiscale a tal proposito si può e si deve, a maggior ragione dopo la scelta del Governo Conte II e del Governo Draghi di puntare sulla circolazione e cessione dei crediti d'imposta. il MoVimento 5 Stelle è consapevole dell'impegno e della responsabilità richiesti per attuare le linee programmatiche riportate nel DEF. Conosciamo le difficoltà, le incertezze del momento e le richieste di aiuto che quotidianamente arrivano dai nostri cittadini, ma conosciamo soprattutto le opportunità. *(Applausi)*. Garantiremo pertanto il massimo impegno, collaborando con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, per raggiungere gli obiettivi e fornire risposte concrete nell'esclusivo interesse del Paese e dei suoi cittadini, certi che ce la faremo.

affrontare il documento più importante della politica economica del nostro Paese, il DEF, e lo scostamento di ben 40 miliardi, quindi oltre 200 miliardi, che saranno debito evidentemente, potranno essere riversati completamente nella nostra economia, che già era ferma anche prima della crisi pandemica

uno sviluppo equilibrato e continuativo verso il progresso, al pari degli altri Paesi europei. La pandemia è stata e continua a essere una tragedia. Il bilancio dei morti,

tutti scossi da questa ondata spaventosa, ma anche da tutti gli effetti psicologici, depressivi e ansiogeni che ne sono derivati. Di questa cosa ci dovremo occupare, soprattutto per i giovani e per i bambini che non sono potuti andare a scuola durante il *lockdown*, ma anche per gli anziani, che, impauriti, sono dovuti rimanere nelle loro case. Soprattutto dovremo dare risposte a tutte le categorie economiche alle quali non abbiamo ancora

Lo dovremo fare in un modo intelligente e con una tempistica assolutamente precisa. Questa mattina è uscita la bozza del *recovery* nella quale si parla della divisione dei compiti. Il MEF monitorerà e i Ministeri e gli enti locali attueranno gli investimenti e le riforme necessarie. La *governance* sarà a strutture operative direttamente responsabili per realizzare nei tempi quanto previsto. Le tre parole che possono essere usate come *slogan* saranno monitoraggio, rendicontazione e trasparenza.

limitato - se n'è discusso ieri in Commissione bilancio - e sarà inferiore a quello auspicabile.

molte cose, ma dovremmo aver riformato la pubblica amministrazione e la giustizia. Questi temi costituiscono priorità da decenni e quindi occorre trovare un modo perché ciò avvenga. Tali riforme avverranno solo grazie a una presa di coscienza da parte di tutti

Non si fa così: non si rilancia un Paese completamente, com'è necessario, stando fermi oppure cercando di schivare le responsabilità; questo non può esistere. Faccio un esempio, perché poi non ci sono altre persone che legiferano, ma siamo noi e il Governo. Stiamo dicendo che occorre semplificare

le generazioni più giovani, avranno questo fardello da portare avanti e dovranno restituire queste risorse, quindi non possiamo sbagliare. Ieri in Commissione dicevo che bisogna bruciare le navi,

Questo è chiaro a tutti i livelli: non possiamo sbagliare noi qua, ma non possono sbagliare neanche nei Ministeri o negli enti attuatori e locali. Non possiamo sbagliare. Vi dico una cosa che mi è capitata qualche giorno fa nel mio Comune. Sapete che la piattaforma dell'INPS, parlando di reddito di cittadinanza, non dialoga con quella dei centri per l'impiego? Vi sembra possibile? Abbiamo da da correre e da lavorare tutti come matti, perché, se abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione efficiente, non possiamo che fare così. Lo dico a me stessa, ma direi che è un problema centrale. La motivazione è che o si fa così o andiamo alla malora e sinceramente non voglio essere quella che scarica la responsabilità su qualcun altro. Mettiamoci tutti di buona lena. di buona lena. Adesso vorrei parlarvi del problema turismo e di un aspetto che mi ha molto preoccupato. L'ambasciatore americano a Roma

«riaperture con rispetto regole e sicurezza (...) con senso di responsabilità dei cittadini cittadini sfibrati, noi in strada con comprensione (...) verso chi esercita pacificamente le proprie prerogative democratiche (...) hanno subito perdite importantissime delle proprie libertà individuali». Quindi, il Capo della polizia, non la senatrice Erica Rivolta della Lega, sta dicendo che c'è questa sofferenza grandissima.

la prudenza, le misure di sicurezza, bisogna fare in modo di riaprire il prima possibile, altrimenti queste realtà saranno morte per sempre. Sottolineo un altro punto. L'industria del turismo è la prima che può ripartire in tempi brevi, perché, appena sarà possibile il movimento tra le Regioni e con gli altri Paesi, i turisti (tranne quelli americani, a meno che l'ambasciatore non cambi idea) continueranno a venire nel nostro Paese, perché è unico e solo noi possiamo offrire la qualità dei servizi, la bellezza dei luoghi, l'importanza dei monumenti. Questo settore va assolutamente supportato,

Signor Presidente, signor Sottosegretario, innanzitutto mi permetta di esprimere il mio apprezzamento per la sua presenza. Devo dire la verità: questa mattina abbiamo avuto nostalgia di un esponente del Governo e del MEF. Abbiamo avuto il piacere della presenza della Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, ma è importante che una persona competente e autorevole come lei sia oggi qui in Aula, soprattutto per rispetto all'opposizione. In questo clima di concordia nazionale, cui noi abbiamo dato un nostro contributo, è importante che tutti possano parlare ai soggetti interessati, in questo caso al MEF. Quindi, grazie, sottosegretario Durigon. Signor Sottosegretario, questo è un DEF molto ambizioso ed è anche pieno di ottimismo. I numeri ce li ha raccontati in sede di Commissioni congiunte il ministro Franco. Negli investimenti si prevede, per il prossimo triennio, un incremento del 3,2 per cento. Ciò significa riportare il livello degli investimenti al periodo precedente alla bolla finanziaria Lehman Brothers del 2008-2009. Si parla di una crescita del PIL addirittura del 4 per cento per il 2022, il che significa riportare il livello del PIL a quello precedente allo scoppio di questa pandemia. Noi, signor Sottosegretario, condividiamo lo spirito di questo DEF, ne apprezziamo alcuni spunti, ma non possiamo evitare di esprimere alcuni dubbi e alcune perplessità. La domanda centrale è come come realizzare i punti previsti, gli obiettivi previsti ed indicati nel DEF, affinché non diventino carta straccia o un libro bianco dei sogni. Ebbene, signor Sottosegretario, noi oggi vogliamo darle dei suggerimenti per garantire un'autentica crescita poderosa. la crescita poderosa non la si può fare senza riforme strutturali, come hanno detto diversi colleghi prima di me. Se, infatti, vogliamo garantire una ripresa della competitività, dobbiamo avere il coraggio di porre in essere le famose riforme che attendiamo da trent'anni. Per titoli, vorrei partire dalla burocrazia. Lo ha detto molto bene la collega Rivolta: digitalizzazione e, come ha spiegato il ministro Brunetta, snellimento delle procedure. Troppi nulla osta, troppi uffici, troppi funzionari che interagiscono si sovrappongono nelle varie procedure. Questo complica la situazione. Pochi giorni fa parlavo con un imprenditore del settore edilizio che, per l'abbattimento di una struttura abbandonata da trent'anni

anche per l'assunzione di responsabilità degli enti locali. I sindaci non firmano più nulla, perché hanno paura che il giorno dopo, qualunque provvedimento loro adottino, venga bloccato dalla procura, con conseguenze giudiziarie importanti. Il secondo settore, sottosegretario Durigon, sono gli investimenti. Dobbiamo dirlo a chiare lettere: se lei oggi avesse un capitale e volesse investire nel suo Paese, cioè in Italia, lei lo farebbe? Io penso che ci voglia coraggio e fiducia e che lo Stato debba darli, soprattutto ai fondi stranieri che vogliono entrare in Italia a investire e non solo sugli *asset* strategici, ma anche sugli altri. Tutti i *report* delle agenzie, pubbliche e private, dicono che noi dobbiamo intervenire sulla legge fallimentare. infatti, un fondo straniero vuole investire su diversi *asset*, se salta uno dei suoi progetti, saltano a catena tutti gli altri. In America esiste *Chapter* 11,

una delle 126 procure della Repubblica, legittimamente e in piena autonomia, può alzarsi e dire la sua. Lei si renderà sicuramente conto che rispetto agli altri Paesi questo non è attrattivo e che i fondi stranieri hanno paura a venire in Italia non perché non vi sia certezza del diritto, ma perché non vi è chiarezza delle norme, che si complicano e intersecano tra loro.

Bisogna insistere su questo, nonché sul rinnovamento e sulla ristrutturazione dei centri per l'impiego. Il reddito di cittadinanza ha un valore sociale inclusivo? Sì. Sotto l'altro profilo (quello della politica attiva del lavoro) è invece del tutto carente, come ha detto poco fa la collega che mi ha preceduto.

abbiamo il più basso tasso di occupazione. Questi sono i numeri con cui interagiamo quotidianamente. Il nostro auspicio è che si vada veramente verso le riforme. Apprezziamo le parole del ministro Franco che in Commissione ci ha detto che

di lottare contro il potere di interdizione degli interessi organizzati che spesso, purtroppo, hanno agito a discapito della crescita diffusa. *(Applausi)*.

Tutto è stato infatti rinviato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che però non è allegato. Sappiamo che tra pochi giorni il presidente del Consiglio Draghi lo dovrà consegnare in Europa e questo ci preoccupa molto. Ricordo che proprio in sede di discussione del PNRR Fratelli d'Italia aveva chiesto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza fosse allegato al DEF. Se così fosse stato, oggi avremmo avuto qualcosa di cui discutere. È invece evidente a tutti che senza PNR e PNRR stiamo parlando praticamente del nulla.

Si dà larga importanza, come era evidente che fosse, alle conseguenze dovute alla crisi pandemica, in particolare alle cosiddette seconde e terze ondate del Covid-19 e a tutti gli interventi che si sono resi necessari per il contenimento.

dopo la scorsa estate, ma il Governo Conte II non fece assolutamente niente. Fratelli d'Italia aveva presentato emendamenti, aveva detto più volte che era necessario intervenire prontamente, soprattutto dove

vero che ha sostituito il commissario Arcuri con il generale Figliulo e abbiamo certamente valutato positivamente questo cambio, ma su tutto il resto è andato e sta andando in assoluta continuità. Nel DEF c'è scritto che le speranze della ripresa economica in Italia sono tutte legate al piano vaccinale,

A questo proposito, dobbiamo sottolineare tutto il tempo che si è perso sul piano vaccinale, ed è costato non poco, molte vite umane. il tempo che ha perso il commissario Arcuri, che rincorreva le primule, i gazebi, presentandoci grafici in cui si vedevano queste primule meravigliose,

tenere colui che noi riteniamo sia l'artefice di questo grande disastro, sia sul piano vaccinale che sulla gestione della pandemia, vale a dire il ministro Speranza, che continua a rimanere al suo posto, continuando con la stessa ricetta,

assolutamente più aggressivo. Sentiamo dire che si deve ancora chiudere, chiudere e chiudere. Invece noi riteniamo che sarebbe fondamentale che questo Governo smettesse di parlare di chiusure, soprattutto per tutte

sembra aver raggiunto una forma di coesistenza col virus». «Si riscontra - prosegue il DEF - una maggiore resilienza dell'economia, verosimilmente riconducibile anche alla capacità di adattamento degli operatori, sia sul piano delle scelte produttive e organizzative che su quello Allora come mai in queste settimane abbiamo visto tanti operatori economici, tante tante persone che vivono - o, meglio, che vivevano - del proprio lavoro manifestare nelle piazze? Come mai, se in questo DEF è scritto che ormai il sistema produttivo ed economico ha trovato un modo di operare insieme al virus, che non è poi più così dannoso? *(Applausi)*. Ma vi siete resi conto? Ma avete visto le persone che stanno manifestando e che chiedono la cosa più dignitosa, più onesta

Ci dovete rispondere. Qual è la vostra *ratio*? su questo scostamento che avete chiesto ancora una volta faremo la nostra parte di patrioti, perché ci rendiamo conto che 40 miliardi di euro sono fondamentali per dare un sostegno alle categorie produttive. Certo,

volete aiutare il sistema produttivo o volete ancora dare mance, prebende e aiutare gli amici degli amici. Fratelli d'Italia vuole credere. Siamo patrioti, faremo la nostra parte, ma siamo molto preoccupati da ciò che è contenuto nel DEF. Siamo molto preoccupati di aver visto che, oltretutto, è aumentata la pressione fiscale nell'anno 2020, che è un'assurdità: non si lavora e siete anche capaci di aumentare

Senatore Airola, credo che tutta l'Assemblea sia assolutamente convinta della sua affermazione.

nei minuti che ho a disposizione voglio proporre due ragionamenti. Il primo è un percorso che può sembrare un esercizio astratto, ma che credo, invece, possa essere utile a mettere a fuoco non solo quello che è successo, ma anche, per quel che resta da fare, ciò che occorre operare con le risorse che mettiamo a disposizione con questo ulteriore scostamento di bilancio.

di questo evento inedito e tragico che ha colpito l'intero pianeta. Ma in questo anno dietro l'angolo non c'è mai stata la fine della pandemia.

turistica e una stagione invernale, un anno di esercizi pubblici sostanzialmente chiusi, ma sapendo anche quali sarebbero stati i settori che avrebbero potuto continuare a lavorare perché essenziali? Insomma, una valutazione preventiva ma complessiva, mettendo a fronte di questa una stima di quelle che sarebbero state le risorse necessarie per fare questa traversata nel deserto, e anche le risorse che ragionevolmente avremmo potuto mettere a disposizione attraverso degli scostamenti di bilancio per contenere i danni e le ricadute negative. I dati I dati sostanzialmente parlano in questi termini: per superare un anno, ovviamente non coprendo tutto quello che è mancato in termini di fatturato, ma salvaguardando la tenuta del Paese nel suo complesso, probabilmente servono - dico servono perché credo che questo conteggio sia valido tuttora - circa 450 miliardi, a fronte di una capacità straordinaria di indebitamento del Paese, che peraltro viene sorretta in questa straordinarietà anche dall'Europa, di 200 miliardi 200 miliardi di debito, che abbiamo fatto e che facciamo oggi concludendo questo *rally*, dopo un anno, considerando tutti gli scostamenti. Questi 200 miliardi come li avremmo utilizzati? A che cosa avremmo dato risposta? Quali sarebbero state le priorità se non fossimo stati costretti a inseguire la pandemia, mese per mese? state tre in modo particolare: la copertura dei costi fissi; il sostegno alla liquidità delle imprese; il sostegno della cassa integrazione. Sostanzialmente parlo del mantenimento della capacità produttiva attraverso il sostegno alla forza-lavoro e il mantenimento in essere degli *asset,* che determinano e sostengono la capacità di produrre del nostro Paese. Sì, probabilmente questo può apparire un ragionamento astratto fatto oggi, però credo ci aiuti a capire quali sono le risposte che dobbiamo dare con questo ultimo scostamento di 40 miliardi; le risposte che dobbiamo aprire e sulle quali ci dobbiamo concentrare per mantenere ancora la nostra capacità produttiva, sia riguardo agli *asset* sia riguardo alla forza lavoro. Lo ripeto: costi fissi e liquidità. Il secondo ragionamento che voglio fare è relativo alle riforme strutturali. Su questo voglio sottolineare incidentalmente il valore del grande patto di solidarietà che si è raggiunto in Europa tra le Nazioni, perché i Governi hanno compreso che l'Europa non è solamente un mercato interno, ma un sistema economico complesso con delle interdipendenze interne, che ha necessità di essere sorretto e aiutato per avere un'efficienza complessiva, avere un'efficienza complessiva, il che significa intervenire per ridurre le disomogeneità e quindi dare aiuti e sostegni in modo disomogeneo per andare a sostenere quei pezzi del sistema che ne determinano la debolezza complessiva. Questo spiega perché all'Italia viene assicurata dal Next generation EU la fetta più significativa di risorse. L'Europa inizia finalmente a ragionare come sistema sociale ed economico, non solo rivolto verso le regole del mercato interno, ma valutando la propria capacità di competere nei mercati internazionali. Parlo quindi di un'Europa che guarda complessivamente alle filiere produttive che sono presenti nel continente, che si confrontano con le altre filiere presenti nel mondo.

facendo anche dei passi inediti come l'istituzione dei titoli di debito europeo, seppur ancora circoscritti alla pandemia e non resi strutturali. In questo quadro ci vengono richieste le riforme. Al di là del fatto che in questo Documento manca il Piano nazionale delle riforme, che è sostituito dal PNRR, la sostanza c'è. Credo che la pagina 14 del DEF,

sulla semplificazione e sul riordino in materia di *start-up* e PMI innovative, sulla revisione organica degli incentivi alle imprese, sulle disposizioni per lo sviluppo delle filiere per favorire l'aggregazione tra imprese e per la revisione del decreto legislativo

Decidere i contenuti di quei collegati è il compito che ci aspetta, come Governo e come Parlamento, ma soprattutto come forze politiche. Diamo un'accelerata, per collocare l'Italia, nel dopo pandemia e nel dopo Covid, in un percorso di rilancio, non solo dell'Italia, ma dell'intera Europa.

mesi dallo scoppio della pandemia, l'economia della montagna è quella che ha pagato il prezzo più alto, per le restrizioni e le limitazioni. Mentre le località di mare, fortunatamente, hanno potuto godere della parentesi tra la prima e la seconda ondata e adesso si apprestano alla nuova stagione, grazie all'avanzamento della campagna vaccinale, la stagione sciistica è coincisa con le fasi più acute della diffusione del virus. In pratica nei nostri territori è saltata un'intera stagione, con impianti e alberghi chiusi e l'intero indotto che non ha potuto far lavorare un solo giorno tutti gli operatori. Come sappiamo, tutto questo ha avuto conseguenze pesanti per i lavoratori stagionali, comprese le professioni della montagna, come le guide alpine e i maestri di sci, che non sempre sono rientrati nelle tipologie di lavoratori che hanno avuto accesso alle varie forme di sostegno al reddito. Per questo, già in autunno, quando era ancora in carica il Governo precedente, avevamo sollecitato un'attenzione particolare ai nostri territori, che si è tradotta poi negli aiuti a fondo perduto per la filiera della neve, contenuti nel decreto sostegni, varato dal nuovo Governo Draghi. Ricordo che quelle misure furono concordate in una fase nella quale si credeva ancora che la stagione sciistica sarebbe potuta partire dopo il periodo natalizio. Per questo oggi non serve soltanto confermarle, nei provvedimenti che saranno finanziati con questo ulteriore scostamento di bilancio. Occorrono, da un lato, un sostanzioso rafforzamento di quelle risorse e, dall'altro, una revisione dei criteri per la quantificazione degli aiuti. In particolare è necessario trovare un meccanismo che calcoli la perdita reale, come abbiamo detto, pesa soprattutto per i mancati introiti del primo trimestre 2021. Siamo consapevoli dello sforzo che è stato fatto portando questo scostamento a 40 miliardi di euro. Dall'inizio della pandemia lo Stato si è indebitato per circa 175 miliardi di euro, ma non sempre queste risorse sono purtroppo riuscite a centrare l'obiettivo del sostegno alle imprese. A maggior ragione occorrono criteri che distribuiscano le risorse, in proporzione alle perdite effettivamente subite, ma oggi credo che occorra lavorare di più su proroghe e moratorie, per alleggerire le imprese e le famiglie dal carico fiscale e favorire così l'accesso al credito. È un tema di giustizia sociale, ma anche un tema di tenuta del tessuto produttivo nei territori di frontiera, che, non dimentichiamolo, si devono confrontare con la concorrenza e quindi anche con i regimi fiscali e gli aiuti che ricevono gli operatori economici dei Paesi confinanti. sempre nell'ottica, importante, che nella prossima legge di bilancio si intervenga sulla quota di compartecipazione delle Regioni e delle Province autonome al risanamento dei conti dello Stato. Con l'ultima legge di bilancio, per via delle minori entrate erariali, nella Valle d'Aosta ad esempio è stata lasciata in cassa parte consistente della quota di compartecipazione. Queste risorse sono state essenziali per garantire il funzionamento di tutta una serie di servizi che sono interamente a carico delle Regioni a statuto speciale, come la scuola, la sanità e la Protezione civile. Nel DEF che oggi ci accingiamo per tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome la quota indicata è di appena 100 milioni. È una cifra sicuramente insufficiente, quindi chiediamo che venga rinegoziata e rivista per continuare a garantire questi servizi essenziali. In conclusione, signor Presidente, vorrei fare una riflessione sulle riaperture.

Questo è un esempio ulteriore di come la realtà della montagna non sia ancora, dopo quattordici mesi di pandemia, presa nella giusta considerazione. È chiaro che un ristorante in una località montana non può far cenare i clienti all'aperto in questa stagione, a meno che questi non si accomodino con i cappotti, la sciarpa e i guanti, oppure si chieda ai ristoratori di dotarsi di stufe per riscaldare i *dehor.* Ma con che faccia, in un settore che è già in ginocchio? Per provvedimento chiederemo un'ulteriore attenzione alla realtà della montagna. Lo ripetiamo da mesi, ma le risorse dei provvedimenti fin qui messi in campo purtroppo non sono ancora sufficienti per salvare un intero settore turistico. Per questo anche la nostra Regione, seguendo l'esempio del Sud Tirolo, sta lavorando a un *pass* che consenta di fare attività anche negli nei luoghi chiusi. il mio auspicio è che ogni scelta tenga conto delle specificità, anche climatiche, dei diversi territori. La montagna ha sofferto più di tutti, dedichiamole l'attenzione che merita.

quello in esame è l'ennesimo scostamento di bilancio che ci apprestiamo a votare, ma in realtà a debito si aggiunge debito. Il grande debito pubblico italiano ha che fare con

Tutto questo determina un quadro a tinte fosche, con poca speranza (non mi riferisco al Ministro, passatemi la battuta).

in apparenza tecnico e neutro, intitolato «Sensitività rispetto alle variabili demografiche». Non so se i colleghi della Lega abbiano avuto modo di dare un'occhiata, però questo Ministro sostiene che far entrare più immigrati è un ottimo modo per ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL. Vi risparmio tutta la narrazione e le disquisizioni macroeconomiche; la conclusione è che l'incremento del flusso netto migratorio di un terzo rispetto al previsto

che non hanno accesso nemmeno alle case popolari in tanti dei nostri Comuni a causa di leggi inique. Perché non investire sulla natalità? Perché non investire su leggi che favoriscano la famiglia, sugli asili nido e su tantissime altre proposte che la destra italiana e i patrioti - lo voglio sottolineare - di Fratelli d'Italia sostengono da sempre? Ecco, riteniamo - lo dico ai rappresentanti del Governo - sia a dir poco vergognoso. Fratelli d'Italia si batterà con ogni mezzo per contrastare la deriva immigrazionista di questo Governo, che è perfettamente in linea con il Governo precedente. *(Applausi).* PRESIDENTE.

perché è richiesta - e il PNRR ce lo racconta molto bene - una radicale trasformazione del nostro Paese sul piano *green*, digitale, di coesione, delle competenze richieste agli italiani, e anche una grandissima sfida sul piano sanitario, che forse ancora stiamo parzialmente sottovalutando. La salute degli italiani è, infatti, il presupposto in base al quale può essere realizzato tutto quello che nel DEF stiamo raccontando. È per questo che come Italia Viva stiamo raccomandando, chiedendo, mettendo in atto un piano di investimento massiccio sulla sanità.

per riformare il fisco, la giustizia, la pubblica amministrazione, il mercato del lavoro. Non dobbiamo dimenticare che tutto questo avverrà nei prossimi cinque anni e che non toccherà solamente a noi.

e in particolare allo scostamento, la richiesta di scostamento - lo sappiamo - è stata resa possibile, come tutte le precedenti che abbiamo approvato quest'anno, dalla applicazione della clausola del "*general escape clause"*, che dà a tutti gli Stati europei quegli spazi di manovra per poter intervenire. L'Italia ha fatto molto per fronteggiare l'epidemia, compreso l'attuale scostamento; abbiamo investito 180 miliardi in interventi a favore della sanità, delle imprese, delle famiglie. Questi 180 miliardi 180 miliardi hanno aumentato il nostro debito, poi analizzeremo come potrà continuare ad essere sostenibile. I 40 miliardi che verranno autorizzati oggi con lo scostamento serviranno per le misure del decreto imprese, a favore, in particolare, delle delle imprese, sui costi fissi, per favorire il credito e la liquidità, ma anche per aiutare le famiglie più in difficoltà, per aiutare finalmente, come è nello spirito di questo nostro periodo e del Next generation EU, i giovani. L'Italia, come gli altri grandi Paesi europei, ha investito molto, secondo le stime del Fondo monetario internazionale, oltre l'11 per cento del PIL in misure di sostegno dell'economia. Il Fondo monetario internazionale ci tratteggia anche un quadro mondiale degli interventi che non sono esattamente comparabili con quelli europei, perché abbiamo due livelli di intervento, quelli nazionali e quelli europei, ma dobbiamo sapere che

perché ciò avverrà temporalmente dopo la reintroduzione del Patto di stabilità e crescita, che dovrebbe essere introdotto nel 2023 e che ci pone un altro obiettivo, quello che l'Italia deve avere primariamente, ovvero la revisione del Patto di stabilità e crescita. Il presente scostamento contiene anche una novità molto importante, che è l'ulteriore indebitamento netto di circa 6 miliardi nel periodo 2025-2034, che andranno a costituire il fondo di investimento complementare. il fondo di investimento complementare. Tale fondo finanzierà quei progetti interessanti e prioritari riproposti dalle amministrazioni dello Stato che però risultavano eccedere le misure complessive destinate all'Italia nel progetto Next generation EU.

delle risorse di altri fondi complementari, come React-EU, per 15 miliardi e appunto di queste ulteriori risorse pari a oltre 31 miliardi del fondo di investimento complementare. Da questo punto di vista, il PNRR, come deve, aiuta moltissimo il cuore di questo DEF, che è la crescita. Il PIL, soprattutto negli anni 2021-2022, risente molto positivamente dell'impatto delle misure di spinta del PNRR, incrementando anche rispetto ai tendenziali di +0,5, e attestandosi a livelli interessanti: il 4,5 per cento nel 2021 e il 4,8 per cento nel 2022. Sul 2022 dobbiamo dire che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sollevato qualche perplessità, ma comunque ci piace vedere questa

sul perché il PNRR non sia in grado di imprimere una crescita duratura, consistente e solida al nostro PIL. Il PIL è dirimente per quanto riguarda la sostenibilità del debito. Il rapporto debito-PIL

per assestarsi nell'orizzonte programmatico al 152,7 per cento, ma ci vorrà un decennio per arrivare ai livelli di debito del rapporto debito-PIL pre-crisi e ancora non basta, perché tutti noi ricordiamo i ragionamenti che facevamo in quest'Aula poco più di un anno e mezzo fa e sapendo benissimo che il nostro debito era già alto e al limite della sostenibilità prima della crisi.

agli scenari avversi, che esistono. Noi, oggi siamo pronti a sostenere questo sguardo in avanti e, però, dobbiamo contestualmente guardare con senso di realismo agli scenari

tuttavia, che non possiamo governare noi. Solo pensando alla pandemia sappiamo benissimo che ci sono rischi di nuove varianti, che il piano vaccinale prosegue spedito grazie al nuovo Governo, ma che abbiamo, comunque, dei problemi di approvvigionamento. E sappiamo anche benissimo due cose importanti: il patto di stabilità e crescita e i programmi di acquisto della BCE dal 2023 vedranno un altro approccio rispetto a quelli di sostegno che vediamo noi.

il percorso di vaccinazione e abbiamo un piano importante. Sappiamo che questo anno ha modificato radicalmente condizioni di vita, di salute, di futuro e di prospettiva. Ha cambiato non solo la convivenza

cento delle piccole imprese che rappresentano più del 20 per cento dell'occupazione strutturale è a rischio, soprattutto nel terziario e nelle filiere produttive molto esposte alla concorrenza internazionale. ci sono i temi del turismo e degli aspetti culturali di questo Paese. Dentro questa situazione percepiamo tutti - ogni senatrice, ogni senatore, ogni parlamentare, ma anche chi ha rappresentanza esterna

Voteremo il Documento di economia e finanza (DEF) votiamo lo scostamento per poter fare un intervento importante a sostegno delle imprese, del lavoro e delle professioni, con tutto ciò che ne deriva.

del PNRR alla fine di aprile, ma perché lì abbiamo determinato la nostra unità di Paese e la nostra visione

Allora noi dobbiamo sapere (ne siamo tutti consapevoli) che abbiamo un Paese in attesa di queste nostre scelte, in attesa di questo orientamento, in attesa della nostra coerenza in queste scelte.

a sottolineare un aspetto che questo Senato e questo Parlamento hanno conquistato nel dibattito e nella costruzione del *recovery plan*, che riguarda uno dei *gap* fondamentali di cui soffre il nostro Paese e che, se non affrontato, non ci metterà nella condizione di crescere e di rimettere al centro il lavoro con una piena occupazione di qualità: l'aumento dell'occupazione femminile. Non mi stancherò mai di dirlo, come tutte noi e tutti noi; lo abbiamo anche votato, ma bisogna rimetterlo al centro di questa scelta e non perché lo diciamo solo noi.

di risposta a ciò che questo anno di pandemia ha messo straordinariamente in visibilità per tutta la società, cioè dove sono collocate le donne nelle loro attività.

anche un altro asse di ragionamento, che c'entra con il fatto di mettere al centro l'obiettivo della piena e buona occupazione nel nostro Paese. Perché alla fine di cosa parliamo quando parliamo degli investimenti? Vogliamo creare lavoro di qualità. creare lavoro di qualità. Ma anche qui, per rispondere all'asse fondamentale e alla visione che ci ha dato il Next generation EU, c'è esattamente la filiera trasversale della conoscenza, senza la quale anche questo non attraversa assolutamente la messa a terra della transizione ecologica, della transizione digitale e di tutto il resto. Questo è l'altro elemento.

Noi abbiamo bisogno di due grandi scelte che dobbiamo fare insieme, Parlamento e Governo: dobbiamo davvero costruire un patto sociale e un patto istituzionale, perché abbiamo bisogno, per rilanciare il Paese, delle Regioni e dei Comuni. Abbiamo bisogno di questo e penso che ci faremo promotori insieme ad altri - me lo auguro e guardo la mia Capogruppo - del fatto di istituire una Commissione speciale bicamerale che accompagni e monitorizzi (oggi,

bicamerale è fondamentale da questo punto di vista, ma lo è soprattutto il patto di rilancio. Questo è un punto della politica, non è un guardare indietro a Ciampi, ma è guardare all'esigenza vera ed è anche l'auspicio per cui è nato questo Governo di emergenza, il Governo Draghi.

nel tempo assegnatomi cercherò di rappresentare il mio punto di vista sul Documento di economia e finanza e di rappresentare anche quelle che potrebbero essere, a mio avviso, le conseguenze della politica economica del Governo in cui si inserisce il DEF. Com'è noto, il DEF rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica. Per legge, questo importantissimo documento programmatorio deve essere accompagnato da determinati documenti e da tutte quelle misure che, in qualche modo, incidono sulle entrate o sulle uscite. Essendo, infatti, una stima che il Governo fa e che il Parlamento deve valutare su quello che sarà l'andamento del Paese dal punto di vista economico, ovviamente si deve basare su elementi che devono essere in qualche misura noti al Parlamento e, quindi, valutabili compiutamente. In particolare, per legge il DEF deve essere accompagnato dal Piano delle riforme, perché è ovvio che queste ultime possono incidere sulle minori uscite, così come deve essere accompagnato da tutte quelle norme e da quei provvedimenti rilevanti dal punto di vista delle entrate. In particolare, il DEF prevede e menziona esplicitamente la rilevanza del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tuttavia, di questo Piano non conosciamo nulla, se non ciò che abbiamo conosciuto dal precedente Governo: già di per sé era piuttosto fumoso e, comunque, questo Governo ha detto di volerlo cambiare in molte sue parti.

come avevamo chiesto? Personalmente, io ho lasciato agli atti la mia richiesta in Commissione, perché il Presidente della Commissione finanze si facesse promotore col Governo per avere un'anticipazione, le schede, i progetti per poter valutare compiutamente il DEF, ma nulla di tutto questo è stato fatto. Quindi, la domanda che segue immediatamente è: che cosa state nascondendo. Come mai l'attività, che sicuramente viene fatta dal Governo, viene fatta non alla luce del sole. Che cosa state nascondendo? Qual è il piano nascosto che cercate di portare più avanti possibile, senza che il Paese e il Parlamento lo conoscano. Per cercare di dare risposta a questa inquietante domanda e, e, quindi, venendo anche a quelle che possono essere le conseguenze della politica economica in cui si inserisce questo Documento di economia e finanza, vorrei entrare brevemente nel dettaglio di quello che si può comprendere anche senza la presenza di quegli importanti allegati di cui parlavo prima. In particolare,

l'obiettivo di medio termine), nel DEF che ci viene presentato oggi si chiarisce che questa parentesi andrà scemando. Non è detto che nel 2022 la clausola generale di salvaguardia venga prorogata e il Governo non si è voluto impegnare, come invece era stato chiesto in Commissione, a portare

è, infatti, l'obiettivo di questo DEF? È chiarire che il successivo sentiero di avvicinamento all'Obiettivo di medio termine prevede di riportare il rapporto tra debito pubblico e PIL verso i livelli pre-crisi per la fine del decennio. Per fare questo, il sentiero è molto stretto. Cito qualche dato molto sinteticamente per non annoiarvi. Si prevede un decremento dell'indebitamento netto rispetto al 2021, sia in valore assoluto, che rispetto al rapporto con il PIL, di 100

che i 200 miliardi di euro sono di prestito sia nella parte cosiddetta a fondo perduto (perché gravano sul bilancio dell'Unione Europea, che poi dovrà essere ripianato con i bilanci degli Stati membri), sia nella parte

il Patto di stabilità tornerà a essere stringente e quindi dovremo seguire lo stretto sentiero previsto nel DEF. Allo stesso tempo, la BCE smetterà il programma di acquisto dei titoli di Stato italiani e, quindi, di nuovo, per poterci finanziare sul mercato ci sarà sicuramente il problema degli interessi e dello *spread*. Inoltre, se teniamo a mente quanto avvenuto improvvidamente con lo scorso Governo, cioè il rafforzamento Fondo salva-Stati (il famigerato MES, il meccanismo europeo di stabilità), capiamo che il prestatore di ultima istanza sarà quel Fondo che presta - sì - quando gli Stati sono in difficoltà, ma a fronte di cessioni di sovranità.

ossia che uno dei compiti del suo Governo sarebbe stato quello di consentire ulteriori cessioni di sovranità dell'Italia a favore dell'Europa. Non vorrei che la conseguenza di questi tasselli fosse il

A me preme che queste cose restino agli atti. Signor Presidente, colleghi, io vi ho avvertito.

sapendo che fuori il Paese sta aspettando, sta soffrendo e sta resistendo, ci carica di una particolare responsabilità. Oggi a nome di Forza Italia, oltre

Ce la stiamo mettendo tutta, ponendo davanti a tutto la salute, accanto al sostegno per la ripartenza economica, per affiancare l'azione del Governo, portando come Parlamento le istanze dei territori

Quindi vaccini, vaccini e vaccini, aiuti economici diretti e indiretti, grazie alle moratorie e ai crediti di imposta, per vincere la grande sfida di superare l'emergenza e garantire il rilancio. Quando abbiamo deciso di sostenere il governo Draghi, lo abbiamo fatto con totale spirito di servizio, determinati a dare al Paese nel suo momento più difficile la guida più autorevole, più credibile e più corretta, che riuscisse *in primis* a creare stabilità, divergenze da parte di ogni movimento politico, per lavorare insieme al superamento dell'emergenza sanitaria e, di conseguenza, sociale ed economica. Forza Italia porta il proprio contributo quotidianamente, attraverso i propri rappresentanti al Governo e in Parlamento, e lo fa con proposte chiare e concrete che l'Esecutivo dimostra di condividere, inserendole negli indirizzi di Governo. Penso al tema del lavoro flessibile, della reintroduzione di *voucher* di emergenza per il lavoro, ad esempio, proposti dal vice ministro Pichetto Fratin, per far lavorare immediatamente i nostri giovani o chi è rimasto senza lavoro, combattendo nel frattempo il lavoro nero e illegale senza tutele.

(medici, infermieri, professionisti della sanità, farmacisti, Protezione civile, alpini), con un sistema integrato che vede affiancate tutte le realtà ospedaliere in campo. tutela della salute vede Forza Italia affiancare la decisione del Governo di fornire un *green pass* per la libera circolazione, un *pass* della libertà, come a noi piace chiamarlo *(Applausi)*. La proposta è di creare un'applicazione di semplice utilizzo che consenta l'accesso ad eventi sportivi, culturali, fieristici, matrimoni ed eventi in genere. Il Paese ha bisogno di sostegno immediato, ha bisogno di sentirsi al sicuro e per farlo c'è necessità che il Governo, supportato dall'azione del Parlamento, metta in atto ogni possibile intervento per trasformare un indebitamento necessario nella leva per la ripartenza. Insomma, il debito deve trasformarsi in un vero e proprio acceleratore di ripresa e in questo senso infrastrutture e sistema immobiliare possono fare la differenza. Penso, ad esempio, alle *smart city*, le vere città del futuro e penso al centralissimo tema della rigenerazione urbana cui stiamo lavorando e che Forza Italia ritiene fondamentale per il benessere e la crescita armoniosa.

il *bonus* sport e salute, che avrebbe la doppia utilità di sostenere palestre e centri sportivi, consentendo la ripresa fisica e morale dopo la malattia alle persone di ogni età. Per l'emergenza immediata è pronto un altro scostamento di 40 miliardi, quello che siamo oggi votando, per un secondo decreto sostegni per non dimenticare e lasciare indietro nessuno. Penso alla montagna, ad esempio, per la quale stiamo cercando di compensare i mancati introiti di una stagione mai cominciata, nonostante gli investimenti messi in campo. Questo Governo dovrà lavorare per gettare le basi di una visione prospettica complessiva che passi da un sistema rivoluzionario di riforme e di investimenti pubblici: pubblica amministrazione e semplificazione (ce l'abbiamo), giustizia (ce l'abbiamo), fisco (ce l'abbiamo), piano industriale, scuola e formazione, transizione ecologica. transizione ecologica. Quest'ultima dovrà essere e sarà il più grande volano. Per questo, ben venga il nuovo Ministero, che dovrà diventare centrale per lo sviluppo di un mondo nuovo, un mondo che dovrà vedere il pubblico e il privato legati da una grande alleanza con l'ambiente, tutelato proprio grazie al progresso e all'innovazione. Supportare e incentivare le imprese, dalle più grandi a quelle micro, durante il percorso di transizione, sarà l'unico modo per raggiungere gli obiettivi che ci chiede il nostro buon senso, prima che l'Europa, per realizzare quel sistema virtuoso in grado di conciliare lavoro, produzione, coesione sociale e rispetto dell'ambiente. Quale migliore auspicio, proprio oggi che si celebra la Giornata mondiale della Terra? Proprio la crescita economica diventa, quindi, un fattore abilitante della sostenibilità ambientale e sociale. C'è bisogno per questo di certezze e programmazione, perché il mondo *post* pandemia, come hanno ricordato tanti colleghi, non sarà più lo stesso e noi non dovremo più essere gli stessi. Come ha detto giustamente il presidente Draghi nel suo primo intervento alle Camere, sarà necessario sapersi adattare per poter crescere, la politica *in primis*. È fondamentale, come ha ben sottolineato il collega Floris, che è seduto accanto a me, puntare sul capitale umano, sulla formazione, a partire dalla scuola primaria fino all'università,

per i bus turistici fermi, per gli ambulanti, per i commercianti, per i professionisti, per le partite IVA. La pandemia ha cambiato il mondo e l'Italia deve tornare al centro, attraverso la valorizzazione dell'infrastruttura immateriale che possediamo solo noi, il *made in Italy*, quel «fatto in Italia» che deve continuare ad essere la migliore garanzia di qualità e unicità dei nostri territori e dei nostri prodotti. Noi non smetteremo di lavorare affinché tutti possano tornare a lavorare. Forza, Italia!

Presidente, colleghe e colleghi tutti, in questa estesa maggioranza siamo tutti qui per risolvere i problemi dell'Italia e degli italiani. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, ma sensibilità diverse fanno sì che ci sia un dibattito nell'individuare il modo migliore per risolverli. Questo Documento di economia e finanza il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso ha il gravoso compito di tracciare le linee di intervento per il futuro; un futuro che deve essere di ripresa, di ritorno alla normalità, facendo i conti con una crisi sanitaria che ha determinato un disastro economico e sociale. Vorrei, quindi, soffermarmi sul mio modo di vedere alcune soluzioni. Il problema sanitario è stato, a mio avviso, vittima di un errore di base macroscopico; mi riferisco alle cure domiciliari nei primi giorni di malattia. Abbiamo preso atto di questa problematica, abbiamo votato tutti insieme in Senato un ordine del giorno che va nella direzione di favorire le cure domiciliari. Dobbiamo tuttavia crederci tutti insieme. Vi sono medici che ormai, a partire da aprile 2020, hanno curato decine di migliaia di persone. Tra queste persone fortunatamente - loro dicono purtroppo - i morti si contano sulle dita di una mano. Allora, signori, facciamo tesoro di queste esperienze e affianchiamo alla strategia dei vaccini la strategia (l'arma, direi) che già si è dimostrata efficace, quella delle cure precoci nei primi tre giorni di malattia. Soltanto con valide ed efficaci cure possiamo permetterci di affrontare la crisi sanitaria. Tornando al DEF, approveremo in un ulteriore scostamento di 40 miliardi di euro, necessari per aiutare il tessuto economico stremato dalle chiusure; un tessuto economico che, se non riparte, non può essere indennizzato all'infinito. Il miglior sostegno all'economia è la riapertura delle attività economiche, in particolare di quelle ricettive, ma evitando regole poco comprensibili - io le chiamerei regole arbitrarie - per chi vive la vita di tutti i giorni e vede chiaramente le contraddizioni.

legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, occorre una vera semplificazione. Tutti siamo d'accordo sul fatto che la burocrazia sia una piaga di questo Paese, ma paradossalmente continuiamo a complicare la vita dei nostri concittadini con regole sempre più assurde leggi talvolta scritte male che lasciano spazio ad interpretazioni, che bloccano il Paese, come ad esempio sta succedendo per il *superbonus* 110 per cento. Dovremmo mettere mano tutti insieme a queste regole. Per rilanciare questo Paese occorre aiutare le imprese nella loro liquidità e nell'accesso al credito, ma anche migliorando i tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione e garantendo il pagamento dello *stock* di debito residuo. Occorre avviare un percorso di riforma fiscale, ma affiancandola ad un coerente processo di riforma strutturale della riscossione *(Applausi)*, con particolare riferimento alla cancellazione dei crediti fiscali inesigibili e alla possibilità di dilazionare le somme dovute, sospese e non riscosse. Bisogna mettere in atto una vera pacificazione fiscale nel rapporto tra fisco e contribuente e implementare le misure deflattive del contenzioso in essere. Non mi dilungo oltre, signor Presidente, perché noi della Lega ed io come piccola imprenditrice vediamo chiaramente dalla base quali sono le difficoltà del tessuto economico e la

lavoriamo tutti insieme - ripeto - senza preconcetti ideologici nell'interesse di questo nostro bellissimo Paese.

la paura. Il Covid ci ha resi stanchi tutti; la corsa col Covid ci ha reso stanchi tutti. Molti sono oramai rassegnati e pensano che non sia possibile più scollinare, vedere la cima della montagna. Invece, con questo scostamento da 40 miliardi di euro noi stiamo veramente vedendo la cima della montagna e stiamo dicendo che è possibile tornare nuovamente a correre; lo faremo con maggiore agilità, con maggior forza, con maggiore consapevolezza. Questi 40 miliardi saranno destinati a chi in questo periodo ha sofferto di più economicamente: stiamo parlando quindi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi. Questo è importante, ma è soltanto un tassello del *puzzle* che stiamo componendo assieme per dare una visione di uscita definitiva dalla crisi economica causata dal Covid. Questo è uno degli ultimi tasselli,

degli investimenti sul *recovery*, stanno indirizzando la politica economica dell'Europa. È una politica economica che l'Europa deve necessariamente cambiare e non può più essere quella che non è stata in grado di aiutarci di fronte alle gravissime crisi economiche del 2008 e del 2011. Cari colleghi, mi vengono in mente le parole del presidente Draghi, quando ha detto che occorre lasciare un buon pianeta e non solo una buona moneta.

La crisi di Governo che abbiamo vissuto all'inizio del 2021 stava per vanificare completamente il precedente scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro. Adesso sappiamo però dove intervenire. Dobbiamo innanzitutto rendere i ristori più veloci e proporzionati alle vere perdite subite. Per fare questo, già con il decreto sostegni abbiamo abbandonato la logica dei codici Ateco e abbiamo finalmente guardato al fatturato annuale, ma adesso bisogna fare di più. Quindi l'auspicio è che, con le nuove misure, possiamo fare riferimento alle proporzionali riduzioni dei margini delle imprese, e quindi degli utili di impresa, nonché ai costi fissi.

questo è stato per lui un grande problema e adesso è contento che ci sia definitivamente un cambio di logica. Con i 40 miliardi di euro, però, non arriveranno soltanto ristori alle imprese e ai lavoratori,

due misure cardine, volute fortemente dal MoVimento 5 Stelle. La norma Spagna è destinata ai piccoli Comuni, che per troppi anni hanno visto il disinteresse della politica. Tale norma diventa il fulcro del Piano rigenera Italia, voluto dal MoVimento 5 Stelle, che prevede un miliardo di euro ai Comuni, elargiti con stanziamenti da 100.000 a 500.000 euro, a seconda degli abitanti dei Comuni. Con quelle risorse, i nostri sindaci potranno fare interventi di manutenzione e di sostenibilità ambientale; potranno mettere in sicurezza le scuole ed efficientarle energeticamente; potranno terminare una pista ciclabile; ciclabile; manutenere una strada o togliere quelle buche che ogni giorno i genitori e i piccolini affrontano per andare a scuola oppure al lavoro; potranno realizzare un impianto fotovoltaico su una proprietà comunale e - perché no? - diventare capofila per la realizzazione di una comunità energetica in quel Comune, con con tutti i benefici del caso. *(Applausi)*. Abbiamo ricordato prima il superbonus al 110 per cento, una misura che è stata in grado di spalancare due porte, quella del rilancio dell'edilizia, con tanti lavori di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, e quella della cessione, della certificazione e della circolazione del credito di imposta: questa è la vera novità. al 110 per cento ha avuto sicuramente un primo periodo di tentennamento e nessuno lo nega, ma è anche vero che adesso sta volando e lo vedono tutti. Abbiamo superato un miliardo di euro di lavori siamo ben oltre 1,5 miliardi di euro di progetti, che diventeranno quindi crediti aumentati del 10 per cento nei confronti dello Stato. Soprattutto, l'intero Paese è disseminato di cantieri, da Nord a Sud. Pensate che, dall'inizio dell'anno ad oggi, stiamo parlando di un aumento del 500 per E lunedì prossimo è anche la volta di un cantiere di una piccola impresa in provincia di Avellino, che è riuscita finalmente a capire il funzionamento del *superbonus*

Quello del *superbonus*, però, non è un ragionamento fine a se stesso, perché noi vogliamo ampliare il perimetro nel quale riconoscere la circolabilità dei crediti d'imposta. Il MoVimento 5 Stelle

affinché questi diventino una moneta fiscale con cui poter pagare beni, servizi e magari un domani fare la spesa e pagare l'ingegnere, il dottore, l'avvocato.

particolare e caratterizzato da eccezionali fattori di rischio a breve, medio e lungo termine dovuti agli effetti della pandemia. Un rischio a breve termine è soprattutto quello di nuove varianti del virus e quello connesso all'andamento più o meno veloce ed efficace della campagna vaccinale; più a lungo termine il rischio proveniente dalla necessità di ridurre gli squilibri finanziari conseguenti alla pandemia. Il Governo ci consegna un DEF molto ambizioso; dipenderà tutto da come l'Italia sarà in grado di impegnare le risorse europee.

come anche la proposta del collega Misiani di istituire una Commissione bicamerale per accompagnare questo processo per garantire trasparenza e collaborazione tra Governo e Parlamento. Poi sarà fondamentale attuare le riforme della pubblica amministrazione, della giustizia, del fisco, sulla concorrenza e sul lavoro e gli ammortizzatori sociali. Vedo due criticità:

un approccio professionale e veloce da parte della pubblica amministrazione. Il secondo rischio è - a mio avviso - da ravvisare nella necessità di rientrare nel debito, essenziale una volta superata la pandemia. La ripresa si gioca su scelte strategiche di politica industriale, che negli ultimi due decenni l'Italia

economica del 2007 avevamo già - nel primo decennio degli anni Duemila - una stasi della produttività. Sarà infine necessario trattare con la Commissione europea il *temporary framework* sugli aiuti di Stato: bisogna senz'altro estendere la durata degli stessi

con un approccio molto pragmatico e professionale. Per questo sono fiducioso che gli obiettivi posti dal Governo in questo DEF si realizzeranno davvero.

civile del proprio territorio, dove insistono ovviamente differenti problematiche, diverse sensibilità. Certo, importanti provvedimenti - come quelli di oggi sottoposti all'attenzione del Senato - avrebbero meritato un'Aula con tutti presenti ad ascoltare in silenzio; quel silenzio che si addice a un contesto che si propone di trovare delle soluzioni; il silenzio che ha il valore di rispetto per gli italiani che soffrono quotidianamente sulla loro pelle, fisicamente, moralmente, economicamente - tutto su di loro - gli effetti della pandemia. L'avete detto quasi tutti: 40 miliardi di indebitamento sono tanti e, aggiunti a quelli che abbiamo già approvato tra il 2020 e il 2021, arrivano quasi a 200 miliardi. L'avete detto tutti: questi soldi sono indebitamento che ci porteremo avanti negli anni. L'avete detto tutti: bisogna fare le riforme necessarie, per cui cui ho la sensazione - spero positiva - che tutti voi abbiate più o meno contezza che questo provvedimento non è a sé stante

e la normalizzazione della vita quotidiana di ciascuno di noi: è importante tornare alla vita normale, è importante riprendere in mano la nostra vita e avere le quotidianità che la vita ci propone. Ma quando saremo tutti vaccinati, quando la pandemia sarà a riposo, cosa resterà di questa Italia, con tutti i soldi che abbiamo versato, con tutto quello che abbiamo cercato di apportare ma che, se guardate bene e state ben attenti - i vostri territori lo dicono e lo richiamano - pare quasi non esserci stato? stato? Ci sono delle mancanze ancora oggi che vengono reclamate; ci sono settori che non sono stati considerati. Perché perché le normative poste in essere sono state spesso oggetto di una discussione troppo lunga; perché il decreto sostegni - come ho detto prima - stanzia risorse per 32 miliardi, ma vedrà la luce a maggio, dopo 3.000 emendamenti;

finché ci sono debiti c'è vita, perché devi rimboccarti le maniche per onorarli. A questo proposito, permettetemi di aprire una parentesi e di rivolgere un abbraccio al senatore Pittoni, che ha perso il suo papà oggi. Mi ha fatto venire in mente mio padre ed è per questo che l'ho ricordato.

il tavolo, a due mani, a quattro mani, a sei mani, il patto sociale, il patto del diavolo? Facciamo quello che volete, basta che ci spicciamo, perché altrimenti alla fine il problema non sono gli italiani là fuori che hanno bisogno di avere i soldi, ma siamo noi qui dentro.

dobbiamo essere utili e, per poterlo essere, dobbiamo essere efficaci. E forse l'importanza di questo scostamento, che porterà un ulteriore indebitamento, la contezza che andiamo a indebitarci. Ma questi debiti non devono farci paura: dobbiamo essere capaci di affrontarli indipendentemente dagli schieramenti, dalle nicchie, delle spillette, dalle giacche, dai territori, perché l'Italia è una e dobbiamo rimetterla in piedi, perché la malattia se ne andrà e dovremo essere capaci di fare quello che non siamo stati purtroppo capaci di fare negli anni precedenti. Non punto il dito contro nessuno: chi è arrivato prima di me aveva di fronte una situazione economica, sociale e morale totalmente diversa, ma il nostro è un Paese un po' arretrato rispetto a un'Europa che prende i soldi ma ha già le riforme, mentre noi non le abbiamo. Non possiamo continuare a dire che le riforme le faremo. Vi faccio un esempio banale: la legge europea da pagina 50 a pagina 60, al capitolo 8, porta le infrazioni sul codice degli appalti. Non se ne cura. Noi portiamo il PNRR con l'infrazione europea,

Ci mettiamo a fare una riforma della pubblica amministrazione? Giustissima. Una riforma della giustizia? Necessaria. Riforme del lavoro, del fisco? Necessarie. Siamo rimasti indietro. Dobbiamo muoverci, ma stavolta dobbiamo farlo sul serio: non possiamo muoverci solo a parole

e arriveremo a dei livelli per cui non basterà buttare dentro i soldi, perché non solo non li avremo e non saremo capaci di restituirli, ma passeremo alla storia come il problema. Ben vengano 40 miliardi, ne vengano anche 100, onorare i debiti, lavorare a testa china.

243 del 2012, nonché di indicare quale proposta di risoluzione relativa al Documento di economia e finanza intende accettare. Avverto che è in corso la diretta televisiva RAI. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2 (testo 2) relativa al Documento di economia e finanza nel 2021, presentata dai senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone e Unterberger. Il Governo esprime, invece, parere contrario sulla proposta di soluzione n. 1, relativa al Documento di economia e finanza, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori del Gruppo Fratelli d'Italia. Il Governo esprime ancora parere favorevole sulla proposta di soluzione n. 100, presentata alla relazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, dai senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone e Unterberger.

Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per il proficuo dibattito sulla richiesta di scostamento avanzata dal Governo e sul Documento di economia e finanza. Come risulta evidente dalle posizioni emerse e dalla lettura delle diverse proposte di soluzioni, esistono opinioni differenti sulle misure prese dal Governo e su quelle in via di preparazione. L'andamento dell'economia italiana e internazionale, condizionate tutt'ora dall'epidemia da Covid-19 e dalle misure necessarie a contenerne la diffusione, richiede da parte di tutti uno sforzo volto ad assicurare il massimo grado di unità e di impegno per l'uscita dalla crisi. Il Documento di economia e finanza inquadra la richiesta di scostamento in previsione economica e di finanza pubblica ed evidenzia l'impatto che le misure di contenimento dell'epidemia hanno avuto e avranno sull'economia. Come anticipato nei giorni scorsi dal ministro Franco, nel 2020, dopo la forte caduta registrata nel primo trimestre, il PIL in termini reali ha nettamente recuperato nel trimestre estivo, per poi tornare a scendere nell'ultimo trimestre. Il calo di fine 2020 è dipeso da un inasprimento delle misure restrittive per contenere la diffusione dell'epidemia. Secondo le stime ufficiali dell'Istat, il 2020 si è chiuso con una caduta del PIL pari all'8,9 in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali. Le stime tendenziali contenute nel DEF, che tengono conto della creazione del Piano di ripresa e resilienza presentato in gennaio e del decreto-legge sostegni del mese scorso, indicano la crescita annuale del PIL del 2021 pari al 4,1 per cento, a fronte del 6 per cento contenuto nel quadro programmatico della NADEF, pubblicato nel settembre 2020. La revisione al ribasso è dipesa da un quadro epidemiologico più severo delle attese e sostanzialmente in linea con lo scenario più sfavorevole contenuto nella NADEF. Per fronteggiare l'incertezza del quadro epidemiologico ed economico e per minimizzare i rischi connessi con il perdurare di questa fase, il Governo ritiene necessario irrobustire il percorso di crescita per uscire dalla crisi. Dopo aver dato un primo impulso al rilancio dell'economia mediante il decreto-legge varato lo scorso marzo del 2021, denominato sostegni e all'esame del Senato, sulla base del precedente scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, è necessario, infatti, predisporre interventi immediati di sostegno all'economia che, oltre ad accelerare nell'immediato l'avvio della ripresa, assicurano che questa sia duratura, potendo contare nel medio termine su un ingente impiego di risorse assicurato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sottosegretario, la interrompo per ricordare che decorre da questo momento il termine di mezz'ora per presentare eventuali emendamenti a tale proposta. per la maggioranza e il Governo è quella di sostenere i vari settori economici per il tempo necessario e di continuare a compensare le imprese e i lavoratori più danneggiati dalle misure di restrizione sanitarie, al fine di evitare la chiusura definitiva di molte posizioni lavorative e di aziende. Queste ragioni hanno portato il Governo, congiuntamente alla presentazione del DEF, a richiedere al Parlamento di autorizzare un nuovo scostamento dal percorso di rientro verso l'obiettivo di medio termine ai sensi della legge n. 243 del 2012. L'Esecutivo quindi ha ritenuto opportuno annettere al DEF una nuova richiesta di autorizzazione al Parlamento, per ampliare il ricorso all'indebitamento rispetto a quanto previsto finora, scegliendo inoltre di avvalersi della possibilità di inglobare il Programma nazionale di riforma all'interno del Programma nazionale di ripresa e resilienza. Pertanto, il PNR non è stato presentato separatamente, ma è stato sostituito da una trattazione riguardante le riforme all'interno del PNRR, che è in corso di definizione e sarà presentato nei termini previsti alla Commissione europea, previa comunicazione al Parlamento. Il Governo quindi, pur nell'auspicio che il miglioramento delle condizioni epidemiologiche ed economiche rendano quello di oggi l'ultimo intervento di tale portata, intende richiedere per l'anno in corso l'autorizzazione a uno scostamento la cui entità è di 40 miliardi e contestualmente l'autorizzazione a uno scostamento di circa 6 miliardi per gli anni del periodo 2022-2033, finalizzato al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento delle spese per investimenti pubblici. È facilmente intuibile, pertanto, come il Governo intenda utilizzare lo scostamento richiesto per intraprendere un programma di spesa molto ambizioso, che ritiene essenziale per sostenere l'economia in questa fase emergenziale e per assicurare una ripresa stabile e duratura. Le risorse richieste con lo scostamento saranno utilizzate con una duplice finalità. In primo luogo, in continuità con quanto fatto con lo scorso decreto, il Governo ritiene essenziale proseguire e sostenere l'economia con grande determinazione, compensando anzitutto i lavoratori, le famiglie e le imprese più danneggiati dalle misure restrittive che si sono rese necessarie. In secondo luogo, parte delle risorse dello scostamento sarà utilizzata per accompagnare e rafforzare la risposta dell'economia nelle prime fasi della ripresa dei prossimi trimestri, essendo fondamentale tornare presto a crescere a ritmi sostenuti e in modo duraturo. Si stanno in particolare definendo i dettagli degli interventi che saranno contenuti nel prossimo decreto-legge, anche sulla base dei contributi emersi dall'attento esame degli ordini del giorno che sono stati approvati dalla Camera e dal Senato sui precedenti provvedimenti economici varati dal Governo.

Il decreto di prossima approvazione conterrà nuovi contributi a fondo perduto, compresa una compensazione per i costi fissi, e destinerà risorse al rafforzamento della resilienza delle aziende più colpite dalle dalle chiusure, alla disponibilità di credito e alla patrimonializzazione delle imprese. Sono allo studio interventi a favore dei giovani, per l'acquisto della prima casa, e delle famiglie più in difficoltà, anche attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse per gli enti territoriali. La strategia che il Governo intende mettere in atto con questo nuovo scostamento non si esaurisce, tuttavia, nell'anno in corso. Infatti la seconda direttrice della strategia uscita dalla crisi ha un orizzonte pluriennale e si baserà su un forte impulso sugli investimenti. Come ha anticipato nella scorsa audizione anche il ministro Franco, a breve finanzieremo il PNRR, che, oltre a delineare una serie di riforme strutturali, consentirà di programmare e finalizzare investimenti per oltre 190 miliardi. Ciononostante, il Governo ritiene opportuno rafforzare il programma di investimenti del PNRR con lo stanziamento di ulteriori risorse nazionali, destinate a una serie di progetti aggiuntivi considerati prioritari, che non hanno trovato capienza nell'ambito dei fondi europei. In particolare, le risorse del Piano complementare sono destinate a progetti che, seppur ritenuti prioritari, non è stato possibile includere nel programma europeo e che saranno, comunque, corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi (*target e milestone*), monitorati e controllati dalle autorità nazionali con le stesse modalità previste per il PNRR. L'approccio basato su *target* e *milestone* secondo una *timeline* predefinita, infatti, permette di monitorare tutte le fasi di realizzazione di un intervento pubblico e di identificare tempestivamente le cause che possono determinare il blocco degli investimenti, oltre a garantire la massima trasparenza sull'impiego delle risorse. Parallelamente alle misure di sostegno dell'economia, è nondimeno necessaria una prudente gestione della finanza pubblica per intraprendere un percorso di progressiva riduzione del debito; percorso indispensabile anche alla luce del contesto europeo in cui si troverà ad operare la politica di bilancio nei prossimi anni. anni. Le condizioni finanziarie per l'emissione dei nostri titoli di debito sono distese, anche grazie ai rilevanti programmi di acquisto da parte della BCE. Tali misure continueranno ad essere operative

ci aspettiamo che anche il prossimo anno rimangano tali. Sebbene riteniamo convintamente che tali regole dovranno essere oggetto di un ripensamento, certamente torneranno in vigore nei prossimi anni finanze pubbliche in ordine in tutti i Paesi dell'Unione europea. Sarà, quindi, necessario avviare una riflessione per guidare il futuro rientro della situazione attuale di eccessivo indebitamento; rientro che potrà avvenire solo mettendo in atto senza indugi il piano di investimenti richiamato e rivolgendo particolare attenzione alla spesa corrente, che dovrà fornire un contributo importante al ripensamento dei conti pubblici. Rispetto alle considerazioni dei colleghi intervenuti nel corso del dibattito, che ringrazio per il contributo recato alla discussione, intendo effettuare alcune precisazioni, chiedendo scusa se non riuscirò a farlo puntualmente per tutti. tengo a rimarcare in questa sede, che rappresenta la massima espressione della democrazia, che il Governo ha ben chiara la centralità del Parlamento e della imprescindibilità di una sua continua interlocuzione nelle scelte. In merito all'osservazione relativa all'assenza di alcuni documenti di corredo del DEF, mi preme indicare che, in data 20 aprile scorso, sono stati inviati il rapporto sulla stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, previsto dall'articolo 3 della legge n. 196 del 2009, e il documento delle spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome, entrambi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, sempre con riferimento a quanto emerso dagli interventi precedenti, ricordo che in ambito europeo è in corso un dibattito sulle regole di bilancio e che c'è piena consapevolezza di tutti i Paesi dell'euro e dell'Unione europea in generale che eventuali azioni individuali dei singoli Paesi sarebbero prive di efficacia e probabilmente controproducenti. Circa le osservazioni in merito alla necessità di una visione prospettica per sostenere il periodo di crisi di oggi, pieno di rischi e volto alla crescita per domani, si ribadisce che l'intento del Governo è quello di affrontare l'emergenza guardando al futuro e alla strategia del Paese 2030-2050, come affermato anche dal presidente Draghi nelle sue ultime comunicazioni dello scorso febbraio. Ribadisco altresì che il Governo ha sempre sostenuto che gli interventi per la ripresa e la resilienza possano attingere a una strategia integrata fatta non solo di PNRR, ma anche di programmazione europea, il cui utilizzo verrà migliorato, e da ulteriori risorse di bilancio. Con riguardo all'esigenza di fornire certezza in questa fase di particolare difficoltà, anche attraverso l'allungamento del rimborso delle garanzie a trenta anni, tengo a precisare che il Governo sta agendo in questa direzione. Infatti, sta valutando possibili misure per consentire l'allungamento dei prestiti e l'estensione temporale delle garanzie pubbliche. Queste misure devono essere compatibili col *temporary framework.* Dal dibattito è emersa anche l'esigenza di avviare una riforma fiscale più equa e organica. Anche in questo caso, voglio rassicurare che la riforma del fisco e in particolare dell'Irpef è una priorità del Governo, che a tal fine si avvarrà dell'ingente e prezioso lavoro svolto dalle Commissioni di Camera e Senato in materia. Quanto, infine, agli interventi dei colleghi in merito alle tematiche di carattere fiscale, mi preme evidenziare che la pressione fiscale in rapporto al Pil si è attestata nel 2020 al 43,1 in aumento di sette decimi di punto rispetto al 2019. Questo andamento dell'indicatore di pressione fiscale nel corso del 2020 dipende non da modifiche normative (ad esempio, aumenti di aliquote) che hanno comportato aumento del prelievo tributario e contributivo, ma da fattori di tipo tecnico. Nel 2020 le entrate complessive nella pubblica amministrazione includono una stima di alcuni versamenti tributari e contributivi del 2020, che il Governo ha sospeso e differito agli anni successivi, con le disposizioni introdotte per sostenere i contribuenti e le attività economiche più severamente colpiti dalle misure di restrizione a seguito dell'emergenza economica sanitaria. La riclassificazione di queste entrate dal 2020 è stata effettuata per assicurare una corretta registrazione dei flussi in base al principio della competenza economica, in coerenza con quanto previsto dal sistema europeo dei conti. Si tratta di circa 8,1 miliardi di entrate tributarie e di 1,5 miliardi di contributi sociali. Per lo stesso motivo le entrate 2020 includono anche 700 milioni a titolo di imposta sui servizi digitali (imposta la cui scadenza è prevista per il prossimo 16 maggio). Questi flussi hanno contribuito a innalzare il livello delle entrate nel 2020 e si sono riflesse nell'aumento della pressione fiscale calcolato nel 2020 rispetto all'anno precedente. Ricalcolando la pressione fiscale al netto delle entrate tributarie e dei contributi riassegnati al 2020 e al netto del trattamento integrativo,

- il più alto grado di unità, collaborazione e dialogo tra tutte le forze del Paese. Si tratta di una sfida difficile, ma noi pensiamo che questo Paese sia in grado di affrontarla e superarla. Chiediamo per questo un largo sostegno e un voto comune del Parlamento sulla richiesta di scostamento e anche sul sottostante Documento di economia e finanza, che presenta le previsioni su cui si fonda la richiesta di scostamento. L'auspicio del Governo è che il nuovo scostamento di bilancio che chiediamo al Parlamento di approvare raccolga il sostegno di tutte le forze politiche e sia l'ultimo prima di una generale ripresa della nostra economia. Grazie anche alla piena attuazione del piano di vaccinazione, il Paese potrà avviarsi lungo un sentiero di ripresa che consenta di superare uno dei periodi più difficili della storia repubblicana.

di sciogliere le criticità strutturali che hanno caratterizzato l'economia italiana prima della pandemia. Per raggiungere questi obiettivi occorre grande coraggio nelle riforme indicate nel percorso: velocizzare la macchina giudiziaria, ridurre il costo del lavoro e iniettare competenze nella pubblica amministrazione attraverso la formazione del personale e un piano di assunzioni che guardi soprattutto agli enti locali e alle strutture periferiche. Ma ciò non basta, serve anche un ripensamento della politica industriale per aumentare la competitività dell'Italia. Nel DEF si collega poi la sostenibilità del debito a questa importante capacità di crescita: una scommessa doverosa, purché non si trasformi in un azzardo. Per questo motivo, sarebbe opportuno immaginare con l'Europa anche un piano alternativo di rientro dal debito (discorso, questo, strettamente intrecciato con quello sul Patto di stabilità). È impensabile che, dopo tutto quello che è successo, prima o poi si torni alle regole esistenti,

175 miliardi di euro di maggior indebitamento dall'inizio della pandemia, cui andranno aggiunti 120 miliardi non a fondo perduto del *recovery*. Per questo, dobbiamo rendere sempre più efficienti i criteri di distribuzione di queste risorse. Il cosiddetto decreto sostegni ha avuto il merito di aver sostituito i codici Ateco con le perdite di fatturato tra il 2019 e il 2020. Credo però che questo lasso temporale non sia adeguato. Capisco la motivazione di chi dice che, lasciando tutto inalterato, gli aiuti andranno in automatico e senza intoppi burocratici, ci vogliono elementi perequativi. Ritengo che la soluzione ottimale sia far decidere alle aziende il periodo di riferimento, scegliendo tra l'anno solare 2019 e l'anno solare 2020 o, in alternativa, tra i dodici mesi che vanno da marzo 2019 a marzo 2020, a quelli che vanno da marzo 2020 a marzo 2021. In questo modo non si renderebbe giustizia a coloro che nel 2021 non hanno lavorato neppure un giorno. E ciò vale soprattutto per l'economia di montagna, che è stata la più colpita dalle restrizioni degli ultimi mesi. Sarebbe però un errore pensare che queste risorse, per quanto importanti, possano risolvere il nodo liquidità, che è la vera questione per la sopravvivenza delle imprese. Secondo il *report* Svimez-MCC delle oltre 200.000 imprese che hanno contratto prestiti garantiti nel periodo Covid, 67.000 con redditività buona e indebitamento sostenibile sarebbero scese di categoria senza quei prestiti e almeno 56.000 sarebbero finite nella classe peggiore, ossia con redditività bassa, forte debito e poca liquidità. Per questo occorre prolungare e potenziare le misure a sostegno della liquidità, non solo con i contributi a fondo perduto, ma anche con l'allungamento degli ammortamenti e crediti d'imposta. modo, va rafforzata nel medio termine la loro patrimonializzazione e la diversificazione delle fonti finanziarie. Intanto, già nella conversione del primo decreto sostegni, si deve lavorare sul filone dei costi fissi e sulle questioni legate ad affitti (Tari, IMU, TOSAP, canone Rai). Tra gli emendamenti presentati in Senato ce ne sono diversi che vanno in questa direzione. Mi colpisce, invece, che nel decreto sostegni non sia stato affrontato a sufficienza il tema dei lavoratori stagionali. Nella sola Provincia autonoma di Bolzano nel 2020 gli stagionali sono stati occupati per appena tre mesi e mezzo, contro gli otto mesi degli anni precedenti. Si calcola che le persone che da gennaio non hanno più la copertura della Nuova prestazione Per questo mi auguro che questo scostamento di bilancio serva anche per rinnovare e prorogare questo ammortizzatore sociale. Il migliore aiuto però, signor Presidente, sono le aperture in sicurezza. I cittadini hanno compreso il primo *lockdown*, perché in quel momento era giusto che si chiudesse: non avevamo mascherine, non avevamo neppure disinfettanti, non avevamo i posti in terapia intensiva e non sapevamo nulla delle modalità di trasmissione del virus. Anche in autunno lo abbiamo compreso: non c'era una diffusione così capillare dei test rapidi e, soprattutto, mancavano ancora i vaccini. Adesso però i tamponi sono accessibili a tutti e sui vaccini la macchina organizzativa sta funzionando al netto dei ritardi nelle consegne. bene, quindi, che almeno sulle attività all'aperto ci sia un allentamento. Forse si poteva farlo anche prima, visto che la scienza ci dice che su 1.000 contagi solo uno avviene all'aperto. Anche sui luoghi chiusi, però, si deve fare qualcosa, allentando ulteriormente la morsa sulle limitazioni ai diritti individuali costituzionalmente garantiti. Il Sudtirolo ha implementato un progetto che in qualche modo ricalca e anticipa quello del *pass* vaccinale. L'obiettivo è creare delle Covid *safe area* per cinema, teatri, palestre, ristoranti e altri luoghi chiusi, il che vuol dire consentire l'accesso a persone che sono state già vaccinate o che si sono sottoposte a tampone veloce nelle settantadue ore precedenti. L'idea è che l'azienda sanitaria rilasci alle persone vaccinate un QR *code* su carta o via *e-mail* o SMS. Le persone che invece hanno fatto un tampone possono inserire i risultati del test negativo nel *database* dei test Covid Covid dell'azienda sanitaria. Possono essere presi in considerazione anche i test fai da te, purché eseguiti in presenza di persone a ciò autorizzate. A quel punto le persone negative presenteranno il loro QR all'entrata della *Covid* *safe area*, dove uno *scanner* simile a quello che troviamo negli aeroporti indicherà una luce verde per consentirne l'accesso o uno rosso, se i requisiti non sono invece soddisfacenti, ad esempio se sono trascorse più di settantadue ore dall'effettuazione del tampone. Questo sistema è un fortissimo incentivo a fare i test diventa così uno strumento di monitoraggio costante e capillare, perché intercetta anche tutte quelle persone che non hanno mai fatto un test diagnostico per la paura di essere messe semmai in quarantena; adesso che gli si offre libertà, sono intenzionate a fare i test, per cui i focolai sono molto più facili da individuare subito. Noi potremmo fare da laboratorio, per cui spero davvero che il Governo nazionale non voglia opporsi a questa opportunità. Francamente cittadini e operatori economici, dopo tutto quello che hanno patito in questi mesi, lo vivrebbero come un ingiustificato atto vessatorio. Si dia allora la possibilità di seguire questa strada: a guadagnarci possono essere tutti. È

Signor Presidente, noi siamo molto convinti dalla svolta impressa da questo Governo. erano tre timidezze che temevamo rispetto all'azione del passato Governo, che rischiavano di trascinare il Paese nell'oblio, e devo dire che le abbiamo superate o le stiamo superando. Naturalmente bisogna insistere. Le timidezze erano le seguenti: quella legata alla ripartenza, quella legata alla mancata scommessa sulla crescita e quella sul piano vaccini. vaccini. Le abbiamo superate ragionando e senza spacconeria e credo sia merito di questo Governo, in particolar modo del Presidente del Consiglio. leggere quello scienziato di Montanari definire Draghi come Bolsonaro fa rabbrividire, perché è una sciocchezza enorme. Finalmente invece ci si sta avviando, irreversibilmente, verso la normalità; d'ora in avanti sarà un crescendo e non si tornerà più indietro. avremo naturalmente a cuore la gestione dell'emergenza sanitaria e non dimenticheremo che la priorità sarà ancora investire sulla sanità. Il Governo ha preso una decisione politica, ascoltando naturalmente gli scienziati, ma senza farsi sostituire e deresponsabilizzare: si riduce sensibilmente la fase della compressione dei diritti (era ora) e si rilanciano le attività sociali, culturali ed economiche. Senza questa azione immediata avremmo potuto fare tutti gli scostamenti possibili, tutte le misure economiche possibili, non saremmo riusciti a rilanciare la nostra economia. Ripartire e vaccinare a ritmi forsennati sono due azioni indispensabili, da affiancare a provvedimenti economici e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui discuteremo la prossima settimana con il Presidente del Consiglio. Abbiamo il dovere di pensare anche ai non garantiti, a chi non riceve comunque a casa uno stipendio o una pensione. Non Non è democratico un Paese in cui qualcuno può decidere di non andare a lavoro perché non si sente al sicuro e un altro, invece, non può permetterselo perché altrimenti non guadagna e muore di fame. Per questo il prossimo decreto sostegni, Presidente, non potrà essere la fotocopia di quello che stiamo esaminando già oggi in Senato. Serviranno misure forti di aiuto alla liquidità e alla capitalizzazione delle imprese; servirà, ad esempio, un'ulteriore proroga della moratoria dei mutui. È impensabile che si possa chiedere di onorare gli impegni con puntualità in una situazione economica ancora ferma. ferma. Bisognerà, poi, insistere con una serie di misure che accompagnino la ripartenza: l'esenzione da Tari, COSAP, TOSAP. Scommettere sulla crescita: dimostra di voler fare così questo Governo, con questo DEF e con il nuovo scostamento. È stata la timidezza del passato Governo su questo tema a determinare un punto di rottura qualche tempo fa e la fine di quell'esperienza. Il punto di dissenso era sul fatto che immaginavamo che quel PNRR

con più investimenti pubblici. E chi dice che nulla è cambiato mente sapendo di mentire. Eravamo noi a invocare quanto ora si sta facendo: uscire dal debito con la crescita. È finito il tempo dei sussidi, Presidente, a volte inevitabili, ma che non possono rappresentare la normalità di un Paese. Il debito del Paese non è irrilevante; oggi il debito è buono - l'ho sentito dire da tanti interventi - e va finalizzato alla crescita, ma dovremo essere bravi ad abbandonare questa percezione quando sarà necessario. Abbiamo a disposizione tre *recovery* da sfruttare al meglio: quello europeo da 210 miliardi e due domestici: i 181 miliardi risparmiati dagli italiani durante la pandemia, che soltanto creando un clima di fiducia riusciremo a mobilitare, e più di 120 miliardi di euro per la realizzazione delle opere pubbliche bloccati dalla burocrazia. Naturalmente, per investire queste risorse economiche sarà necessario intervenire con un'azione riformatrice forte che rada al suolo la burocrazia e migliori l'efficienza della pubblica amministrazione. Signor Presidente, la pandemia ha toccato tutti, ma non ha colpito tutti allo stesso modo. L'Ipsos ci ha segnalato un dato allarmante: il ceto medio, un tempo corpo centrale del nostro Paese, si sta erodendo; cento degli italiani ha difficoltà per gli acquisti alimentari; il 16 per cento ha difficoltà a pagare le bollette; il 37 per cento ha difficoltà a far fronte ad una spesa imprevista; 1 milione di posti di lavoro sono andati perduti, soprattutto tra le donne e i giovani; è aumentata sensibilmente la quantità di giovani scoraggiati. sono ottimista sulla ripresa: c'è e ci sarà, ma non sarà scontato farne parte. Se non gestita bene, questa fase rischia di aggravare le diseguaglianze e di crearne di nuove. Dobbiamo evitare che non tutti i gruppi sociali, i lavoratori, le imprese, i territori a partire dal Sud e dalle aree interne siano attrezzati a prendere questo vento. L'aumento del PIL è una condizione necessaria, ma non sufficiente; dovremo lavorare anche sugli aspetti relativi all'organizzazione sociale, famiglia e scuola *in primis*, per consentire ai penalizzati di poter partecipare a questo rilancio.

Signor Presidente, il Documento di economia e finanza costituisce sempre il principale strumento di programmazione della finanza pubblica, ma il DEF 2020 rappresenta - possiamo dirlo - un *unicum*, perché delinea un quadro macroeconomico condizionato dagli effetti dell'emergenza pandemica e perché considera due ulteriori provvedimenti, ovvero il decreto-legge con misure di sostegno e di rilancio, legato alla proposta di scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro, e l'adozione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alle risorse del DEF si aggiungono quelle previste dal programma Next generation EU e quelle del cosiddetto "fondone" di investimenti complementari per finanziare gli interventi programmati nella versione finale del PNRR, ma non coperti né dai prestiti né dalle sovvenzioni del *recovery*. Il DEF contempla anche alcuni scenari di rischio, come una limitata efficacia dei vaccini rispetto alle varianti del Covid, con le ipotesi di conseguenti ulteriori misure di limitazione delle attività economiche e sociali, nonché un potenziale di rischio - aggiungiamo noi - che potrebbe essere quello di mancare l'obiettivo di vaccinare l'80 per cento della popolazione entro l'autunno.

ottimistico, per non dire infondato, se consideriamo, ad esempio, la contrazione del PIL registrata nel primo trimestre del 2021 con un meno 1,2 per cento. Inoltre, le proiezioni del DEF sulla ricaduta occupazionale risultano così modeste da essere preoccupanti. Questo ci ci ricorda solo una cosa: la ripresa si costruisce con le riaperture. E ci chiediamo, dunque, come pensa il Governo di conciliare la previsione della progressiva riduzione del rapporto debito-PIL e l'incremento del PIL con quelle mazzate economiche - scusate l'espressione - stabilite ieri, con il mantenimento alle ore 22 del coprifuoco e quelle riaperture finte, solo per bar e ristoranti che hanno spazi esterni. In tal modo si condannano all'agonia economica, almeno fino al 1o giugno, tutte quelle attività del settore che non hanno spazi esterni e si rischia di

di tassi di crescita sostenuti e di una programmazione di interventi duraturi, esattamente quello che non c'è nel DEF. Scusate, ma tutto il resto non è un documento di programmazione ma, oserei dire, un azzardo da tavolo da gioco. Nel 2020, infatti, il PIL ha registrato una caduta dell'8,9 per cento. Si tratta di una contrazione dell'attività economica senza precedenti storici in tempi di pace e questo amplifica la drammatica contraddizione, rilevata dal DEF, della crescita della pressione fiscale

quindi non capisco come le vostre previsioni di una diminuzione della pressione fiscale si avvereranno. Comunque: auguri! La caduta dell'economia nel 2020 è dovuta alle misure restrittive, alla contrazione dei consumi privati, alla perdita di quasi un milione di posti di lavoro e all'impennata delle nuove povertà, che hanno colpito le famiglie italiane: un *record* negativo assoluto. È alle famiglie italiane che si dovrebbe pensare e invece sono escluse dal PNRR, mentre notiamo - lo diciamo con polemica - che il Governo sostiene, all'interno del DEF, che per aumentare il PIL abbiamo bisogno di un maggior flusso di immigrati, con un un terzo. Fratelli d'Italia pensa invece che il Governo dei migliori dovrebbe mettere al primo posto gli italiani, favorire la natalità e la demografia e dare più risorse alle famiglie, alle imprese, agli artigiani e ai lavoratori.

nella migliore delle ipotesi una dichiarazione di buone intenzioni. Vogliamo dire che è una scommessa sul debito buono? Il tempo delle scommesse però è finito! Quello che serve è una crescita solida, una visione organica e delle riforme reali, che nel DEF non ci sono, mentre di quelle accennate, come la riforma fiscale e della pubblica amministrazione, non conosciamo né linee, né contenuti, come non si conoscono - ed è grave - i contenuti del PNRR, che il Gruppo Fratelli d'Italia aveva chiesto di allegare al DEF, come avevamo chiesto che ci fosse del tempo per discuterne in Parlamento. Questo tempo, però, non ci sarà: il piano andrà direttamente a Bruxelles e nessuno conosce i dettagli, esattamente come, in questo DEF,

Ricordiamo che è stato grazie al voto favorevole delle opposizioni che sono stati approvati i precedenti scostamenti. Una cosa deve essere chiara: noi non votiamo per il Governo ma per l'Italia e non dovete chiedere un voto al buio senza spiegare come spendere questo ulteriore indebitamento! Né possiamo accettare di scaricare ulteriori debiti su figli e nipoti, continuando a spendere male o sperperando in *bonus,* mancette e marchette che non favoriscono la ripresa della Nazione, come è accaduto con il Governo precedente che ha varato *bonus* improduttivi e microinterventi tra i più disparati per un totale di 170 miliardi, frutto di scostamenti spesi in mille rivoli per cui oggi nessuna categoria può dire di essere stata davvero ristorata rispetto ai danni subiti. Avviandomi alla conclusione, la somma degli scostamenti fatti fin qui non è solo un'estensione del debito pubblico per rispondere alla crisi pandemica - lo sappiamo - ma, con la gestione sbagliata della spesa, rappresenta un eccesso di debito pubblico, perché anche nel fare debito serve serietà, distinguendo quello necessario da quello voluttuario. Per capirci - non vi arrabbiate - monopattini e biciclette sono voluttuari. Per questo Fratelli d'Italia continua a chiedere che tutte che tutte le risorse, ogni centesimo del prossimo scostamento, vadano unicamente al nostro tessuto produttivo, che non si buttino via i soldi in riffe di Stato come il *cashback*! Piuttosto chiediamo indennizzi

(la guerra è al Covid ma siamo in tempo di pace), però il pensiero va alla ricostruzione post-bellica, quando il Governo decise con il prestito chi avrebbe ricostruito l'Italia. Si disse che sarebbero stati gli operai.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il Documento di economia e finanza rappresenta senza dubbio l'atto più significativo, più importante, per verificare la sostenibilità della finanza pubblica. Rappresenta il cuore della programmazione economica e sociale del nostro Paese, non è un atto burocratico o tecnico, contiene scelte politiche fondamentali per il futuro dell'Italia. I dati tendenziali e programmatici misurano con chiarezza gli effetti sulla crescita e sull'occupazione, nonché le azioni necessarie sul versante economico per rimettere al centro un nuovo sviluppo fondato sulla conversione ambientale, sociale e finanziaria del nostro Paese.

ed altri) hanno ricordato con grande chiarezza e con forza l'esigenza di un nuovo progetto industriale, un'esigenza indispensabile per individuare i nuovi assi portanti delle nuove filiere produttive, perché solo individuandoli potremo connettere formazione, ricerca e università ad un nuovo modello di sviluppo economico e sociale. Per noi, colleghi, è insostenibile e sbagliato per l'Italia contrapporre le azioni ed i progetti per garantire la coesione sociale con le misure espansive per favorire nuova crescita economica: sono due facce della stessa medaglia. Colleghi, nel conflitto sociale, con tassi di povertà crescenti, nel dilagare della solitudine e nell'allargare la forbice delle disuguaglianze, non si realizza un terreno fertile per nuove opportunità e per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia. La pandemia ha prodotto la recessione più ampia dal Dopoguerra a oggi (8,9 punti percentuali di PIL in meno) e in Italia, già prima della pandemia, problemi strutturali irrisolti rallentavano la crescita e ampliavano le disuguaglianze. Per il Partito Democratico garantire al Paese una speranza, non un'illusione, e una nuova programmazione sociale ed economica costituisce la radice del nostro impegno, nel Governo Draghi e nel Paese. Per noi è da irresponsabili usare e piegare le tante sofferenze presenti nel Paese per una gestione del consenso. Per noi è indispensabile trasformare le sofferenze, la rabbia, la solitudine in nuove opportunità per uscire dalla pandemia. Ai giovani, alle donne, al Mezzogiorno dobbiamo orientare la massima attenzione e realizzare i progetti strutturali più efficaci per ritornare a crescere. Diciamo no a un assistenzialismo di facciata, che per gestire il consenso chiude le sofferenze e la solitudine in un recinto. Queste sono per noi le basi di una democrazia; queste sono per noi le radici anche del nuovo europeismo, che riveda il Patto di stabilità e favorisca gli investimenti sostenibili e compatibili con le diverse transizioni ambientali, ecologiche, digitali e sociali, necessarie per garantire un futuro a questo Paese. La credibilità del presidente Draghi, del Governo, delle istituzioni italiane è fondamentale e decisiva anche per rendere sostenibile il nostro debito. Non si deve scalfire con l'inutile propaganda da coprifuoco; in gioco c'è il destino dell'Italia. Senatore Salvini, il Partito Democratico non prende lezioni da nessuno. *(Applausi).* Soprattutto non accetta la critica di ipocrisia. Non confonda l'ipocrisia con la responsabilità. Vogliamo riaprire le attività economiche e sociali, lo vogliamo tutti; lo vogliamo fare in sicurezza per non sprofondare in una nuova ondata pandemica, e soprattutto lo vogliamo fare scegliendo la responsabilità. Anche la Lega sa scegliere tra responsabilità, Governo e irresponsabilità e opposizione. *(Applausi)*. Sono decisioni che vi attendono e ci attendono insieme al varco degli italiani. Colleghi, non se ne esce. Dovremo saper scegliere insieme il nuovo volto dell'Europa e dovremo saper scegliere di staccarci insieme dall'idea sbagliata di un'Europa che nuovamente ricentralizza confini e Stati. Non abbiamo nulla a che vedere con l'Europa di Orban e dei suoi soci e seguaci; quell'Europa non garantisce futuro. Per queste ragioni, insieme a voi, dobbiamo realizzare questa nuova sfida e sostenere il nuovo volto dell'Europa per garantire un futuro ai nostri giovani. Di fronte a noi c'è una sfida molto difficile; le sofferenze possono produrre disordine. Di fronte a noi ci sono anche, però, nuove opportunità per progettare il futuro dell'Italia. Possiamo dire che il DEF ha al suo interno due grandi opportunità, 40 miliardi di euro per aiutare i settori più colpiti dalla crisi pandemica, attraverso le misure per favorire la liquidità delle imprese. I dati industriali ci confermano con forza e nettezza nel primo trimestre che c'è una ripresa possibile per l'industria, l'edilizia, la manifattura, il *packaging*, l'industria che esporta; ma c'è una crisi violenta sui servizi, sul turismo, sul commercio. A loro dobbiamo dedicare l'impegno più importante *(Applausi)* per garantire un abbattimento dei consumi, dei costi fissi, ripristinare misure che avevamo anche introdotto, a cominciare dal credito di imposta sulle locazioni per gli immobili commerciali e turistici. ai banchi del Governo - sul turismo serve un investimento strategico, su una filiera fondamentale per recuperare Prodotto interno lordo. L'Italia è una piattaforma naturale. Dobbiamo evitare di disperdere la nostra rete alberghiera, il nostro patrimonio genetico dell'accoglienza, la nostra capacità di crescere nelle dorsali più importanti del turismo italiano. Lì non bastano gli interventi di sostegno; servono sostegni precisi agli investimenti e lo Stato deve farsene carico perché, dietro l'angolo, con la ripresa del turismo c'è una crescita possibile di PIL, di lavoro, di occupazione, di benessere. È per che diciamo con forza che la sfida più importante è rappresentata dalle riforme. I 230 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza richiedono una stagione riformista, richiedono la capacità di leggere questi straordinari cambiamenti: la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, della concorrenza, del fisco sono iniziative fondamentali per dare velocità, coerenza, motore alla realizzazione di progetti così importanti, perché solo attraverso un rilancio degli investimenti potremo garantire nuova crescita economica.

fino al 2024 non recupereremo i tassi di occupazione antecedenti alla crisi pandemica; quindi, decidiamo insieme: serve una Commissione per valutare attentamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza. il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questo Piano dobbiamo individuare dei coefficienti e delle priorità che, secondo noi, devono riguardare l'occupazione e il contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile. Pensiamo ad un Paese nel quale torni ad essere normale l'ambizione di far nascere un figlio. Colleghi, pensiamo ad un Paese nel quale lo Stato riduca le distanze con i giovani e offra loro nuove opportunità per la formazione, il lavoro, la ricerca. Pensiamo ad un Paese che investa nella formazione, che contrasti la povertà non solo con il reddito di cittadinanza, ma anche con un reddito di formazione, centrale nelle riforme degli ammortizzatori sociali. Pretendiamo un Paese nel quale intraprendere una professione, progettare un'impresa torni ad essere normale e semplice e la pubblica amministrazione, anziché ostacolare, favorisca i progetti per una nuova economia sociale. Vogliamo progettare un Paese che sappia, con lo sviluppo della scienza, della formazione, della ricerca, produrre i vaccini necessari per proteggere tutti noi da eventuali varianti pandemiche e da nuove pandemie. Riteniamo che occorra restituire centralità alla medicina di base, per troppo tempo messa ai margini dalle riforme sanitarie. Pensiamo alle cure domiciliari, al nuovo volto del sistema sociale e sanitario nel territorio, in grado di formare e favorire sintesi anche tra le giovani generazioni. Si vince insieme con le riforme e il riformismo può incontrare nuovamente il suo popolo. Facciamo qui uno sforzo insieme per essere all'altezza. Per queste ragioni, il Gruppo Partito Democratico dichiara il voto favorevole sulla risoluzione per lo scostamento e esprime un apprezzamento sul Documento di economia e finanza.

parto da un'inevitabile considerazione politica: ieri mattina il Capogruppo della Lega ha voluto richiamare tutti noi alla responsabilità, peraltro con un richiamo improprio, perché fuori dal perimetro delle scelte e dei provvedimenti del Governo, in quanto riferito al disegno di legge Zan. Ieri pomeriggio la Lega si è astenuta su un decreto del Governo su un punto fondamentale della vita di questo Esecutivo: il governo della pandemia, mettendo in difficoltà tutto il Governo e gli stessi Ministri della Lega. La contraddizione credo sia palese e clamorosa, ma c'è un punto politico: è ovvio affermare che nessuno può immaginare di stare in una maggioranza e, a seconda delle proprie convenienze, dei sondaggi, della irrefrenabile tentazione di cavalcare qualunque protesta, fare quello che vuole, lanciare *ultimatum*, mettere in difficoltà il Governo. Noi lo sappiamo che questo è il Governo Draghi e non il Governo Conte. Forse è Salvini che non sa che questo non è il Governo Salvini. Questo schema di gioco è infantile, irresponsabile e oggettivamente insostenibile. Decidete che parte volete fare perché questa non è una commedia. Non possiamo giocare con i sentimenti, la rabbia e le difficoltà di un Paese. Qui si gioca la responsabilità, che involontariamente ieri il Capogruppo della Lega ha richiamato e che oggi suona come un richiamo allo stesso partito della Lega. Noi votiamo convintamente il DEF e lo scostamento. Il DEF è un'impresa coraggiosa e una scommessa che si fonda su due punti fondamentali: la sconfitta

la possibilità di dare un futuro al Paese. Per la riforma della pubblica amministrazione la parola chiave è competenze. Bisogna dare ai Comuni, alle Province e alle Regioni le competenze necessarie per realizzare quegli investimenti, trovando le forme più celeri e trasparenti. È una scelta inevitabile. Serve, inoltre, perché il caos in cui è l'assetto fiscale del Paese è evidente a tutti e dobbiamo diminuire il peso sul lavoro e sulle imprese

una nuova politica industriale che abbia al centro, come architrave, la transizione ecologica e, sulla base di questo, superare gli incentivi a pioggia per le imprese. trovare la chiave per produrre una crescita non solo sostenibile, ma che sia in grado di dare nuovo lavoro. I dati del DEF ci dicono che il tema dell'occupazione è il più critico e serio. Proporremo che il Governo si metta alla prova per produrre un piano straordinario per il buon lavoro, la buona occupazione e contro la precarietà. Al centro ci devono essere il Sud, le donne e i giovani. È su questo che possiamo dare fiducia al Paese. Siamo di fronte a scelte di grande spessore e di valore strategico. Ciò di cui ha bisogno l'Italia è un nuovo compromesso sociale, basato sulla valorizzazione dei beni comuni: la sanità e la scuola sono beni comuni su cui dobbiamo fare investimenti strategici in grado di dare futuro La digitalizzazione e la lotta alle disuguaglianze: è su questo che si può fare un nuovo patto sociale, in cui le imprese, le forze intermedie, i sindacati, il Governo e la Repubblica italiana trovino obiettivi concreti per fare quel salto che diversamente non riusciremo a fare. È necessario andare avanti nella costruzione della nuova Europa. Abbiamo cominciato, l'Europa ha fatto cose importanti; adesso dobbiamo cambiare il Patto di stabilità, senza il quale non c'è un futuro. È importante la proposta di Draghi sugli eurobond per gli investimenti; è importante ridare un senso e una direzione di marcia

Ci sono troppi Paesi che non riescono a recuperare i vaccini e il piano fatto per quei Paesi non sta funzionando; occorre un salto di qualità e avere la capacità di guardare avanti. Infine, credo

a dare una risposta di qualità, se vogliamo costruire una speranza. Ho sentito - e concludo - che alcuni colleghi dicono che la scelta del Governo sulle riaperture è ideologica. No, colleghi: per governare

Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, non mi richiamo ai numeri del DEF, perché sono stati ampiamente trattati dai colleghi del mio Gruppo, i senatori Perosino, Damiani e Saccone e le

per sottolineare che ci accingiamo ad approvare un ulteriore indebitamento di 40 miliardi nel 2021 e un ulteriore di indebitamento medio di sei miliardi annui per il periodo 2022-2033, per finanziare perlopiù investimenti pubblici. Ora - mi riallaccio a quello che ha detto il senatore Errani - non sta a me qua richiamare la responsabilità delle dichiarazioni; però dobbiamo capirci tutti bene una volta per tutte. Siamo in una maggioranza e tutti abbiamo aderito senza indugio all'appello del Presidente della Repubblica, che ha richiamato tutti i partiti a un senso di responsabilità e a non mettere bandierine; non siamo però nemmeno in una gabbia dove non è consentito esprimersi. Quindi, nel dibattito politico accettate che ci possa essere anche qualcuno che dice quello che pensa, magari non perfettamente in linea. L'importante è andare avanti e guardare oltre. Da questo punto di vista, richiamiamo anche le parole del ministro Franco, che, preannunciando il provvedimento del DEF, ha detto che questo aveva un effetto *shock* sull'economia.

fatto presenti nel corso delle audizioni numerose che ci sono state in Commissione bilancio: abbattere i costi fissi, introdurre una fase di moratoria chiedere all'Europa una proroga del *temporary* *framework*. Se non riusciamo a portare a casa questi risultati, infatti, vano è il nostro parlare. vano è il nostro parlare. *(Applausi)*. Non si tratta qui di riaprire, perché farlo senza ripartire non serve assolutamente a niente. Le aziende, specialmente quelle più colpite, nel settore dei servizi, del turismo e della ristorazione,

perché - lo ripeto - vana è una riapertura, se non c'è una ripartenza. Su questo, dobbiamo permettere alle aziende, quelle piccole, che mantengono la struttura portante del nostro Paese a livello economico, di essere pronte a questa fase di rilancio e di rimbalzo, che sicuramente ci sarà.

miglior uomo che in questo momento possa degnamente e ottimamente rappresentare gli interessi degli italiani, specialmente nei confronti dell'Europa. *(Applausi)*. Possiamo dire tutto del professor Draghi. Ci sembra un uomo saggio, un uomo prudente. Sicuramente, nella sua saggezza e nella sua prudenza, sarà anche in grado di riprendere in mano alcune determinazioni che, allo stato attuale, in questo momento, sembrano necessarie. Non

il breve periodo. Dobbiamo traguardare il medio-lungo periodo per portarci fuori da queste secche. Si è parlato di debito buono.

Prendete in mano, signori del Governo, la questione del *voucher* per i lavori stagionali o dell'agricoltura. Sblocchiamo, in un certo qual senso, tutto quello che può favorire una ripresa effettiva e un rilancio del settore dei servizi. Non capisco perché si tardi a liberare queste energie, che ci sono. La produzione industriale italiana di questo primo trimestre è migliore di tante altre a livello europeo. Quindi, i nostri imprenditori, nonostante questa situazione, questa difficoltà e la carenza di liquidità, ancora confermano la validità del nostro sistema e della nostra struttura economica, specialmente nelle aree più sviluppate del Paese.

Abbiamo visto però che nell'ultimo anno gli italiani hanno fatto ricorso a una loro caratteristica principale, che è la parsimonia. Le giacenze medie nei conti correnti degli italiani non sono mai state alte. Chiaramente era tutto bloccato e chiuso, ma questo dimostra, ancora una volta, che se liberiamo queste energie, mettiamo in campo risorse e flussi ingenti di denari che vanno a favorire lo sviluppo e la ripresa.

se non ci sono freni e si tolgono i blocchi e i divieti vari, anche i servizi si riprendono immediatamente e rapidamente. bisogna mantenere vive le imprese per farle ripartire appena saranno tolti i vincoli. Servono sostegni finanziari immediati.

è un rischio che vale la pena assumerci, visti anche il rilevante ruolo e la vicinanza dell'istituzione europea. Non occorre che richiami puntualmente i singoli provvedimenti, come la moratoria dei prestiti, la proroga dei termini e i *voucher*, in quanto sono tutti argomenti che sappiamo essere all'attenzione dell'Esecutivo

d'arte italiane, vero patrimonio mondiale dal punto di vista storico, architettonico e culturale. Non lo dico per drammatizzare, ma non ce la fanno più.

con il decreto-legge di ieri), ma anche ottimismo. Noi di Forza Italia siamo ottimisti e abbiamo fiducia nell'Italia e negli italiani.

Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo alla proposta di risoluzione presentata e, quindi, al Documento di economia e finanza.

asprezze e battaglie ideologiche, anche se ciò naturalmente non significa rinunciare alla nostra identità (ribadisco che questo non ci è stato chiesto), né arrendersi al conformismo e, quindi, rinunciare a esercitare il diritto di critica. Infatti, se facessimo così, renderemmo il tutto di questa maggioranza inferiore alla somma delle sue parti. Nel motivare la mia dichiarazione di voto, vorrei muovere dal mio ultimo intervento in quest'Aula. In quell'occasione mi accadde di far notare che la richiesta che veniva fatta coralmente (ma credo, forse, in particolare alla forza politica in cui mi onoro di militare) di sostenere la prospettiva di un'Unione europea sempre più integrata e che sarebbe approdata a un bilancio unico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione, se rivolta specificamente a noi, era male indirizzata. Il problema rispetto a questa visione ideale, infatti, non era e non poteva essere una nostra preclusione ideologica, che non c'è e che, se ci fosse, sarebbe tutto sommato irrilevante nel grande disegno europeo, ma, viceversa, la strenua preclusione politica della Germania che da sempre si oppone a questo progetto di solidarietà. A tale preclusione credo sia difficile girare intorno. Non è una critica, ma un dato fattuale, quello che espongo. Questo dovrebbe essere ormai chiaro ma *pro futuro -* lo diventerà ancora di più quando la SPD perderà le prossime elezioni tedesche, dopo le quali peraltro anche il PPE non starà benissimo, ma non entriamo in queste tristi vicende. Ne consegue, però, una cosa che riguarda noi e il dibattito di oggi, cioè il fatto che non dovremmo razionalmente aspettarci di essere sostenuti nei periodi di recessione da altri che da noi stessi la valutazione del DEF, come in generale quella dell'orientamento di politica economica del Governo, va fatta alla luce di questo dato di fatto. Da quell'intervento sono passati tre mesi e sono stati fatti altri passi avanti (rilevanti, direi). Il 24 marzo 2021 abbiamo appreso che: «il coordinamento europeo va sempre cercato e va rafforzato, ma se non funziona in questi momenti dove il tempo è prezioso, occorre anche trovare le risposte da soli». Questa è una dichiarazione saggia, estremamente opportuna e tempestiva del signor Presidente del Consiglio, che peraltro viene incontro a una cosa che questa forza politica ha sempre affermato. *(Applausi)*. L'idea L'idea è che il coordinamento debba essere un mezzo e non un fine e il fatto di avere un primo Ministro che finalmente afferma quest'idea, che di per sé è lapalissiana, è rivoluzionario. È un'idea rivoluzionaria e liberale e un segno di buon senso: la ricerca del coordinamento non deve assorbire più risorse di quanto il coordinamento possa procurarne o liberarne, altrimenti si determina una inefficienza. Esiste evidentemente anche un rendimento di scala decrescente dell'integrazione politica. Ora, pur precisando che non è una critica a nessuno di noi, visto che siamo tutti qui e partecipiamo alla discussione perché accettiamo di operare all'interno di un contesto di regole date, la liturgia del semestre europeo, che oggi celebriamo con la stazione del DEF, a me non sembra un esempio particolarmente virtuoso. Non voglio annoiarvi con citazioni erudite dalla letteratura scientifica, ma personalmente continuo a pensare che questa rigida calendarizzazione di documenti programmatici e questo scrutinio europeo, che in circa un decennio non è riuscito di fatto ad aumentare la convergenza macroeconomica fra gli Stati membri, siano un esempio chiaro di coordinamento che assorbe o distrugge risorse, anziché liberarne. Lo è a mio avviso ancora oggi, ma naturalmente lo era ancora di più quando questa liturgia era il veicolo di quelle prescrizioni politiche irrazionali che un tempo tutti propugnavano e che oggi sono rimaste orfane, cioè quelle dell'austerità. Naturalmente però lealtà e senso delle istituzioni significano anche operare all'interno di regole la cui razionalità forse è dubbia, ma ci è facile farlo, perché vediamo che il mondo ci sta venendo incontro, a noi che abbiamo sempre detto quello che era nei libri di macroeconomia, e lo sta facendo con una rapidità impressionante, direi promettente. Sei giorni fa abbiamo appreso che la sostenibilità del debito pubblico non dipende più, come in passato, dall'andamento dei tassi di interesse che permettono di servire i costi della raccolta, ma dalle prospettive di crescita. Ecco, quest'affermazione, sempre del Presidente del Consiglio, è interessante, anche se tutto sommato mette in evidenza aspetti che finora, nel dibattito sulla dinamica e sulla sostenibilità del debito pubblico, erano stati sottaciuti: per esempio, il ruolo che l'esplosione del costo del debito, verificatasi all'inizio degli anni Ottanta, ha avuto nel determinare il raddoppio del rapporto debito-PIL in circa dieci anni. Eppure, non si tratta di enormi novità, da un punto di vista concettuale. Voglio fare una citazione: si spera che questo articolo abbia dimostrato che quello dell'onere del debito è essenzialmente il problema della crescita del reddito nazionale. Questa citazione viene da un articolo del 1944 di Evsej Domar, un economista keynesiano. Non abbiamo quindi fatto una grande scoperta, scoprendo che la crescita economica è fondamentale nel garantire la sostenibilità del debito. La domanda, in questo come in altri casi, è perché ora: nel 1944, che è anche l'anno della Conferenza di Bretton Woods (un altro dato storico che spesso viene evocato), si stava concludendo, come sappiamo, una guerra. È veramente triste constatare che, per arrendersi all'ovvio, gli esseri umani prima debbano combattersi tra loro o, come nel caso attuale, essere sopraffatti da catastrofi naturali che nel linguaggio corrente continuiamo a paragonare a un evento bellico: sono ad esso paragonabili non solo e non tanto nel tributo di vittime umane, cui deve andare il nostro ricordo, quanto nelle conseguenze economiche. Il debito oggi è a volumi postbellici; più esattamente, però, lo era anche prima della crisi pandemica. se, da un lato, non è strano che oggi si riscoprano le ragioni della crescita, come si scoprivano nel 1944, lo è che si sia aspettato fino ad oggi per affermare l'esigenza della crescita e che, per tanti anni, si sia continuato sulla strada dell'austerità.

il Covid-19 ha dato una ragionevole via di fuga ai nemici dell'ovvio, cioè agli amici dell'austerità, perché consente di dire che, siccome oggi è tutto diverso, allora finalmente si può fare quello che in realtà si sarebbe dovuto fare già da prima, però scordiamoci il passato e ci permettiamo di esprimere minime critiche, pur nel giudizio positivo che diamo all'intervento del Governo; infatti agli atti - a noi sembra che non venga compreso un dato che pure dovrebbe essere evidente. Ricordiamo il tempo in cui si rimproverava ai Governi di avere il pilota automatico e che i mercati li avrebbero costretti a procedere comunque sulla strada delle riforme, che poi erano i tagli (quelli che servivano a consegnare in mani private pezzi crescenti di stato sociale e di intermediazione del risparmio)? Esiste, però, un'eterogenesi dei fini, una nemesi: oggi è la Banca centrale europea ad avere il pilota automatico. Sono sempre i mercati a indurre questo regime e sono sempre loro, in qualche modo, gli artefici del pilota automatico, per il semplice motivo che, ove la BCE smettesse di sostenerli acquistando i titoli del debito pubblico, crollerebbero, il che,

finanza è il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica e ci restituisce un quadro chiaro e preciso degli interventi adottati nell'anno passato, primo anno terribile della pandemia, e uno di quelli che metteremo in campo nel 2021 e negli anni seguenti. I riferimenti e le cifre contenuti nel DEF sono incontrovertibili e consentirebbero a tutti di fare un'analisi obiettiva circa le politiche economiche di contrasto alla crisi messe in campo dal Governo Conte II, lungo tutto il 2020, e dal Governo Draghi, negli ultimi due mesi. Sono numeri, tabelle e dati che sono al di sopra della propaganda che alcuni fanno e continuano a fare sui *media* e sui *social*. Rivolgo quindi un appello a tutti: parliamo di fatti e cerchiamo di dare informazioni precise e fedeli ai cittadini. Nell'anno 2020 l'indebitamento aggiuntivo contratto dallo Stato per fronteggiare l'emergenza economica e sanitaria causata dalla pandemia, utilizzando risorse interne, quindi non provenienti dall'Europa, è stato di 108 miliardi

Agli enti territoriali ne sono andati 10,8; alla sanità 8,2; a tutto il capitolo delle politiche per la famiglia e le politiche sociali, che comprende anche il reddito di emergenza, ne sono andati 6,1; infine, alla scuola 2 miliardi. Quindi, nel 2020 il Governo Conte II ha destinato 64 miliardi su 108 alle imprese e agli operatori economici, a testimonianza di quanta attenzione ci sia stata per il comparto, al di là delle chiacchiere e delle menzogne propalate a piene propalate a piene mani negli ultimi mesi. A tutto questo si aggiunga che con il decreto-legge cura Italia del marzo 2020 e con il successivo decreto-legge liquidità abbiamo aperto lo spazio alla moratoria dei mutui per le imprese, che ancora oggi investe un valore di 158 miliardi.

garantiti dal Fondo per le piccole e medie imprese, per un totale di 155 miliardi, e da SACE per quelle più grandi, per un totale di 23 miliardi. Riassumendo, stiamo parlando di numeri molto grandi: 130 miliardi di scostamento nel 2020 (i 108 di cui ho parlato prima e i 22 di scostamento

Sono numeri freddi, che possono non dire niente, ma è importante il totale generale: facendo appunto il calcolo, dal 2020 al 2026, grazie al percorso che è stato delineato dal Governo Conte II e fisiologicamente ripreso tal quale dall'attuale Esecutivo senza alcuna discontinuità (checché se ne dica), il nostro Paese ha potuto e potrà mettere in campo risorse per quasi 450 miliardi Voglio sottolineare che ancora oggi le misure economiche che stiamo adottando seguono la filosofia di intervento e gli schemi adottati dal Governo Conte, al punto che gli stessi 40 miliardi dello scostamento di cui ci occupiamo oggi e che costituiscono la base finanziaria del decreto-legge sostegni-*bis* serviranno anche a prorogare tutte le suddette misure per la liquidità messe in campo dal precedente Esecutivo e che ha potenziato quelle soluzioni innovative che l'attuale Governo non può fare a meno di prorogare. Inoltre, tutte queste misure serviranno a dare respiro agli operatori economici messi in ginocchio da questa crisi e da questa pandemia. Se serviranno altre misure, le adotteremo senza alcun problema, perché nessuno dovrà mai essere lasciato indietro. Va tutto bene? Assolutamente no: sono ancora vaste le sacche di sofferenza causate dagli effetti economici della pandemia, tra l'altro, si aggiungono a problematiche di cui già il nostro Paese soffriva. Tanto ancora vogliamo e dobbiamo fare e noi del MoVimento 5 Stelle siamo in questo Governo proprio per continuare a mettere in campo provvedimenti che tutelino le vite dei cittadini e le attività economiche, che potenzino la sanità e la scuola pubbliche *(Applausi)*, che inneschino e fortifichino un modello di sviluppo che ponga al centro la persona, basato sulla sostenibilità, sul rispetto dell'ambiente, sull'economia circolare e sulla transizione ecologica. Proprio a tal proposito, ci siamo tanto battuti per l'istituzione del nuovo Ministero, quello della transizione ecologica, che ieri abbiamo approvato in via definitiva qui al Senato. Vogliamo un Paese più giusto, più solidale, più equo, più sicuro, più attrattivo e più stimolante per chi vuole fare impresa. Siamo al Governo, in una maggioranza composita - e non è semplice - proprio per continuare a progettare il Paese del futuro e per difendere le conquiste degli ultimi mesi. Ho sentito proprio ieri, in Commissione bilancio, un esponente dell'opposizione attaccare ancora una volta il reddito di cittadinanza e il *cashback*. Certamente ci vuole davvero coraggio a prendere queste posizioni e a farlo dopo un anno terribile, come quello della pandemia, e dopo la plastica dimostrazione dell'estrema efficacia di questa misura, che che ha consentito a tre milioni di nostri connazionali di non precipitare nell'abisso della disperazione, in un momento drammatico come quello causato dall'emergenza sanitaria. Signori detrattori, se non volete credere a noi o ai cittadini, almeno provate a leggere i documenti dell'OCSE, che nel rapporto intitolato «Going for growth» ha evidenziato, testualmente, che il reddito di cittadinanza è stato in grado di «migliorare radicalmente la rete di sicurezza sociale, introducendo maggiori benefici per le famiglie, insieme a condizioni più rigorose». *(Applausi)*. Tra l'altro, sempre l'OCSE ha lodato anche il taglio del cuneo fiscale che abbiamo fatto con il precedente Governo e il piano *cashless*,

di euro di gestione del contante, ovviamente nel lungo periodo. Signor Presidente, torno ai numeri di prima e al loro significato politico. Abbiamo messo in campo quasi 400 miliardi di euro di risorse fino al 2026, tra protezione sociale e investimenti, più altre centinaia di miliardi di euro di garanzie per la liquidità. È un risultato storico, un cambio di paradigma e un'occasione di sviluppo che il Paese attendeva da anni e che deve utilizzare al meglio, per creare lavoro e benessere. Ieri, in audizione, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che, anche grazie a queste misure, nel 2022 gli investimenti pubblici in valore assoluto torneranno finalmente al livello registrato -

Una giovane coppia: 31 euro di spesa di consumo e 184 euro di bolletta. Una famiglia: 213 euro di consumo e 474 di bolletta. Una parrucchiera: 106 euro di consumo e 351 di bolletta. Un *pub* chiuso: 264 euro di spese per l'energia e 892 di bolletta. Un'attività commerciale: 500 euro di gas naturale e 1.076 di bolletta. Un ristoratore: 4.800 euro di spese di energia 12.500 tra spese varie, tasse, oneri di sistema e quant'altro. Una palestra: 34 euro di consumo e 235 di bolletta. Ecco dove sono i problemi degli italiani, che non vedete, perché questo accade nel Paese vero. Invece, nel vostro Paese dei padroni, accade che si dovevano revocare le concessioni ai Benetton e invece partecipiamo, con i soldi degli italiani, ad un'asta con Abertis. Dov'è la sinistra, quella che con Speranza, D'Alema e Bersani governa con Draghi e con Giorgetti, che oggi non ha voluto sentirsi dire che la società pubblica Invitalia (Arcuri) è socia di ArcelorMittal, un padrone che licenzia un lavoratore colpevole di aver pubblicato un *post* che commentava favorevolmente una *fiction* televisiva

Draghi teme i fantasmi del suo passato? Profumo è ancora lì, amministratore delegato di Leonardo, una partecipata dello Stato quotata in Borsa. Lo sapete che MPS (sempre del MEF ha dovuto accantonare 400 milioni per le cause miliardarie in corso? Certo che lo sapete, Draghi lo sa! Voi state governando per il sistema, nel sistema. I vostri scostamenti, i vostri soldi fanno dei giri immensi e poi finiscono nelle tasche dei soliti. Votiamo no. Presidente, L'Alternativa c'è voterà contro al DEF perché prefigura un sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine eccessivamente rigoroso. Nondimeno, per responsabilità

per certificare i crediti d'imposta, quindi sostanzialmente creare una moneta fiscale, e impegnare il Governo nelle sedi opportune ad aprire la discussione per la revisione delle regole fiscali che sostengono il patto di stabilità e crescita. Ciò per evitare che la nuova applicazione del patto di stabilità comporti l'adozione di regole di rientro dal debito in modi e tempi non condivisi da tutti gli Stati che possano

comunque non è corretta, anche perché non ci consente la valutazione attraverso il PNRR. Voteremo invece a favore dello scostamento di bilancio, perché è giusto dare ossigeno alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini.

né il modello di sviluppo né i trattati dell'Unione europea. Abbiamo sostenuto il presidente del Parlamento europeo Sassoli quando ha fatto una proposta che l'Italia non ha accolto

impensabile, perché sarebbe stata una violazione del trattato europeo, come se questo fosse intoccabile. Il tema è delicato, di carattere economico (e io non sono un economista), ma soprattutto politico; della politica però ha una visione diversa ognuno di noi, mentre non è così per le questioni giuridiche, su cui mi vorrei soffermare, riguardando la carta di Sant'Agata dei Goti "Dichiarazione su usura e debito internazionale" del 1997, che è stata sottoscritta da un autorevole *pool* di studiosi provenienti da vari Paesi. Pur riconoscendo il sacrosanto principio per cui i debiti vanno onorati, essi fanno emergere nella dichiarazione quattro fondamentali principi di giustizia in tempi non sospetti, perché fuori dal pericolo e dalla situazione Covid: innanzitutto, la priorità del diritto alla vita; l'universale destinazione dei beni della terra; la fondamentale esigenza di equità, che non permette di assumere solo il profitto come criterio ultimo; e il fatto che vadano sempre prese in considerazione innanzitutto le esigenze dei più deboli. Muovendo da questi presupposti, la Dichiarazione enumera alcuni principi di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, che costituiscono la fonte dell'ordinamento internazionale, come prescritto dall'articolo 38, comma 1, dello statuto della Corte internazionale Ebbene, rispetto alla questione del debito contratto a seguito della grave pandemia in corso, si impone l'applicazione e il rispetto, oltre che del principio del diritto alla vita, di almeno altri due principi: principi: quello dell'autodeterminazione dei popoli e quello del *favor debitoris*. Sull'autodeterminazione dei popoli qualunque contratto non può essere siglato se una delle parti esercita un'ingerenza sulla debolezza dell'altra. Pertanto, la scrittura dei trattati non è...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

specificare che non ho fatto altro che riportare sotto forma di emendamento due osservazioni, votate favorevolmente dalla maggioranza parlamentare presente in Commissione finanze, che erano volte - come l'emendamento in questione - a implementare un'infrastruttura digitale che garantisca le certificazioni dei crediti d'imposta anche come mezzi di pagamento di beni e servizi (sostanzialmente introduca la strada per la moneta fiscale). L'altro capoverso aggiunto impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi opportune per affrontare la discussione di una revisione delle regole fiscali che sostengono il Patto di stabilità e crescita, per scongiurare il rischio che l'adozione di regole di rientro dal debito - in modi e tempi non condivisi da tutti gli Stati - possa ingenerare effetti prociclici a detrimento delle prospettive di crescita economica. Questo secondo capoverso è particolarmente rilevante;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

Signor Presidente, c'è una vicenda legata al nome del celebre tenore Enrico Caruso che in queste ore sta fortemente indignando gli animi nel mondo della lirica italiana e non solo, perché Caruso è stato e resta tenore tra i più grandi, amato in Italia e osannato all'estero. Quest'anno ricorre il primo centenario della sua morte e per l'organizzazione delle iniziative in ricordo è stato istituito dal Ministero della cultura un comitato nazionale per le celebrazioni. trasparente *iter* relativo alle nomine dei membri di tale comitato costituisca un danno al valore della memoria e si aggiunga alla beffa di un'allarmante e impunita ignoranza. È una pura operazione politica, quella orchestrata da Franceschini, che usa a proprio consumo la figura di un artista al quale dovremmo invece rispetto e cura della sua eredità. Innanzitutto, nell'elenco dei componenti del comitato c'è una "teoria" di nomi dovuti, ma è palese e sconcertante l'assenza dei testimoni di Caruso, cioè di chi per preparazione o per esperienza diretta ha davvero vissuto il tenore. Caruso non è forse nato a Napoli? Non è morto a Napoli? Non è legato alla località casertana di Piedimonte Matese, dove visse la sua famiglia, e a Sorrento, dove soggiornò prima di morire e dove esiste, nelle sale di un ristorante, l'originale museo che raccoglie cimeli, dischi originali, caricature? Al teatro San Carlo di Napoli, città che conserva le sue spoglie, oltre che al Metropolitan di New York, che ha visto sul palco le sue portentoso esibizioni? E allora perché, colleghi, nella lista non si legge alcun rappresentante di questi mondi carusiani, parte viva della storia umana e professionale del cantante? Il Ministro o pecca di analfabetismo musicale, ignorando chi sia Caruso, o di opportunismo politico, posizionando su poltrone strategiche e redditizie in termini di visibilità personaggi della propria corte, in quella che invece non è una monarchia, perché Enrico Caruso è patrimonio democraticamente universale. In entrambi i casi, il ministro si macchia di un reato grave contro la cultura del nostro Paese, anzi Caruso, definito "la voce dei due mondi", meriterebbe un comitato di respiro internazionale, che coinvolga quanti lo amano e lo conoscono. Il pronipote Federico ha scritto una lettera aperta ai responsabili per lamentare tutto ciò. D'altra parte, il direttore del giornale *on line* «Toscana Today» ha chiesto come la consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali abbia potuto assegnare 90.000 euro al Comitato per le celebrazioni di Caruso il 23 febbraio 2021 se quello ancora non esisteva. Insomma, parafrasando la celebre canzone di Lucio Dalla «Caruso», al Ministero della cultura certe prassi clientelari per nulla logiche e per nulla trasparenti sono diventate «una catena ormai che scioglie il sangue dint'e vene», ma per l'indignazione.

Quando pensi di avere potere sull'altro e lo perdi tutto ciò che ti resta da fare è pensare al potere sulla vita e la morte. è, purtroppo, la solita espressione della volontà di potenza dell'uomo sulla donna. Il mio intervento è rivolto a portare all'attenzione dell'Assemblea l'ennesimo caso di violenza contro una donna avvenuto nei giorni scorsi e conclusosi, purtroppo, con un epilogo più tragico. Si tratta di due miei concittadini di Sarno, nella provincia di Salerno, ma residenti a Marino, in provincia di Roma. Il marito, un carabiniere, si è tolto la vita dopo aver sparato più volte alla moglie, Annamaria. Lei era un'insegnante molto conosciuta e benvoluta nella comunità di Sarno, dove la notizia ha sconvolto i cittadini uniti nel dolore per l'accaduto. Annamaria era molto impegnata nel sociale e voglio ricordare anche il suo impegno civico e politico rivolto *in primis* alla difesa dei diritti delle donne. Le ricostruzioni giornalistiche parlano di un rapporto che, purtroppo, è sfociato nell'esito più drammatico, connotato, da parte del marito, da gelosia, pedinamenti e continui controlli al cellulare. Tale comportamento è frequente nei casi di violenza contro le donne e spesso anticipatorio di conseguenze fatali. Per questo la massima attenzione va data ai cosiddetti reati spia. Le istituzioni sono continuamente al lavoro per tentare di contrastare l'accadimento di episodi come quello di cui è stata vittima Annamaria. Da una relazione che abbiamo approvato ultimamente in Commissione femminicidio emerge come la diffusione della violenza contro le donne rappresenti nel decennio 2008-2018 una vera e propria strage con ben oltre 1.600 uccisioni. Oggi ci troviamo costretti ad aggiornare i dati sul femminicidio: nel corso di quest'anno, a causa della pandemia, si sono registrati numerosi aumenti. Ci troviamo di fronte a un fenomeno che non è più un'emergenza occasionale, né un fatto privato, ma una tragedia sociale e cronica ormai strutturale, che sta travolgendo la nostra società civile. Senza una vera e propria trasformazione culturale che parta dalle scuole e che permetta di superare gli stereotipi promuovendo la diffusione di atteggiamenti e linguaggi rispettosi di identità e differenza di genere, questa battaglia non potrà essere vinta. La sfida reale è promuovere una profonda trasformazione culturale che investa la società partendo dalle basi (scuola e famiglia) e che sappia coinvolgere ogni aspetto della vita relazionale. Insegnare alle giovani alle giovani generazioni la parità dei diritti e il rispetto dell'identità di genere rappresenta un obiettivo imprescindibile per deviare il percorso... (*Il microfono Signor Presidente, il sistema delle banche sta attraversando già da qualche decennio una profonda trasformazione individuabile nel processo di concentrazione che stanno perseguendo, dettato principalmente dall'introduzione delle grandi innovazioni dell'era digitale, dall'esigenza di maggiore competitività con i grandi gruppi internazionali e da qui nasce la necessità di un netto taglio alle spese. Tutto ciò produce l'effetto inesorabile della riduzione degli sportelli e, di conseguenza, toccherà inevitabilmente il posto di lavoro di migliaia di dipendenti, su cui bisogna urgentemente predisporre un piano di reintegro. Il 29 dicembre scorso BPM ha annunciato la chiusura di 300 filiali nel corso del primo semestre del 2021. Tra queste troviamo anche quelle filiali che nelle piccole località rappresentano un importante riferimento per la permanenza delle già poche attività esistenti. Motivo in più, per questi piccoli insediamenti, di andare verso un inesorabile spopolamento, cui la politica nazionale e locale ha il compito e il dovere di dare soluzioni tangibili e urgenti. Così ad Accadia, piccolo centro dei Monti Dauni in provincia di Foggia, che, come tanti che seguono la stessa sorte, meriterebbe grande attenzione e sviluppo per la sua storia e le sue bellezze paesaggistiche, ma che invece vede ora chiudere la sua unica banca con cui lo stesso Comune ha sempre intrattenuto rapporti di tesoreria. solo significa spegnere poco alla volta le residue speranze di ripopolamento di queste aree, ma rappresenta anche un colpo alla permanenza di coloro che, amando la propria terra, resistono e sperano in un futuro migliore. Un ruolo sociale che verrà a mancare anche per quei clienti di maggiore fragilità, quali gli anziani, che avrebbero notevoli disagi a recarsi presso i Comuni vicini. Vorrei rivolgere un appello al Ministro dell'economia e delle finanze, affinché si adoperi per questi piccoli Comuni nel garantire loro almeno una filiale come servizio alla cittadinanza, già fortemente penalizzata e verso cui tutti dobbiamo compiere ogni sforzo, consapevoli del grande valore che rappresentano.

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per esprimere, a nome mio, del Gruppo di cui mi onoro di far parte Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e - mi voglio augurare - di tutta l'Aula, il pieno sdegno nei confronti delle gravissime insinuazioni che il sottosegretario alla giustizia Macina ha proferito nei confronti di Giulia Bongiorno e di Matteo Salvini di Giulia Bongiorno e di Matteo Salvini *(Applausi)*, ai quali va tutta la nostra solidarietà, in quanto persone correttissime, tanto nella vita quanto nel lavoro. Noi siamo qui, Presidente, richiamati a un elevato atto di responsabilità, a un elevato senso delle istituzioni, per tirare fuori l'Italia da questa difficoltà e da questa pandemia. purtroppo ci ritroviamo il Sottosegretario, in perfetto stile grillino, a tirar fuori ancora una volta la storia del complotto e la storia delle insinuazioni. comprensibile e soprattutto non è rispettoso nei confronti del presidente Mattarella e del presidente Draghi. A maggior ragione, questo attacco diventa del tutto incomprensibile quando ci ricordiamo che il problema del problema ce l'hanno a casa loro e si chiama Beppe Grillo. *(Applausi)*. Mi sarei aspettato che una donna, nonché Sottosegretario alla giustizia, avrebbe proferito alcune parole nei confronti di Beppe Grillo, che in un suo video scandaloso è stato in grado di dileggiare una ragazza e la sua famiglia, di offendere tutte le donne e di calpestare secoli e secoli di civiltà giuridica. *(Applausi)*. Tutto questo non è bastato a distrarre la sottosegretaria Macina alla giustizia. Tra l'altro aggiungo, Presidente, che Beppe Grillo, nell'ottimo stile che lo contraddistingue, cioè quello di un *clown*, riesce a essere forcaiolo alla bisogna, quando lui non c'entra, e garantista quando invece lui c'entra. Basta con questa cultura del sospetto, basta con questa cultura che

del senatore Pepe, che ha parlato testé. È oggettivamente sconcertante vedere quel che è accaduto oggi, con il rilascio di quell'intervista da parte dell'onorevole Macina, parlamentare sottosegretario alla giustizia. È una vergogna che un Sottosegretario alla giustizia approfitti del suo ruolo per mettere in campo quegli argomenti, soprattutto donna, che è la cosa peggiore e davvero più sconcertante: soprattutto donna! Devo dire, però, che lo sconcerto aumenta se si tiene presente che è anche un avvocato, che dovrebbe conoscere il meccanismo dei procedimenti penali. Quelle parole lasciano ovviamente allibiti chi conosce quei meccanismi e sa perfettamente che il comportamento della magistratura non si mette in discussione solo per un atto di piaggeria nei confronti del capo. Il capo ha sbagliato. Sarebbe stato più logico chiedere scusa, senza stare lì ad aggiungere niente. Invece, ha voluto richiedere il sostegno e il sottosegretario Macina si è ovviamente affrettata a dare quell'aiuto che era stato richiesto.

È sconcertante questo atteggiamento, così come il liquidare così sbrigativamente un attacco che è stato fatto alle istituzioni, alla magistratura. Quella magistratura che in tante circostanze ha voluto difendere, ha voluto in qualche maniera elogiare, quando fa comodo come è stato ben detto. È un atteggiamento a doppio binario: quando fa comodo, si diventa giustizialisti; quando fa comodo, si diventa garantisti a difesa di qualcuno, introducendo argomenti che non c'entrano nulla. E soprattutto, si attaccano le persone che sono state vittime di questi attacchi e che sono state poste alla gogna mediatica (cosa di cui ho parlato anche nell'intervento dell'altro giorno qui in Aula). Si attaccano quelle persone che, invece, hanno sempre chiesto che i processi non si svolgano in Parlamento. Quelle stesse persone che erano state attaccate, in maniera così

usi il suo ruolo, per di più essendo avvocato e dunque dovendo conoscere la materia, per attaccare una senatrice della Repubblica, nonché avvocato, facendo gravissime insinuazioni sulla sua correttezza di avvocato, è veramente una cosa intollerabile

di esecrazione e una correzione. Non è possibile e non è accettabile una cosa di questo genere. Il Ministero della giustizia deve assicurare il buon funzionamento della giustizia, non fare insinuazioni contro l'avvocato che ha il torto di difendere una ragazza che

Signor Presidente, io cambio argomento e mi rivolgo a lei e a quest'Assemblea per informarla che a Palermo è stata scoperta l'ennesima residenza *lager*, dove dipendenti insultavano e prendevano a botte e calci i disabili affidati alle loro cure. Ci sono stati degli arresti, grazie al lavoro dei carabinieri della stazione di Palermo Brancaccio, che ringrazio di cuore. Ovviamente, tutto è emerso grazie alle riprese delle telecamere, che hanno registrato maltrattamenti sistematici e vessazioni continue, spintoni, urla e insulti nei confronti di questi pazienti affetti da paralisi spastica. Un vero e proprio inferno, signor Presidente. Nel video si vede un operatore che prende la testa di un paziente e la sbatte violentemente contro un muro; un altro paziente trascinato per terra, tirato per i capelli; un operatore che tira una sedia a rotelle contro un disabile. vi invito a visionare questi video per rendervi conto dell'orrore di ciò che vi sto raccontando, perché davvero le parole non possono spiegare la rabbia, la sofferenza e la pena che si prova nel vedere queste immagini. Signor Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi di tutti gli schieramenti e dico: ma davvero il Parlamento vuole continuare a far finta di nulla? Dal 2009, per tre legislature consecutive, compresa questa, ho presentato una proposta di legge per l'introduzione delle telecamere in asili nido e strutture che ospitano anziani e disabili. La proposta è sempre arrivata a un passo dall'approvazione, per poi arenarsi e cadere nel dimenticatoio. Mi chiedo e vi chiedo: perché? Cosa stiamo aspettando? E non mi si venga a parlare di tutela della *privacy*, perché di fronte a comportamenti così disumani e violenti nei confronti di soggetti deboli e indifesi non c'è *privacy* che tenga. Mi

Grazie,